2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge recante: «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale».

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme in principio di materie di intelligenza artificiale. Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024. Il provvedimento, composto da 26 articoli distinti in sei capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

preliminare, rispetto alla discussione del G7, esattamente legata a questo punto. Siccome stiamo discutendo di un punto che potrebbe essere oggetto di una deliberazione in sede di G7 e poiché è una materia estremamente delicata e complessa, che ha bisogno, prima che si passi all'articolato, di una discussione in sede parlamentare, mi permetto di rivolgere un appello alla Presidenza e altri anche agli altri Gruppi. Chiediamo di poter calendarizzare, nella seconda metà di giugno, una sessione di dibattito con mozioni dedicata al tema dell'intelligenza artificiale e ai relativi provvedimenti da adottare.

quanto detto adesso dal presidente Borghi, cioè quanto sia importante che l'Assemblea si occupi di un tema che ha un'incidenza enorme sul futuro, sul mondo del lavoro, sul mondo dell'impresa, sulle amministrazioni centrali e periferiche e quindi sulla vita dei cittadini. Io non credo si possa pensare di arrivare ad una posizione del Paese, che sarà espressa, ovviamente, dal Governo in sede di G7,

complessiva. Pertanto, anche il MoVimento 5 Stelle chiede, come fatto in Conferenza dei Capigruppo, che si calendarizzi con l'urgenza necessaria, in considerazione dei tempi del G7, una sessione dedicata al tema dell'intelligenza artificiale.

successivo intervento del presidente Patuanelli mettono in evidenza l'atteggiamento contraddittorio della stessa Presidenza. La prego di informare il presidente La Russa in merito. Oggi la Presidenza informa l'Assemblea del collegamento del disegno di legge quando da giorni chiediamo che essa non sia più ostaggio di questa ossessione dei pieni poteri che la Presidente del Consiglio chiede, costringendo la maggioranza a questo tipo di sedute.

ci si dice che non è arrivato il momento, ma il momento oggi arriva semplicemente perché noi, al termine della giornata, prevista dal vecchio calendario con termine alle ore 20, non abbiamo altro all'ordine del giorno. Immagino che tutte le colleghe e tutti i colleghi vogliano partecipare domani alla commemorazione di Giacomo Matteotti alla presenza del Capo dello Stato. Immagino vogliano esserci tutti, anche se alcuni non hanno proprio nel cuore questa commemorazione

però che il calendario che avevamo previsto oltre una settimana fa è finito. Chiediamo anche, come abbiamo già detto ieri, di rivedere

agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***

sul modo di procedere dei lavori, rinnovandole la richiesta che abbiamo già fatto nei giorni precedenti, di conoscere in anticipo quali sono gli emendamenti che la Presidenza ritiene di non mettere in votazione perché decide di applicare il cosiddetto canguro. come senatori chiamati ad argomentare gli emendamenti presentati, abbiamo almeno il diritto di sapere qualche minuto prima quali saranno i testi messi in votazione. Abbiamo Abbiamo naturalmente contestato l'applicazione del canguro. Noi riteniamo che, in una discussione sulla Costituzione, in una discussione sulla riforma del nostro modello di democrazia, il canguro non dovrebbe assolutamente trovare applicazione.

di trasmettere a tutti i senatori presenti in quest'Aula l'ordine dei lavori, il che significa in sostanza conoscere uno per uno gli emendamenti che verranno "cangurati" e quindi non sarà possibile trattare specificamente con illustrazione, dichiarazione di voto e con un pronunciamento libero e consapevole. Ripeto: è una richiesta che è tanto più solida in quanto la materia trattata è la riforma costituzionale e, soprattutto, in quanto si è anche deciso il contingentamento dei tempi. Quindi, le chiedo per cortesia almeno di conoscere questo aspetto. Sospendiamo i lavori, la Presidenza si prenda mezz'ora di tempo, ma almeno ci trasmetta tutte le informazioni per poter esprimere il nostro voto con consapevolezza.

che nel dibattito di ieri sera qualcuno abbia potuto dire, a proposito dei nostri interventi, che è la solita paginetta trita e ritrita che ognuno ripete. Mi pare che quello che stiamo ripetendo, intervenendo sui diversi articoli, è l'allarme rispetto a una riforma che davvero mette in discussione l'architettura costituzionale. Non è un tema secondario, non è un tema semplicemente di logica di opposizione, ma riguarda il nostro ruolo, il ruolo di quest'Assemblea e il ruolo del Presidente della Repubblica. C'è una rigidità che questa riforma e questo articolo in particolare introduce rispetto alla possibilità

In gioco, appunto, c'è il ruolo del Parlamento e tutti gli emendamenti di cui sono prima firmataria, ma anche gli altri del nostro Gruppo, sono tesi a dare maggiore valore e potere al Parlamento dentro la gestione delle crisi e con esso al Presidente della Repubblica. Infatti, qui c'è un rovesciamento: passiamo dalla sovranità popolare al popolo del sovrano e al Parlamento del sovrano *(Applausi)*, nella migliore delle tradizioni autoritarie che fanno parte, ahimè, anche della cultura della destra di questo Paese. Un Parlamento trascinato, infatti, sarà un organo operativo che deve solo applicare l'indirizzo del Governo, tant'è vero che la maggioranza ci continua a ripetere che questa riforma era nel loro programma (anche se non era così) e, siccome era nel loro programma, la dovremmo per questo accettare perché hanno vinto le elezioni, volendo già nel metodo applicare la riforma che hanno disegnato. Quindi, non ci sarebbe più pluralismo e le maggioranze qualificate avrebbero meno senso. Non a caso, la Costituzione prevede il *referendum* popolare su queste riforme, perché sono garanzie di tutela della volontà popolare, non ostacoli al Governo. il ruolo del Parlamento e affiancano ai Presidenti delle due Camere anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari, consultati dal Presidente della Repubblica nella gestione delle crisi. Vorrei infatti tornare a ricordare il tema è che il suffragio universale e la volontà popolare si esplicano, si organizzano, si mettono in pratica attraverso le organizzazioni politiche (articolo 49 della Costituzione), tramite le quali i cittadini e le cittadine concorrono a determinare

nessuna possibilità di parlamentarizzare le crisi di Governo: è questo il *vulnus* fortissimo che riguarda il nostro ruolo. Io continuo a a ricordarlo rispetto a ciò che questa proposta ci pone. Davvero il Parlamento può essere solo un organo esecutivo della volontà della maggioranza? Una volta che una maggioranza viene meno ed entra in crisi, non è davvero possibile, dentro il pluralismo delle forze politiche che rappresentano la volontà popolare, trovare una via di uscita? Questa è la fine della democrazia rappresentativa e l'articolo 3 segna fino in fondo questo attacco alla democrazia rappresentativa.

Signora Presidente, l'obiettivo degli emendamenti a mia firma è quello di salvaguardare la funzione e le prerogative del Presidente della Repubblica, che sono il vero agnello sacrificale dell'impianto

d'elezione che dalla settima votazione in poi permetterà al Presidente del Consiglio, forte del premio di maggioranza, di scegliersi da solo il Presidente della Repubblica. poi l'articolo 3, che ha una funzione di raccordo rispetto a quello che colpisce la prerogativa più importante del Colle, ossia il potere di scioglimento delle Camere. Si intacca in questo modo lo strumento chiave, quello che consente al Presidente della Repubblica di esercitare la sua funzione di *moral suasion* sulle forze politiche, di essere motore di riserva del sistema, una volta che quello principale si è inceppato. Il Presidente è chiamato a svolgere una mera funzione notarile rispetto a un'eventuale crisi politica, in cui il pallino è soltanto nelle mani del Presidente del Consiglio. È lui che ha il potere di scioglimento delle Camere e non vale, come è stato detto, l'esempio del Regno Unito, della Svezia, della Spagna, perché gli unici Paesi in cui viene riconosciuta al Primo Ministro questa facoltà sono le monarchie e se al Re venisse attribuita tale facoltà, non ci troveremmo più in un regime democratico, ma in uno Stato dai tratti dispotici e assolutistici. Lo spostamento di questo potere dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio avrà come unica conseguenza la perdita di autonomia da parte delle Camere, la loro più totale subalternità alle determinazioni dell'Esecutivo. In situazioni di crisi o di attrito tra il Governo e la sua maggioranza, basterà al Primo Ministro agitare lo spettro dello scioglimento delle Camere per mettere fine alle istanze parlamentari. Noi pensiamo che per aumentare la stabilità del sistema sia sufficiente introdurre il meccanismo della sfiducia costruttiva: si può mandare a casa un Governo a patto che il Parlamento, in simultanea, sia in grado di indicarne uno nuovo. Al riguardo è molto interessante conoscere l'esperienza tedesca: si è ricorso alla sfiducia costruttiva solo due volte, nel 1972 nel 1982. Nel 1969, dopo tre anni di grande coalizione tra CDU e SPD, si formò una maggioranza tra socialdemocratici e liberali che elessero il cancelliere socialdemocratico Willy Brandt. Tre anni dopo, nel 1972, la CDU provò a rovesciare Brandt con un voto di sfiducia costruttiva e fallì per soli due voti. Dieci anni dopo, Helmut Kohl riuscì a prendere il posto del cancelliere in carica i liberali, che si trovavano in maggioranza con i socialdemocratici, votarono la sfiducia costruttiva insieme ai cristianodemocratici ed elessero Helmut Kohl. Pochi mesi dopo, però, ci furono le elezioni anticipate perché la nuova coalizione di Governo potesse essere convalidata da un voto popolare. Vinse effettivamente la coalizione tra cristianodemocratici e liberali, ma questi ultimi persero quasi un terzo dei voti. Cosa significa questo? Significa che la sfiducia costruttiva richiede una coesione, una compattezza, ossia una forte presa di responsabilità da parte del Parlamento. Quando questa non c'è stata, ha semplicemente rafforzato i Governi, quindi è stata a tutti gli effetti un elemento di stabilizzazione del sistema. sistema. Lo ripetiamo ancora una volta: perché non si è cercata questa strada semplice su cui le opposizioni avrebbero potuto convergere? Perché questa volontà di trasformare anche la natura del Presidente della Repubblica da garante dell'unità del Paese a figura espressione di una parte politica con meri compiti di ratifica della volontà di quest'ultima? Perché avete della democrazia un'idea da scontro muscolare e quindi tutte le figure terze di garanzia, a partire dalla più importante, sono un ostacolo o una minaccia. State aumentando la potenza del motore, state togliendo alla macchina freni e cinture di sicurezza e non è possibile che non ve ne rendiate conto.

secondo la quale questa riforma costituzionale non toccherebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, sia totalmente priva di fondamento.

questa riforma, ritengono eccessivi i poteri del Presidente della Repubblica e quindi, in qualche modo, proporre una riforma costituzionale che li limita e che sbilancia il potere dal Presidente della Repubblica al nuovo Presidente del Consiglio eletto. Perlomeno, si farebbe un'operazione di chiarezza, senza invece, come si sta facendo nel corso di queste settimane, richiamare un argomento che non ha un fondamento. Mi dispiace dirlo per l'ennesima volta, ma non si può, nel momento in cui si mette in campo un'ipotesi di riforma costituzionale che limita i poteri del Presidente, innanzitutto su due punti decisivi

vale per la formazione del Governo e vale in realtà - lo abbiamo visto nel corso della giornata di ieri e nei giorni precedenti esaminando l'articolo 1 - per la nomina dei senatori a vita, anche quello, evidentemente, un classico potere presidenziale. Vale però ancora di più per il tema dello scioglimento delle Camere. È chiaro che si fa una scelta di campo: si immagina un sistema politico nel quale la centralità del sistema viene spostata. Mentre oggi la centralità del sistema politico risiede in questo Parlamento e nella facoltà del Presidente della Repubblica

Ancora una volta viene raccontato un inganno; non c'è niente da fare e voi la potete raccontare come volete. Potete raccontare che l'elezione diretta porterà beneficio alla partecipazione popolare - davvero potete dire quello che volete ma i freddi numeri cantano. Domenica scorsa ha votato un piccolo Comune del Nord Italia, una bella cittadina del Nord Italia che si chiama Rovereto.

Lo capite che siamo dinanzi a un crollo del sistema democratico così come l'abbiamo conosciuto? Lo capite che abbiamo dinanzi a noi un problema gigantesco, cioè che mezzo Paese non va più a votare, considera la politica un corpo totalmente estraneo e che questa cosa paradossalmente succede maggiormente quando c'è il meccanismo dell'elezione diretta? Lo capite che, dinanzi a questo problema macroscopico che interroga la qualità della democrazia italiana, le scorciatoie non servono a niente, mentre servirebbe invece un ragionamento serio e articolato su come ricostruire un campo, su come ricostruire un sistema dei partiti, su come ricostruire un equilibrio politico? Lo capite che le scorciatoie non servono? Possibile mai che un dato clamoroso come questo, che dovrebbe vedere questo Parlamento ossessionato dalla ricerca di un qualche rimedio, venga totalmente espulso dalla discussione? Che cosa deve succedere Deve succedere davvero come nell'Ottocento, ossia che vadano a votare solo coloro il cui reddito parte da una certa percentuale in poi e tutto il resto della popolazione non vota? Credo che, dinanzi a un tema macroscopico come questo, questo, la scorciatoia che si sta cercando sia un danno esiziale per la democrazia di questo Paese e mi piacerebbe discutere di questo piuttosto che delle scorciatoie di cui stiamo parlando.

Abbiamo esaminato i primi due articoli, stiamo esaminando il terzo. Il primo articolo toglie uno dei poteri del Presidente della Repubblica; il secondo fa finta di dargli importanza, modificando le modalità di nomina; il terzo torna ad incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, perché va a modificare l'articolo 88, che parla di un potere fondamentale del Presidente della Repubblica: è il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere. Ma voi dovete modificare l'articolo 88 della Costituzione, e lo dovete modificare perché adesso il potere principale di sciogliere le Camere lo dovete dare al Presidente del Consiglio eletto. Sta emergendo sempre di più e si sta delineando sempre di più quella realtà che voi state nascondendo attraverso la vostra campagna elettorale e i vostri slogan, che tutto dicono meno quello in cui consiste questa riforma.

magica "atto dovuto" e la funzione notarile di un Presidente della Repubblica che aveva una norma specifica, che gli dava un potere e lo delimitava anche in ambiti temporali; ora no: si contempla l'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica non ha voce in capitolo. E guardate che c'è una retorica manipolatoria e mistificatrice che emerge anche da come avete scritto questa riforma, perché poi ci arriveremo all'articolo 7, in cui in maniera politicamente ipocrita,

al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Peccato però che nello stesso articolo obblighiate il Presidente della Repubblica a rispondere e a sciogliere le Camere.

che possano volere questa concentrazione del potere né i colleghi della Lega, che difatti vogliono spingere verso una direzione opposta, quella dell'autonomia,

ma mi sorprende che tutta la maggioranza si voglia mostrare compatta rispetto a un programma che è diventato sempre più chiaramente funzionale a tenerla insieme non tanto per una comunione di intenti, ma per uno scambio reciproco di concessioni.

le imprese che vogliono stabilità dovranno affidarsi agli umori di una persona sola al potere, che il giorno dopo potrebbe decidere senza un perimetro di dimettersi, sciogliere le Camere e far tornare tutti al voto? In questa maniera state peggiorando la stabilità e consegnando il Paese e la sua stabilità agli umori di una sola persona.

con i contenuti dell'articolo 7 di questo disegno di legge. Confermano questa lettura incrociata le questioni che sono state dette in quest'Aula ieri nell'intervento del senatore Renzi circa l'insostenibilità, dal punto di vista giuridico, di questa proposta di premierato che, come tale, si manifesta incoerente rispetto a un principio elementare, che i giuristi chiamano del *simul simul*: nel momento in cui vi è l'indicazione diretta da parte dell'elettorato di un mandato nei confronti del capo di un Esecutivo e di un organismo legislativo, venendo meno il potere del Capo dell'Esecutivo, automaticamente decade l'intero impianto. E così laddove esistono dei meccanismi di elezione diretta coerenti e ordinati in cui, nel momento in cui il Parlamento o, nel caso specifico (esistono già dei casi nel nostro Paese), i sindaci, i Presidenti di Regione i Consigli comunali o regionali dovessero sfiduciare il capo dell'Esecutivo, si torna inevitabilmente alle elezioni. In questo caso, invece, per motivi tutti interni alle contraddizioni della maggioranza, non è presente questo principio elementare che - ripeto - ci avrebbe visti favorevoli. Ed è esattamente in questa direzione che andava la proposta di legge che abbiamo depositato e che è abbinata al testo in esame, la quale non è stata presa in considerazione per insipienza politica da parte del Governo, per infilarsi dentro questa contraddizione nella quale noi non abbiamo, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttamente eletto, il naturale ritorno al corpo elettorale. Infatti - leggo testualmente - in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Quindi, già qui viene meno l'attuale facoltà del Presidente della Repubblica. È poi il comma successivo quello che ulteriormente incastra l'intera vicenda: qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente e decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Insomma, qui si sdogana il diritto di fronda: c'è la possibilità costituzionale per un parlamentare eletto in collegamento al Presidente del Consiglio di organizzare la fronda nei confronti del Presidente del Consiglio eletto. Il Presidente della Repubblica viene trasformato in silente spettatore di questo gioco di Palazzo.

o si ha il coraggio e la volontà di andare fino in fondo e stabilire che c'è un nesso causale diretto tra il voto del popolo e l'esercizio del potere, oppure si fa rientrare dalla finestra quello che voi avete dichiarato che sarebbe uscito dalla porta, cioè i giochi di Palazzo, gli accordicchi, i trasformismi e gli equilibrismi parlamentari. Tutto questo è uno dei motivi per i quali

questo articolo, sul quale abbiamo presentato degli emendamenti, tra cui un soppressivo del comma 2, sono un po' la prova provata, la prova del nove, della natura ambigua, poco chiara e instabile di questo disegno riformatore. Abbiamo sempre detto sin dall'inizio di questo processo di riforma costituzionale che noi ci siamo e pensiamo che una riforma costituzionale vada fatta e anche presto. Non ci convince chi dice meglio niente che questa riforma perché, a furia di meglio niente, sono passati undici anni da quando Giorgio Napolitano, appena rieletto, ci diede uno uno schiaffo in faccia, ricordandoci che le istituzioni non stavano funzionando e chiedendo un impegno solenne all'intera classe politica, che lo applaudiva a scena aperta, di

Si pensi alla sciaguratissima riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, l'unica riforma che è passata e che non aveva nessun criterio dietro, se non un becero populismo al quale tutti ci siamo piegati colpevolmente per evitare guai peggiori. Noi pensiamo che la riforma vada fatta; ma va fatta una riforma chiara. Allora, o noi lasciamo che il capo dell'Esecutivo (sia il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica) venga eletto dal popolo, oppure diciamo che non è così. In questa riforma non si capisce. capisce. Quando diciamo che il Presidente della Repubblica può, in alcuni casi, nominare per una sola volta un altro parlamentare,

diventa il capo dello Stato. Pensi, signora Presidente, che Gerald Ford, quando diventò Presidente degli Stati Uniti, era addirittura sfuggito all'elezione, perché il meccanismo prevede che il Vice Presidente sia scelto dal Presidente; tanta è la vicinanza e la comunanza, che agli elettori è chiesto di votare per un *ticket*. Quindi io voto, per esempio, Biden-Harris, perché, nel caso in cui il presidente Biden non arrivasse alla fine del mandato,

non è più il popolo ad averlo scelto; tranne appunto il caso Ford, che è veramente un caso che è passato alla storia, normalmente dovrebbe essere così. Allora, quello che noi diciamo è che la la legislatura dura quanto il Presidente del Consiglio eletto, perché abbiamo deciso che sia il popolo ad eleggerlo. Vogliamo avere un numero due in caso di morte? Allora deve essere eletto anche lui, deve essere previsto dalla legge. Altrimenti dobbiamo decidere che il Presidente della Repubblica è lui che, in una Repubblica parlamentare, decide quando sciogliere le Camere. Questo ibrido non sta in piedi, perché l'elettore ha tutto il diritto di dire: ma, scusate, non avevate detto che dovevo sceglierlo io il Presidente del Consiglio? Adesso mi trovo questo signore o questa è esattamente la situazione nella quale ci troviamo oggi. Se vogliamo fare che il Presidente del Consiglio è scelto dalla maggioranza parlamentare, teniamoci la Costituzione così com'è. Se invece vogliamo passare vogliamo passare a un sistema presidenziale o semipresidenziale, allora facciamolo bene. Ha ragione Renzi a dire: che stiamo facendo? Volete fare il semipresidenzialismo? Prendiamo il modello francese (tutte le parti di questo Parlamento, prima o poi, hanno detto che gli andava bene) e diamo una Costituzione nuova, ma ben fatta, a questo povero Paese.

affermare dal presidente Balboni che questa è una "riforma selettiva", quasi a sdrammatizzarne la portata. Signor Presidente, colleghi, questo è un inganno. Noi abbiamo il dovere di dire, all'Aula ed all'opinione pubblica, che questo disegno di legge, altro che essere fintamente selettivo! Colpisce proprio il cuore della nostra Costituzione, scardina il fondamento della nostra Costituzione, che è il sistema parlamentare. La destra sta tentando una spallata per modificare la natura della nostra democrazia e trasformarla in un regime autoritario. Questo è! E questo noi denunciamo! *(Applausi)*. È un tentativo di rottura netta

di presidenzialismo, ma perché è un presidenzialismo senza contrappesi, che annulla il bilanciamento dei poteri, che annulla le garanzie, che sono fondamentali in democrazia. Non c'è niente di nuovo in questa che la la destra e la presidente Meloni chiamano riforma. In realtà è una regressione, un ritorno indietro ad un tempo vecchio, vecchissimo, dove solo uno comanda e tutto il resto non conta. La discussione degli emendamenti su questi articoli fa cadere tutta l'ipocrisia di una retorica insistita, portata avanti dalle forze della una retorica di bugie che sono spudorate. La prima bugia spudorata è quella secondo cui questa riforma non toccherà in alcun modo i poteri del Capo dello Stato: stiamo vedendo quanto sia falso! Il Presidente della Repubblica perde la sua funzione cardine, che è la facoltà di sciogliere le Camere. Oggi quel potere è del Capo dello Stato, in funzione della sovranità del Parlamento; domani non più. In caso di dimissioni o sfiducia del *Premier*, il Parlamento decreta il suo auto scioglimento, che è automatico e non più prerogativa del Presidente della Repubblica. Egli, perdendo questo potere, perde, di fatto, tutti gli altri. Per questo la vostra è una bugia spudorata. Il Presidente della Repubblica non avrà più autonomia, ma sarà ostaggio del Capo del Governo, che è il *dominus* della maggioranza parlamentare e di tutto il sistema. La seconda bugia: la destra afferma che la legge elettorale non sarà una legge truffa. Poi, però, inserisce addirittura in Costituzione un premio di maggioranza attribuito sempre. Quindi, non è vero

più uno dei voti si potrebbe avere il 50 per cento più uno dei parlamentari e questa sarebbe una truffa mostruosa.

con il clima di continue provocazioni, al limite del bullismo, portate avanti dagli esponenti della maggioranza.

ne siete capaci. Voi dite: dobbiamo fare questa riforma perché è nel nostro programma di governo: in realtà la volete fare proprio perché state tradendo il vostro programma di governo. Non avete alzato le pensioni, non avete abbassato le tasse, state distruggendo la sanità pubblica. Ci tenete qui inchiodati per mesi quando fuori c'è un Paese che aspetta risposte, ma a voi interessa solo fare propaganda. Presidente, questa riforma è un castello di di bugie, un castello storto che non sta in piedi, affastellato di bugie, ma vedrete: saranno i cittadini a farlo crollare.

Un emendamento che dice che il Presidente può sciogliere le Camere soltanto quando risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo, fa una cosa meritoria anche sul piano della chiarezza istituzionale del presente. Non è soltanto una riforma, ma in un certo senso è anche una sorta di interpretazione autentica perché tutti i costituzionalisti, tutti gli osservatori e tutti gli studiosi riconoscono che in questo momento uno dei compiti del Presidente della Repubblica è preservare la vita della legislatura. Noi ci siamo trovati negli ultimi anni, quantomeno nelle ultime due legislature, ma forse ma forse anche prima, anzi senz'altro anche prima, in situazioni nelle quali ci sono state delle crisi chiuse dentro il Parlamento, durante la legislatura, che hanno richiesto anche una certa dose di creatività alle forze politiche e un notevole lavoro di cucitura da parte del Presidente della Repubblica. Molti osservatori e molti molti concittadini si sono chiesti perché se cade un Governo ci si mette così di buzzo buono a tentare di farne un altro. Non si potrebbe tornare a votare, visto che il Governo è caduto? Pensate per esempio alle convulsioni che attraversarono quest'Aula nei giorni della caduta del Governo Conte II. Ricordate la disperata ricerca di numeri, il famoso collega, quello che abitava sugli ulivi e abbracciava gli alberi,

poteva fare più in fretta e andare a votare. La ragione è che, come dicevo prima, tutti gli studiosi e tutti i costituzionalisti riconoscono, tra le responsabilità del Presidente della Repubblica, quella di fare in modo che la conservazione dell'organo costituzionale prevalga. Dunque, fintanto che c'è una maggioranza possibile, il Presidente deve adoperarsi per portare a casa

lavoriamo e viviamo nei palazzi della politica, è stato dato per scontato, gli studiosi l'hanno dato per scontato, probabilmente l'opinione pubblica si è anche chiesta dove si trovasse la ragione giuridica per per questa particolare impostazione. Io penso che metterla per iscritto darebbe un grande contributo alla chiarezza del funzionamento delle istituzioni all'intero corpo elettorale, ai nostri concittadini che ci osservano; ci darebbe la possibilità di spiegare che la prosecuzione e la durata della legislatura per la sua vita naturale è un valore costituzionalmente protetto, non è un'invenzione della dottrina, non è una bizzarria del mondo della politica, ma è cosa buona e giusta. È cosa corretta sul piano costituzionale proprio per il principio della conservazione della volontà popolare in un regime presidenziale. Quindi, se dobbiamo dire che il Presidente Repubblica può sciogliere le Camere, dobbiamo anche dire quando deve sciogliere, cioè quando non c'è più la maggioranza. Qui lo stiamo dicendo chiaramente, lo stiamo mettendo nero su bianco: diamo chiarezza e importiamo nella lettera costituzionale ciò che sta nello spirito della Costituzione e secondo me, quindi, il collega Verducci ha fatto un'ottima opera nella presentazione

Signor Presidente, intervengo semplicemente per dichiarare anch'io, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole a questo emendamento del senatore Verducci, che anche a me sembra importante. Ho condiviso molto la sua argomentazione e l'aver motivato la presentazione di questo emendamento per ricalibrare il sistema istituzionale e, quindi, ridare al ridare al Parlamento e al Presidente della Repubblica, per esempio nella gestione delle crisi, il ruolo che gli spetterebbe. Il senatore Scalfarotto, da parte sua, penso abbia ben inquadrato anche quello che è accaduto negli ultimi anni. Ragioniamo alla luce di quello che è successo, perlomeno

i colleghi, avvenne dentro un quadro di crisi profonda del sistema politico e in quel caso il Presidente della Repubblica che c'era all'epoca, l'onorevole Napolitano, scelse di estendere in maniera significativa i poteri della fisarmonica. Credo che fare una riflessione su questo in maniera seria sarebbe stato - questa sì - un'occasione per questo Parlamento. Io, per esempio, non ho alcun imbarazzo a dire che, dal mio punto di vista, considerai nel 2013 quell'apertura della fisarmonica forse addirittura eccessiva, onestamente non perché penso che fosse un errore da parte del Presidente della Repubblica, ma perché penso che il sistema politico aveva raggiunto un tale livello di crisi che, per quanto probabilmente quell'apertura fosse eccessiva, andasse però dinanzi all'unica soluzione praticabile. Insomma, il tema è esattamente questo. Il punto centrale della riflessione qual è? È un sistema politico sistema politico attorcigliato - mi viene da dire così - attorno a una crisi sistemica, oppure è l'idea di voler superare questi elementi di crisi, per l'appunto, con le scorciatoie? Per tornare al 2013, qual era il problema? I troppi poteri del Presidente della Repubblica o un sistema politico completamente incartato su se stesso? Io penso che se si sbaglia l'obiettivo della questione, poi diventa davvero difficile anche trovare le ragioni di crisi. È come la vicenda del Governo tecnico. Io non li amo particolarmente, faccio parte di un partito politico che ha contestato quasi tutti i Governi tecnici nati negli ultimi dieci anni, che non diede la fiducia al Governo Monti, che non ha dato la fiducia al Governo Draghi e che, per riprendere le osservazioni del collega Scalfarotto, quando è caduto il Governo Conte-*bis* ha detto: piuttosto che fare un Governo tecnico, si torni al voto e si dia di nuovo il potere di scelta al Paese. Paese. Pertanto, da molto tempo a questa parte e per formazione politica appartengo a questa scuola di pensiero. Tuttavia - e lo dico io, che i Governi tecnici non li amo - non si può sbagliare l'obiettivo della discussione. Il problema sono i Governi tecnici in sé o il problema è la crisi del quadro politico, che in alcuni casi rende inevitabile il ricorso ai Governi tecnici? Ci basta agire sul terreno regolamentare, come viene fatto, riducendo i poteri del Capo dello Stato, impedendo i Governi tecnici, imponendo lo scioglimento delle Camere ogniqualvolta si pone un elemento di crisi del Presidente del Consiglio per risolvere i problemi di natura sistemica che hanno attraversato la democrazia italiana negli ultimi vent'anni? Il tema sono i poteri del Presidente della Repubblica o è la crisi della forma partito e del sistema politico? Questo è il punto di fondo *(Applausi)* e su questo a me sarebbe piaciuto fare una riflessione seria in questo Parlamento. Secondo me, onestamente, c'erano le condizioni per mettere in campo un ragionamento su questo, se ognuno faceva lo sforzo di non partire con un elemento preconcetto, ma di provare anche a mettersi in ascolto delle ragioni della controparte politica. Se invece si va avanti con l'accetta, si propongono soluzioni come se fossero dei rimedi certi ad una condizione di crisi che, invece, probabilmente rimedi certi non ne ha, allora penso che si determina un totale cortocircuito. È per questo che poi diventa impossibile anche la ricerca di qualunque forma di mediazione. Questa è l'accusa maggiore che rivolgo alle forze politiche di centrodestra, perché in un Paese così diviso, così lacerato, così attraversato dai fenomeni a cui ho fatto riferimento prima, cioè al fatto che mezzo Paese non riconosce più nessuno di noi, dinanzi a questa situazione di sfacelo si sarebbe dovuto porre il problema di come ricostruire degli elementi che riguardano il tessuto connettivo di una democrazia, piuttosto che andare avanti con l'accetta e fare finta che un dibattito politico serio come questo venga piegato a un interesse di parte. Io penso che sia un errore davvero molto grave. senatore De Cristofaro, ribadire il voto del Gruppo Fratelli d'Italia contro questo emendamento e gli altri simili, anche secondo il parere del relatore e del Governo, facendo una notazione. L'argomento che forse viene toccato maggiormente dall'opposizione è la questione che, secondo loro, con il provvedimento in discussione limitiamo i poteri del Capo dello Stato. Ebbene, oggi il comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione afferma che: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere sciogliere le Camere o anche una sola di esse.». Ebbene, siamo di fronte a 90 pagine di emendamenti presentati dall'opposizione che limitano questo potere.

qualora risulti impossibile; può sciogliere le Camere solo se; a seguito di questo o di quello; nel caso di impossibilità di funzionare regolarmente; solo a seguito di, eccetera. Sono 90 pagine di limitazioni dei poteri del Presidente della Repubblica. Viva la coerenza.

vorrei precisare che questa è una norma di raccordo, quindi una norma necessitata, perché

siccome si continua a dire che noi limitiamo i poteri del Capo dello Stato, forse bisognerebbe leggere gli atti dei lavori dei Padri costituenti e capire perché questa norma è nata e si dice che il che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Questa è una norma che è stata congegnata per restringere i poteri del Presidente della Repubblica perché si temeva allora che il Presidente della Repubblica rinnovare un Parlamento favorevole alla propria rielezione oppure all'elezione di un candidato a lui collegato. Quindi, è proprio tutto il contrario di quello che state affermando, perché questa norma nasce proprio per limitare i poteri del Presidente della Repubblica. Interpretando alcune obiezioni, se il Governo interviene nel merito di questo emendamento, non si considera riapertura del dibattito. Questo lo dico

questione. Colleghi, l'interpretazione è piuttosto autentica: se il Governo interviene nel merito dell'emendamento che si sta trattando, non si considera riapertura del dibattito;

ma almeno per quanto riguarda la Camera che ho presieduto, questa è un'interpretazione del tutto inedita. *(Applausi)*. Adesso vorrei sapere in base a che cosa lei ha dato questa pronuncia. Sulla un articolo del Regolamento? Se lei mi dice a che cosa fa riferimento, mi aiuta a evitare di sbagliare per il futuro, perché è la prima volta da quando sono nelle Aule parlamentari che sento questa interpretazione. Presidente Casini, in questo caso il Governo è intervenuto in una sorta di precisazione, quindi non la consideriamo una riapertura del dibattito. Grazie.

che c'è una regola per cui se il Ministro parla nel merito dell'emendamento non si riapre il dibattito, perché questa è una cosa sconvolgente. Questa circostanza non è mai capitata, a meno che lei non mi citi i precedenti e l'articolo. Se lei me li cita dirò che ho sbagliato io perché probabilmente alla Camera è diverso che al Senato.

dopo l'intervento di cui al comma 1,» - quindi dopo la discussione generale - «prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni» - è evidente che l'oggetto è quello in esame e che queste sono dichiarazioni ulteriori senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare». Mi sembra che non ci sia interpretazione da fare di questo passaggio regolamentare. Ha ripreso la parola il Governo e ha reso ulteriori dichiarazioni nell'ambito dell'oggetto di cui stiamo discutendo; non ha parlato dell'atterraggio su Marte, ma ha parlato sull'oggetto. Questo, comunque, riapre i termini per una nuova discussione: faremo un intervento per Gruppo, perderemo più minuti a discutere delle ulteriori dichiarazioni fatte dal ministro Casellati, dopodiché riprenderemo ordinatamente il voto sugli emendamenti. Credo che ci sia poco da interpretare.

La Presidenza aveva dato una interpretazione. Siccome capisco che le opposizioni insistono su questo, l'articolo 99 dice che, nel caso diverso, si apre una nuova discussione alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Io la parola

è ricorsa ai lavori preparatori della Costituzione. la ministra Casellati è anche la presidente Casellati, nel senso che ha seduto su quello scranno in modo molto autorevole e, quindi, sono certissimo che, quando ho preso la parola, era perfettamente consapevole del fatto che avrebbe riaperto il dibattito. Immagino che abbia voluto farlo. Una persona così esperta che ha presieduto il Senato e fa il Ministro delle riforme costituzionali come può non sapere che, prendendo la parola, riapre il dibattito? Sono stupito anche del fatto che ne stiamo discutendo. Volevo soltanto dire questo, signor Presidente; lo consideri come lei ritiene, ma ci tenevo a dirlo. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e poi il nostro Gruppo si riserva di intervenire - rispettando il suo invito a

non è intervenuta sull'emendamento del senatore Verducci, ma è intervenuta dicendo la sua - ovviamente ci trova assolutamente contrari - sull'articolo nel suo insieme e ha fatto delle valutazioni che hanno riaperto il dibattito. la ringrazio per aver consentito ai Gruppi di intervenire, però c'è un tema che le pongo e chiedo di sottoporlo ancora al presidente La Russa: questi nostri interventi - il mio, quello del presidente Patuanelli, quello del presidente Enrico Borghi - non possono essere conteggiati nel tempo complessivo che i Gruppi hanno *(Applausi)*, perché questo significa sottrarci la parola. In questo momento noi siamo intervenuti semplicemente per mettere in evidenza alla Presidenza che l'intervento della ministra Casellati necessitava nuovi interventi da parte dei Gruppi. Se lei ogni mia vocale e ogni mia consonante la sottrae dalla quantità di tempo che il Gruppo del Partito Democratico ha a disposizione, allora anche non volendo, lei non ci sta consentendo di partecipare al dibattito. Questo è quanto noi contestiamo e su cui insistiamo. Torno a richiederle una convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, perché abbiamo la necessità di capire

Boccia, ovviamente insisterò nel farmi tramite con la Presidenza per la convocazione. Il mio pensiero è che su un argomento così importante e delicato gli interventi sull'ordine dei lavori debbano avere una considerazione: al momento, appunto conteggiati esattamente, e ne siamo tutti consapevoli. È evidente che su una discussione così importante forse bisogna che la Conferenza dei Capigruppo tratti anche questo. ci sono volute giornate di discussione per sentire dal Capogruppo del principale partito di maggioranza e poi dalla Ministra considerazioni che ci fanno dubitare che abbiano contezza della Costituzione vigente. *(Applausi)*. Senatore Malan, ma lei lo sa che oggi, a Costituzione vigente, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere quando gli pare e piace? Lo sa questo? Oggi, a Costituzione vigente, l'emendamento a prima firma del senatore Verducci ripropone sostanzialmente il principio in base al quale le Camere si possono sciogliere da parte del Presidente della Repubblica solo ed esclusivamente quando non sono in grado di formare una maggioranza né di esprimere un Governo. Invece, cosa proponete voi? Ministra Casellati, cosa sta proponendo lei? Propone che le Camere non vengano più sciolte dal Presidente della Repubblica quando non sono in grado di esprimere una maggioranza, ma quando lo chiede il Presidente del Consiglio: questo è il punto. La durata della legislatura dipende non più dalla capacità delle forze politiche di costruire una maggioranza di Governo, ma dalla volontà del Presidente del Consiglio. Questo è il ribaltamento che state praticando e ci viene il dubbio che forse non abbiate neanche ben capito cosa state proponendo: altrimenti, come si fa a dire che questo emendamento e quelli che seguono evidenziano la nostra ipocrisia e la nostra contraddizione? Noi stiamo riaffermando il principio della sovranità e della primazia del Parlamento sul Governo, che vuol dire primazia del pluralismo sull'uno o sull'una. Come fate a risponderci dicendo che questi emendamenti stanno limitando il potere del Presidente della Repubblica? Per cortesia, un po' di serietà!

Borghi, si rivolga alla Presidenza.

che si possono riassumere in una sola: la maggioranza sta procedendo con il cingolato sopra la Costituzione. *(Applausi)*. Voi state procedendo con il carro armato sul bene più prezioso che questo Paese ha, che è la Costituzione, che lo tiene in piedi e unito. Il contingentamento dei tempi della discussione di questa riforma costituzionale che è stato imposto ai Gruppi di opposizione è già di per sé inaccettabile. È stato deciso nelle chiuse stanze della Conferenza dei Capigruppo e quest'Assemblea non ha la minima possibilità di deliberare al riguardo. *(Applausi)*. Deve subire in silenzio e in silenzio rimarrà,

per discutere della riforma costituzionale, la madre di tutte le riforme, che improvvisamente è diventata la zia. Un'altra cosa inaccettabile sta succedendo. Questa discussione nasce per l'errore di un componente del Governo, e parlo di errore perché ritengo

che si apra una discussione. Questa discussione non può essere conteggiata in quello scarsissimo tempo che è rimasto ai Gruppi di opposizione per discutere della riforma costituzionale. Quindi chiedo due cose. Anzitutto, tutto questo tempo deve venire

Quanto alle ultime, la senatrice Maiorino ha detto che il ministro Casellati ha sbagliato. Il ministro Casellati ha diritto di intervenire quando lo ritiene: il Regolamento lo prevede ed è quindi intervenuta. La Presidenza ha dato le sue interpretazioni e mi pare che abbia dato completa soddisfazione a tutti. Aggiungo una cosa sulla questione dei tempi. In ogni legislatura, con ogni Presidenza e maggioranza, i richiami al Regolamento e simili sono sempre stati conteggiati nel tempo contingentato. *(Applausi)*. Ripeto: sempre. In ultimo, devo essere particolarmente grato al senatore Giorgis perché ci ha spiegato che la Costituzione non dice quello che c'è scritto, ma dice quello che pensa lui. E lui è libero di pensarlo. *(Applausi)*. Purtroppo ci sono altri che hanno quest'idea cui la Costituzione dice una cosa, ma adesso noi siamo molto più furbi dei Padri costituenti e le facciamo dire un'altra cosa. L'articolo 88 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i Presidenti: punto, senza alcuna condizione. Ricordo che nel 1994

prendiamo atto della sua opinione, che non è la nostra. Secondo noi la Costituzione continua a dire quello che c'è scritto e non quello che qualcuno ritiene dica.

Signora Presidente, io penso che per cercare...

Presidente. Associandomi alle considerazioni fatte dai Capigruppo dell'opposizione, per consentire un'utile prosecuzione dei nostri lavori, credo sia indispensabile la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, la quale, in questa modalità un po' singolare e un po' aleatoria dell'organizzazione dei nostri lavori, si è detto che sarebbe stata convocata mercoledì; così, senza un orario, senza una puntualità. Esatto, ha ragione il senatore Delrio: quale mercoledì? Sostanzialmente mercoledì? Sostanzialmente noi stiamo immaginando di lavorare alla modifica della Costituzione in una modalità - diciamo così - un pochino abborracciata, nella quale le inevitabili tensioni che la politica porta con sé incrociano anche le questioni di questa mattina - chiudo, signora Presidente - per le quali mi verrebbe da richiamare Talleyrand,

sull'emendamento, a partire dalla considerazione che ha fatto il collega Giorgis riferendosi all'emendamento Verducci, che dice sostanzialmente che, fino a quando non si verifica nell'Aula la possibilità che nasca una nuova maggioranza e quindi nasca un Governo, non si possono sciogliere le Camere; e ciò perché in qualche modo si restituisce al Parlamento quella centralità che dovrebbe avere, come per l'appunto stiamo cercando di dire. Giustamente viene osservato da parte del Governo arriva invece una proposta che sposta nelle mani del Presidente del Consiglio la facoltà di fatto di sciogliere le Camere. Questa cosa dimostra esattamente quello che stiamo cercando di dire da molte settimane, cioè che tale proposta, che è stata immaginata dal Governo, non solo è totalmente differente da quella che piacerebbe a noi - questo mi pare che si sia sufficientemente compreso ma è anche profondamente diversa da quei sistemi puramente presidenziali dove l'autonomia del Parlamento nei confronti del Presidente eletto dal popolo rimane sacra. vuol dire che anche in quei Paesi del mondo dove esiste un sistema di elezione diretta, finanche un sistema di elezione diretta presidenziale, questo questo meccanismo di forte accumulazione dei poteri nelle mani del Presidente eletto dal popolo - si è fatto innumerevoli volte riferimento per esempio al presidente degli Stati Uniti d'America - mette comunque il Parlamento in una condizione di altrettanta condizione di altrettanta forza. Qui il tema è esattamente questo squilibrio. Non viene presentata una proposta che tiene saldo questo principio,

per cui il Presidente eletto dal popolo non solo ha l'investitura popolare, ma ha anche un tale elemento di dominio nei confronti del Parlamento che prima lo trascina cioè grazie a se stesso lo trascina e lo elegge - e poi però lo scioglie, se lo ritiene. Quindi, capite bene il totale cortocircuito e capite bene anche come questa proposta sia una profonda forzatura nei confronti di quei sistemi puramente parlamentari come quello italiano degli ultimi decenni, ma anche in totale distonia rispetto a quei sistemi puramente presidenziali, che a me personalmente non piacciono, ma che perlomeno rispettano il principio cardine dell'equilibrio dei poteri.

del provvedimento e delle modifiche da noi proposte: *magis amica veritas*. Non entrerò - come hanno fatto i miei colleghi prima di me - sulle giravolte del Presidente del Consiglio, del premierato come madre di tutte le battaglie, su quel "o la va o la spacca", fino all'*hic manebimus optime*, vada come vada. Ci sono le elezioni europee, tutto si confonde ed è rumore di fondo, certo non di buon auspicio per il ministro Alberti Casellati. Attenzione, però, perché in quel "o la va o la spacca", evidentemente, lo stesso Presidente del Consiglio, una volta uscito dalla tridimensionalità di un incontro pubblico e diventato lancio di agenzia e titolo di giornale, ha ritrovato il sapore amaro dei pieni poteri del suo sodale, Matteo Salvini, quello che ha ballato una sola estate. È quel momento in cui il favore si trasforma nel suo rovescio, quando gli stessi che ti osannano all'improvviso vengono inquietati da un istantaneo, a volte irrevocabile: ma siamo proprio sicuri? Presidente, se l'agnizione la ritroveremo nelle urne di Fratelli d'Italia o se, invece, ce la beviamo ancora per un po'. Il tentativo del premierato è esattamente questo: provare a prolungare il più possibile, mettendo mano addirittura alla Costituzione, l'orizzonte di questo Governo. Come faccio a durare il più possibile, con obiettivo ventennio, se non cambio la Carta, nella quale peraltro la mia parte politica si è ritrovata sempre il giusto? Facendo mostra, peraltro, di avere acconsentito a un cambio di destinazione d'uso rispetto allo storico obiettivo del presidenzialismo? Leggevo ieri le dichiarazioni di di Almirante in un qualche *blob*: ma come? Vi siamo venuti incontro, abbandonando la nostra storica battaglia del Presidente eletto direttamente dal popolo, e così ci ripagate? Così mi ripagate? Con il risultato camuso di una riforma o pretesa tale, che non è quella che volevate e che certo non è quella su cui possiamo dare la nostra adesione, tanto è grave lo sfregio sfregio alla Costituzione. Quindi, state portando avanti un disegno che non vi corrisponde e sappiamo ovviamente tutti perché: il baratto con la Lega, che pare più uno scambio di prigionieri sul ponte delle spie che un accordo tra alleati, e che, dunque, difendete a testa bassa solo perché ormai vi siete esposti, perché siete andati troppo avanti, perché vi domandate: come faccio ora a tornare indietro? Che figura ci farei? Quello che mi colpisce del loro premierato, però, signor Presidente, è che mi sembra esso suoni anche come un giudizio inappellabile del Presidente del Consiglio nei confronti della sua classe dirigente. Che ci sia un divario, qualcuno lo definisce un abisso, tra il *Premier*, i suoi riconosciuti talenti, e la sua intendenza, con rare e significative eccezioni, è non una malignità, ma un truismo, tanto che questo provvedimento mi pare espliciti proprio la cattiva fede nei confronti dei suoi. È un *simul stabunt*, che lega le sorti dell'intero Parlamento alla forza e al ruolo del Presidente del Consiglio. come se lo stallo alla messicana tra Fratelli d'Italia e Lega - con Forza Italia che, mi dispiace, non ha un ruolo riconoscibile ed udibile in questa riforma - abiti già anche il partito del *Premier*: ma dove andate senza di me, con buona pace di Rampelli. Siete legati a me a doppio filo e, per evitare tentazioni o congiure, dopo di me il diluvio. ci troveremo di fronte a un regolamento di conti interno, spacciato per la riforma di cui il Paese ha bisogno da anni, anzi da decenni, secoli, millenni, eoni. Poi, però, si a va a vedere in filigrana e si trova il filo liso della politica, la vecchia politica, quella di sempre, con l'ambizione personale, l'illusione di interpretare di interpretare chissà quale *esprit du temps*, con tutta la diffidenza nei confronti della vil razza dannata e una *suasion* molto poco *moral*, per durare più a lungo. È il comandamento del potere, che in Italia viene sempre negletto e deriso dalla nostra imprevedibilità, dal nostro scartare di lato, dall'etica del telecomando, che ci ammalia all'istante e l'istante successivo ci fa cambiare canale, condannandoci a un compulsivo *zapping* di cui lamentarci come una maledizione. C'è un momento, Presidente, in quello scintillante e vivido film che è «La chimera» di Alice Rohrwacher, nel quale i tombaroli, di fronte alla meravigliosa statua di una dea in un anfratto della terra, le spezzano la testa, perché l'unico modo di portare via quel ritrovamento era quello di farlo a pezzi e venderlo a frammenti. Ecco, questo furbo sacrilegio nel film viene poi punito. In conclusione, colleghi, siamo ancora agli inizi e vi potrà sembrare lontano il momento della resa dei conti per quello che state facendo in quest'Aula. Ma la sanzione coincide con il momento stesso di questo scasso, non dopo, in un poi che non riuscite a intravedere e che oggi deridete. Pensateci perché, infranta la sua simmetrica integrità, della Costituzione che volete vendere a pezzi agli italiani non restano altro che la vostra ambizione smisurata, la vostra malfidata arroganza e la vostra scarsa fiducia in questo Paese e nella sua gente. Nulla in mano, cocci. *(Applausi)*. Grazie,

il nostro sistema costituzionale, il suo equilibrio e la nostra democrazia rappresentativa vengano colpiti al cuore. Questo è del tutto evidente anche per il dibattito che in parte si è sviluppato nel corso degli ultimi giorni in Aula e nei giorni scorsi anche per le affermazioni della Presidente del Consiglio. Colleghi, il lessico in politica non è una variabile, le parole non sono mai indifferenti e in questo fine settimana la Presidente del Consiglio ha utilizzato una terminologia indicativa di come effettivamente interpreta nella sua testa e per la sua cultura politica la va o la spacca" può essere l'espressione di un liceale prima dell'ultima interrogazione per non avere un debito; può essere l'espressione di uno studente universitario nell'ultimo appello di una sessione, ma non può esistere questa espressione quando parliamo di riforme istituzionali. *(Applausi)*. È infatti la dimostrazione di una prepotenza politica, culturale e anche di una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e del suo ruolo. La nostra Costituzione non è stata scritta con questo principio: è stata il risultato di un incontro tra punti di partenza assolutamente diversi, di una mediazione in un Paese complesso, che aveva su di sé le scorie della dittatura e della guerra. Questo atteggiamento mentale, invece, tradotto con questo tipo di lessico istituzionale sgrammaticato, è seriamente preoccupante per il destino della nostra Repubblica e sicuramente per il prosieguo di un confronto che questa maggioranza non vuole portare non è nemmeno semplicemente il fatto che siamo vicini a un appuntamento elettorale e ciascuno deve esibire la propria bandierina; e allora c'è chi esibisce la sanatoria per la casa, chi quella relativa all'autovelox, chi riparla della separazione delle carriere. Tutto questo non può riguardare una cosa così seria, importante e delicata come la nostra democrazia. E poi, se al "o la va o la spacca", si aggiungono la necessità e la volontà di rivedere i poteri del capo dello Stato, allora il livello di attenzione deve diventare ancora più grande e deve crescere ancora di più. Sì, perché state preparando una concentrazione di poteri in un'unica figura, quella del Presidente del Consiglio, che non ha eguali in nessuna parte del mondo. C'è il rischio - riflettete su questo punto - che il populismo si impadronisca dei gangli vitali della nostra democrazia. Fate apparire oggi il cittadino più in grado di scegliere. Ma, in realtà, state riducendo l'agibilità e la libertà dei cittadini, perché avranno meno spazio per essere protagonisti nel processo democratico. La disintermediazione, il concentrare i poteri nelle mani di una sola figura, può essere un salto nel buio pericoloso, in cui non troveranno spazio i corpi intermedi, le forze sociali, perché tutto ruoterà intorno al ruolo del Presidente del Consiglio. La riduzione di questa partecipazione democratica rischia, appunto, di rendere le nostre istituzioni più fragili, meno plurali, meno rappresentative, meno democratiche e più esposte a pulsioni di mero Del resto, questo è l'*humus* culturale che noi stiamo vedendo in tutto questo periodo: di questo ci parla il vostro atteggiamento sulla RAI, sulla libertà di stampa, sull'aggressione a chi la pensa diversamente, su chi è diverso il fatto di voler ripetere votazioni quando non vi stanno bene, con un conflitto strisciante tra i poteri dello Stato, come per esempio nel caso della magistratura. Tutto questo segnala un'oggettiva insofferenza per una democrazia bilanciata, ma soprattutto la vostra è un'insofferenza ideologica per la nostra Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione e dalla Resistenza.

Presidente, ho assistito con un certo sconcerto e con un po' di incredulità alle dichiarazioni che hanno fatto su questo articolo il senatore Malan e la ministra Casellati, tanto da domandarmi se davvero credono in quello che dicono. Non si può far finta di non capire la portata dirompente della riforma che questo articolo propone. E mi pare non si sia discusso abbastanza nemmeno oggi di questa portata dirompente. Allora, alla ministra Casellati che richiama i dibattiti dell'Assemblea costituente, che tutti noi amiamo e conosciamo molto bene, voglio ricordare che il motivo per cui venne inserito il divieto di scioglimento nei sei mesi prima delle elezioni - cara Ministra - aveva a che vedere con il fatto che l'elezione del Presidente della Repubblica, cioè di quella che Mortati definì la suprema magistratura di persuasione del nostro ordinamento, non doveva in alcun modo essere influenzata da una decisione, come quella di sciogliere le Camere e ricorrere alle elezioni, che, da chiunque presa, può essere un fattore di perturbamento di una cosa così delicata come l'elezione presidenziale. Se è così, se davvero si leggono gli atti della Costituente, quello che voi ci state proponendo è qualcosa che va esattamente contro lo spirito della discussione fatta a larghissima unità nell'Assemblea costituente. Provo a spiegarvelo con parole semplici, facendo ancora una volta finta di credere che ci vogliate ascoltare. Che cosa accade con quello che voi prevedete? Accade che al Presidente del Consiglio, con un'altra parte della riforma, viene attribuito un potere incondizionato di scioglimento delle Camere. Lo scioglimento delle Camere è qualcosa che il Presidente del Consiglio può fare quando vuole. Con l'intervento che fate sull'articolo 88 della Costituzione date, in sostanza, la possibilità al Presidente del Consiglio di disporre lo scioglimento delle Camere anche nei sei mesi precedenti l'elezione del Presidente della Repubblica. Ora, che vi sfugga l'enormità di questa previsione a me pare incredibile. Ripeto che voi volete dare al Presidente del Consiglio, che può sciogliere il Parlamento in qualsiasi momento, il potere di farlo anche nei sei mesi prima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Questo significa consegnare nelle mani del Capo del Governo, oltre a tutti gli altri poteri che gli affidate con le altre parti della riforma, il potere di esercitare un condizionamento indebito e finanche un ricatto sul Parlamento nel momento in cui il Parlamento si accinge a compiere il suo atto più solenne, che è l'elezione del Capo dello Stato. *(Applausi)*. Questo è ciò che fate con questo articolo. Che discussione ci proponete dicendoci che non si limitano i poteri del Capo dello Stato e che si rispetta lo spirito della discussione della Costituente? Andate esattamente in senso contrario. Un'azione come quella dell'elezione del Capo dello Stato, che, attraverso questo articolo, era sempre stata preservata da manovre politiche faziose, da domani diventerà il possibile ed anzi probabile oggetto di manovre politiche faziose, forzanti e squilibrati. *(Applausi)*. Questo fate e non ve ne rendete conto. Se il problema è che non ve ne rendete conto o siete in malafede, questo ci allarma molto; che ve ne rendete conto e ci state dicendo una cosa per un'altra. Il Governo è al telefono, perché probabilmente si farà dare l'interpretazione autentica di questo punto del disegno di legge. *(Applausi)*. Invece, fossi nel ministro Ciriani ascolterei perché, quando queste cose queste cose diventeranno chiare a una parte larga dell'opinione pubblica, indeboliranno fortemente la credibilità del vostro tentativo. Io penso che gli italiani accettano che si scherzi con qualsiasi cosa, ma non con la Costituzione e non con il prestigio, la terzietà, l'autorevolezza, la natura equilibratrice della carica del Presidente della Repubblica. Voi, con questo articolo, mettete l'elezione del Presidente della Repubblica malamente nelle mani non soltanto della maggioranza di turno, ma di chi *pro tempore* si trova a occupare Palazzo Chigi e che avrà nelle sue mani un potere non sufficientemente bilanciato e del tutto illimitato. Aprite gli occhi, non fate questa ferita alla nostra Costituzione.

Signora Presidente, come hanno già detto i miei colleghi, con questo articolo e gli emendamenti ad esso relativi entriamo sicuramente nel cuore del provvedimento. Io aggiungo alle considerazioni poc'anzi rese da molti dei miei colleghi una riflessione che abbiamo già fatto, però la vorrei riprendere perché secondo me calza proprio a pennello rispetto a questo articolo. Stiamo Stiamo provando a ribadire ancora una volta che quello che viene nei fatti fondamentalmente riscritto è l'equilibrio tra i poteri principali del nostro assetto costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento e Presidente del Consiglio.

invece, il potere e le funzioni del Parlamento, aggredire le criticità che pure c'erano, dando maggiori poteri al Parlamento, riconoscendone la centralità, quindi investendo su questa strada e su questo terreno.

lasciate intatto il primo comma, che dice che è potere del Presidente della Repubblica sciogliere le Camere, ma quella funzione, quella prerogativa voi la andate a intaccare successivamente negli altri articoli del disegno di legge e quindi nell'altra parte della riforma, con la quale rendete il Presidente del Consiglio

per garantire terzietà, ruolo di garanzia, funzione, autorevolezza del Presidente della Repubblica, quindi tenete in qualche modo ancora sotto scacco il Parlamento in uno dei suoi momenti vitali più significativi e importanti e lo fate mettendo tutto unicamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Questo fate con questo articolo, ancora una volta: mortificazione del ruolo del Parlamento e soprattutto quasi una delega in bianco solo ed esclusivamente nelle mani del Presidente del Consiglio. È su questo che proviamo a farvi riflettere. Quella che fate è una riforma che non può vivere, lo diciamo veramente in maniera semplice e accorata ma stando al merito, di furbizie e di astuzie; provate a non scrivere quello che volete fare e non ne siete convinti. Ve lo chiediamo ancora una volta: perché non siete chiari ed espliciti, perché non consentite né attraverso il dibattito parlamentare, né soprattutto, a questo punto, nel dialogo con il Paese, una verità su questa riforma? La verità è che voi continuate a mettere in discussione uno dei pochi ruoli che hanno funzionato veramente e che sono amati dal popolo italiano e lo fate per questo. Per questo non avete il coraggio di dire che toccate i poteri del Presidente della Repubblica e le sue prerogative: perché sapete che quella è una figura amata e apprezzata, avete paura delle vostre stesse azioni e non lo scrivete esplicitamente con un po' di furbizia e di astuzia. Provate in qualche modo a far vedere che formalmente non toccate i suoi poteri, ma nei fatti sottraete al Presidente della Repubblica

delicati e difficili della vita del Parlamento. Togliete al Presidente della Repubblica questi poteri, li mettete esclusivamente nelle mani del Presidente del Consiglio e mortificate del tutto il ruolo del Parlamento. Con questo articolo entriamo nel cuore della riforma anche per questo, perché sostanzialmente date una botta importante, decisiva e significativa alla vita, all'autorevolezza e all'autonomia del Parlamento. Presidente, credo che siamo arrivati al momento di dirci le cose schiettamente. Devo dire la verità: ho molto apprezzato il fatto che la presidente Casellati abbia deciso di interloquire con questa Camera, mi sembra Mi sembra anche giusto che poi abbiamo potuto interloquire con lei. È così che si procede, quindi bene. Visto che c'è disponibilità del Governo a parlare, ne approfitterei. ne approfitterei. Adesso stiamo discutendo dell'articolo 3, ma di fatto esso ha un legame strettissimo con l'articolo 7. Lo diceva anche la Ministra: è un articolo di coordinamento. La Ministra ci ha spiegato, nella lezione che ha voluto dare a questa Camera, quale sia stata l'intenzione sul semestre bianco dei Costituenti: evitare che il Presidente della Repubblica che stia per terminare il suo mandato decida di ricorrere alle urne per avere l'elezione di una Camera a lui o a lei amica, in modo tale da farsi rieleggere.

qualche anno fa ha collaborato con la sua allora predecessora, la ministra Boschi. So che cosa significa fare il lavoro che state facendo, lo rispetto profondamente e anzi auspico che vada in porto, perché queste istituzioni oggi non funzionano come dovrebbero. A me dispiace che questa soluzione sia così pasticciata, che gli errori fatti siano così grevi e che crassa appaia proprio la superficialità con la quale ella, signora Ministra, i suoi collaboratori e questa maggioranza avete avvicinato uno sforzo così alto e importante *(Applausi)*che avrebbe meritato ben altra attenzione, riflessione, approfondimento. Mi scusi, signora Ministra, mi faccia capire. Qui c'è una norma che si capisce: «in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere». Benissimo. C'è l'elezione diretta, ma se il Presidente del Consiglio perde la fiducia, si torna al voto: lo dicevamo prima e questo è quello che chiede l'elettore, ossia una consequenzialità tra il voto e l'esito del voto. «in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre (…) lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone».

Che proposta è la proposta che non si può rifiutare? Francamente non l'ho mai vista e mi pare quasi irrispettosa dell'alta magistratura che il Quirinale rappresenta.

o nel caso muoia (qui capiamo che la forza maggiore avanza e c'è impedimento permanente o decadenza), il Presidente della Repubblica può conferire per una sola volta nel corso della legislatura l'incarico di formare il Governo a un altro parlamentare. Può conferire,

la massima attenzione e la massima apertura, però chiediamo che lo sforzo sia all'altezza della responsabilità che ricopriamo. *(Applausi)*. Mi lasci dire, con grande rammarico, signora Ministra, che io purtroppo questa responsabilità, considerato che si mette mano alla Costituzione, come è giusto *ex* articolo 138, in questo caso non la vedo. Vedo dilettantismo, un grande pressappochismo, una grande superficialità e davvero me ne dispiaccio. Grazie,

l'infantilismo. Dobbiamo affrontare un'altra cosa: qui la questione non è, come qualcuno ha detto, se non state capendo o siete in malafede,

Loro possono fare tutto! Poiché io sono Giorgia, posso anche a cancellare dal palinsesto di una televisione uno scrittore che non dice quello che mi piace; piace; posso cancellare anche una conferenza stampa e non accettare il contraddittorio con i giornalisti; posso fermare un treno; posso rivolgermi a un Presidente di Regione insultandolo, durante un saluto ufficiale e formale. E sapete perché lo potete fare? Perché voi siete Giorgia e potete fare

Grazie,

me correttamente e giustamente dal suo punto di vista, che però è anche il nostro, cosa succede quando si interpreta nella maniera sbagliata, com'è stato fatto in tutti questi mesi, una questione così seria come mettere mano alla Costituzione repubblicana…

Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione della Presidenza. Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione della Presidenza. *(Commenti).* Non vedo cosa ci sia da contestare con riguardo a queste parole. O non dobbiamo valutarle?

ai fini della convocazione immediata del Consiglio di Presidenza per le valutazioni di competenza del Consiglio medesimo. Inoltre, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, la seduta sarà sospesa fino alle ore 14. Resta fermo il termine di conclusione dei lavori di oggi per le ore 20, mentre la seduta di domani non avrà luogo, così come non sono previsti lavori per la successiva settimana in vista delle elezioni europee. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 giugno, alle ore 16,

litania, secondo la quale, anche con questo articolo, si limiterebbero i poteri del Presidente, litania peraltro in parte smentita da alcuni interventi della stessa opposizione. Francamente, rispetto all'intervento del collega De Cristofaro, ho apprezzato la sua onestà intellettuale nel riconoscere quello che è stato riconosciuto da tanti illustri costituzionalisti, che si sono alternati nelle lunghe audizioni che ci sono state

delle crisi di Governo, i poteri del Presidente della Repubblica si sono espansi in maniera particolarmente significativa. Rispetto a questo, ringrazio il collega De Cristofaro per aver citato una fase particolarmente complicata e delicata della vita della nostra Repubblica,

per sanare situazioni che invece sono determinate dall'instabilità sistemica, che è il vero ed è il principale problema. Ed è curioso come in quest'Aula così come in Commissione, in diverse occasioni, occasioni, la gran parte delle opposizioni abbia più volte richiamato lo strumento della sfiducia costruttiva, tema sul quale in più di un'occasione

una limitazione delle prerogative del Capo dello Stato. Evidenzio, peraltro, che proprio in questo emendamento si fa richiamo ad una

Il Senato è in numero legale.

Signor Presidente, siamo nel cuore della proposta, perché nell'articolo 3, se ne avessimo ancora avuto bisogno, appaiono in modo molto chiaro gli intendimenti della maggioranza. Le modifiche contenute in questo articolo rappresentano le premesse per trasferire in modo chiaro - impossibile non vederlo - nelle mani del Presidente del Consiglio poteri fino ad oggi custoditi dal Capo dello Stato, e costituiscono l'*habitus* anche per i successivi provvedimenti. Quello che per me è sconcertante è come sia facile per la maggioranza e per il Governo

chiaro), ma con i cittadini e le cittadine. Si continua a dire, a partire dalla Ministra, che non è vero che al Presidente della Repubblica vengono tolti i poteri. Lo abbiamo visto nel togliere il potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori e le senatrici a vita; abbiamo anche visto lo spregio con cui vengono considerati dalla maggioranza e oggi, in modo molto più chiaro, mettendo tra l'altro in parallelo questa riforma con l'autonomia differenziata, è evidente di come la concentrazione dei poteri in mano solo al Presidente del Consiglio toglie di fatto le competenze e le prerogative del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Non siamo stupiti da questo: è da un anno e mezzo che, decreto-legge dopo decreto-legge, messa all'angolo della stampa, della libertà di stampa, noi assistiamo a una ingordigia di potere mai conosciuta nel nostro Paese. Sono chiari anche gli intendimenti è chiaro dove si vuole arrivare: uno sbilanciamento completo di potere e di ruoli istituzionali, cosa esattamente contraria allo spirito che ha animato le Madri e i Padri costituenti quando hanno scritto la nostra Costituzione. Come Partito Democratico, ogni emendamento, anche quelli che ho presentato, volgono proprio ad arginare e fermare una deriva di concentrazione dei poteri che mette in discussione il diritto della partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Addirittura la possibilità del Presidente del Consiglio - come ha ben ricordato il collega Parrin - di far cadere le Camere e influenzare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica la dice lunga su come abbiamo completamente smarrito, quel senso di democrazia partecipata *(Applausi)*, di diritto alla partecipazione, che sono carne e sangue della nostra Costituzione.

cento dei cittadini e delle cittadine decidono di non andare a votare, ben consapevoli di cosa significhi, in modo particolare i giovani. Mi chiedo, con uno sbilanciamento dei poteri come quello prefigurato, che ci vogliono imporre, cosa ne sarà del diritto partecipativo degli uomini e delle donne nel nostro Paese. Non solo. Siamo un Paese forte delle sue associazioni e dei suoi modelli partecipativi: le organizzazioni sindacali confederali rappresentano circa 15 milioni di persone un mondo del volontariato, laico e cattolico, che nessun altro Paese europeo conosce. Cosa sarà tutto questo valore partecipativo, con il potere in mano a uno solo? No, noi non permetteremo tutto questo e che nessuno pensi a man bassa di utilizzare ogni strumento - il premio di maggioranza, il modello del premierato una sottovalutazione totale del diritto di partecipazione dei cittadini - per cambiare in peggio il nostro Paese. Faremo tutto quello che potremo per opporci.

vorrei intervenire, cercando di provare a ragionare, sostanzialmente la modifica di questo articolo sarebbe tendente a interpretare la volontà dei costituenti.

se sciogliere o meno le Camere, perché non è solo una prerogativa del Presidente della Repubblica. Vorrei sottolineare che, visto e considerato che si continua a dire che bisogna essere eletti, quindi con il mandato dei cittadini, se una sola persona eletta dai cittadini può mandare a casa 600 tra deputati e senatori altrettanto eletti dai cittadini, è chiaro che è un potere a dismisura, da questo punto di vista, perché anche i senatori e i deputati sono eletti dai cittadini. Speriamo che la nuova legge elettorale preveda anche le preferenze e che semmai

rinascere nel Paese una molteplicità di soggetti, a partire dai partiti politici, per i quali - sottolineo - dovremmo prevedere anche il finanziamento pubblico, perché possano in sostanza costruire quella capacità di selezione dei gruppi dirigenti ed essere quelle casematte in grado di trasmettere il rapporto tra quello che succede in quest'Aula e la società. Questo è il dato che dovremmo discutere; dovremmo discutere di queste cose. Io

all'autoritarismo è la partecipazione; non ci sono altri mezzi. Fondamentalmente è il livello partecipativo che garantisce la democrazia in un Paese. Per questa ragione, ovviamente, sosterrò questo emendamento, come ho fatto con altri, però insisto che questo è il punto. Discuteremo. La maggioranza vuole imporre questa riforma sbagliata, che è unica al mondo (anche questo la dice lunga), senza nessuna disponibilità al confronto. Anche questo è un modo autoritario per imporre le scelte.

va definito come un vero e proprio disastro di diritto costituzionale. Vorrei far notare, Presidente, che questa riforma - lo dico a lei e per il suo tramite anche ai colleghi di maggioranza - è un tradimento è un tradimento degli elettori della maggioranza, perché è stata data loro l'illusione che si voleva addirittura valorizzare la figura del Presidente della Repubblica. Si parlava di presidenzialismo, di una valorizzazione del Presidente della Repubblica. Bene, si è visto come l'avete valorizzato: avete iniziato smantellando e depotenziando i poteri del Presidente della Repubblica. Il primo tradimento lo avete fatto ai vostri elettori. Ed è un tradimento perché tradisce anche i cittadini che non sono vostri elettori; tradisce quei cittadini, perché state continuando e state perseverando nel mandare avanti degli slogan manipolatori, in cui vi limitate a dire che si farà un'elezione diretta del *Premier*, dando ad intendere che sia lo stesso *Premier* che oggi conosciamo, con i poteri che conosciamo, sottacendo volutamente volutamente il reale contenuto della riforma, ossia che questo *Premier* avrà dei poteri che non ha neppure il Presidente degli Stati Uniti, potrà dimettersi e sciogliere le Camere. E quel Presidente della Repubblica, che in campagna elettorale volevate valorizzare così tanto, non potrà aprire bocca. Presidente, questa riforma è un tradimento. Ma soprattutto è un tradimento dell'anima democratica e pluralista del nostro Paese. Questo autoritarismo è l'antitesi della democrazia ed è l'antitesi del pluralismo. È un tradimento perché vendete anche l'illusione che si possa per legge creare il bipolarismo. Il bipolarismo non si crea per legge; andrete a creare delle coalizioni che sono soltanto una sommatoria di voti, collage di programmi diversi, per cui, come vediamo oggi, la Lega, che vuole il decentramento del potere, voterà per una concentrazione del potere e per una centralizzazione del potere. Noi del MoVimento 5 Stelle, Presidente, non vogliamo essere complici di questo scempio di diritto costituzionale oltre ad essere un tradimento degli italiani, è un tradimento della Costituzione, è un attacco ai poteri costituzionali, è un attacco al Parlamento che non ha precedenti. Presidente, per coerenza, a questo punto la maggioranza ha detto che ha modificato pochi articoli, ma forse ha dimenticato di modificarne uno, che quantomeno è stato di fatto già depotenziato: l'articolo 1 della Costituzione. L'inizio dell'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica democratica».

bisogna poi ripetere delle affermazioni. La ripetizione delle affermazioni, però, non le rende vere. Si sostiene, come molti sanno, che a ripetere una notizia falsa si finisce per farla diventare vera. Allora, di tanto in tanto, noi dobbiamo fare qualche puntualizzazione, perché, se il Ministro interviene, allora si riapre il dibattito e si cercano pretesti regolamentari, mentre quello era anche un modo per dare delle spiegazioni. Ieri siamo arrivati all'assurdo, con i Gruppi di opposizione che si opponevano all'articolo 2, che era frutto del recepimento di una proposta che veniva dalle opposizioni e che, in qualche modo, rafforza la trasversalità della figura del Presidente della Repubblica. Noi siamo ora sull'articolo 3, ma l'articolo 2 proroga, proroga, nel numero delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento, un *quorum* più ampio. Vuol dire che la parte politica che ha la maggioranza del Parlamento, che a rotazione decidono gli elettori, si spoglia del potere di eleggere il Presidente e moltiplica il numero delle votazioni; votazioni nelle quali, essendo alto il *quorum*, si deve cercare una condivisione. Questo è accaduto, ma non lo si racconta. Si dice che c'è il colpo di Stato e che si cancella la democrazia. Mi rivolgo alla senatrice Furlan, che non so se adesso sia in Aula. La senatrice Furlan ha fatto un intervento che io credo meriti una risposta, meriti una risposta, perché è persona che io rispetto, per la sua lunga storia di democrazia sindacale popolare, nel senso migliore del termine, che oggi prosegue nel Parlamento. Ora, descrivere, da parte sua, questa riforma come una privazione di potere ai cittadini è un ribaltamento della realtà. Che qualcuno lo dica strumentalmente, lo capisco, ma voglio rispondere con rispetto al suo intervento, perché non è vero. È esattamente il contrario: Giuseppe Conte divenne Presidente del Consiglio portato da un taxi, senza avere avuto il voto di nemmeno un cittadino. Questa non è la democrazia di un Paese! Questa non è la democrazia!

ricorrenza tragica del Paese, la strage di Brescia, uno degli eventi più orrendi del terrorismo del Dopoguerra, perché poi ci sono stati altri eventi. Organizzare le manifestazioni il 2 giugno, mentre c'è la festa della Repubblica, non è rispettoso del Presidente della Repubblica, il quale, anche con questa riforma della Costituzione, avrà più poteri di un re.

potrà avere dei poteri superiori a quelli del Re d'Inghilterra. Che altro dobbiamo fare? La monarchia? Io sono per la Repubblica, sia chiaro, ma sono aperto anche al dibattito sulla monarchia, se necessario. Il Presidente della Repubblica con questa riforma conterà più del re del C'è anche la canzone di Baglioni, visto che citiamo le canzoni. Cari colleghi, non si può stravolgere la realtà. Non ci sarà Letta presidente del Consiglio europeo, che lo fece fuori Renzi. Come era? «Stai sereno». Non ci sarà un altro tecnico commissario europeo, i vertici che rappresenteranno l'Italia li sceglierà la politica democratica che avrà i voti dei cittadini, non le tecnocrazie o i partiti che perdono le elezioni. *(Applausi)*. Capisco che bisogna trovare un posto a Enrico Letta; ce l'aveva il posto, glielo avete tolto voi, mica noi. noi. Credo che noi abbiamo tutto il diritto di andare avanti nella democrazia sostanziale. Questa riforma è un ampliamento della partecipazione dei cittadini che scelgono chi guida il Governo. Il Presidente della Repubblica guiderà il CSM, le Forze armate, scioglierà il Parlamento, farà 1.000 cose. Noi vogliamo rinnovare la Costituzione. In conclusione, Presidente, il Governo che oggi ha proposto finalmente un disegno costituzionale di riforma della giustizia *(Applausi)*, di cui siamo orgogliosi. Rinnoveremo la Costituzione anche nella giustizia e finirà l'uso politico della giustizia, che ha ostacolato la democrazia del Paese. Signor Presidente, prima di esprimere qualche considerazione anche su quello che ha detto ora il collega Gasparri, ci tenevo a stemperare gli animi dopo quello che è successo stamani, leggendo un testo di Trilussa, nostro collega per un periodo come senatore a vita di questo Senato della Repubblica, anche per far capire che i senatori a vita a volte possono essere particolarmente utili. [**Presidenza del impeccabile. «Ner modo de pensà c'è un gran divario: mi' padre è democratico cristiano, e, siccome è impiegato ar Vaticano, tutte le sere recita er rosario; de tre fratelli, Giggi ch'è er più anziano è socialista rivoluzzionario; io invece so' monarchico, ar contrario de Ludovico ch'è repubblicano. Prima de cena liticamo spesso pè via de 'sti princìpi benedetti: chi vo' qua, chi vo' là… Pare un congresso! Famo l'ira de Dio! Ma appena mamma ce dice che so' cotti li spaghetti semo tutti d'accordo ner programma». Oggi, dopo il momento di tensione qui in Aula, ci siamo ritrovati tutti alla mensa del Senato ed era tutto a posto. Mi fa piacere che Trilussa ci abbia azzeccato, questa, come tante altre volte. altre volte. Mi sento di citare brevemente Cicerone che diceva il potere nel popolo e l'autorità nel Senato e ovviamente, per esercitarla questa autorità dovremmo essere anche autorevoli. autorevoli. Il senatore Gasparri faceva riferimento alla nomina di Conte Presidente del Consiglio. Io vorrei ricordare che i Presidenti del Consiglio tecnici sono stati nominati perché l'esito delle elezioni non era tale da garantire la governabilità del Paese, altrimenti sicuramente non si sarebbe fatto. si poteva anche fare un'altra elezione immediatamente successiva a quella precedente, ma forse non è stato neanche male ricorrere al Governo tecnico. In ogni caso, questo è parte della nostra storia e adesso da lì dobbiamo ripartire e costruire. Ecco, il problema è costruire. Cosa vogliamo costruire? Leggo oggi che, secondo i *report* internazionali, il 71 per cento della popolazione mondiale vive in Paesi dove non c'è una sufficiente democrazia secondo i parametri che si è data l'ONU. Allora questa riforma che stiamo proponendo

Vogliamo essere più democratici o no? Qui non è il problema di essere pro o contro, io posso essere pro o contro, ma il discorso è un altro. Cerchiamo di perseguire un risultato che faccia del bene al Paese. È per questo che tale modo di discutere, secondo me, non porta da nessuna parte. Ci sono illustri costituzionalisti che hanno bocciato una serie di cose in questo provvedimento. Altri, ovviamente, l'hanno pensata diversamente, perché i giuristi notoriamente non sono mai tutti dello stesso parere. Quindi, cosa volete che vi dica? Cerchiamo di lavorare e di fare del bene al Paese. Faccio un'ultima citazione che è di Roberto Calderoli, il quale, nel marzo 2007, diceva: sbaglia l'opposizione quando dice che in Senato si lavora poco, sbaglia la maggioranza quando dice che si lavora, la realtà è che il Senato non fa niente. Vorrei smentire l'attuale ministro Calderoli,

Volevo segnalare alla presidente Rossomando, ma a maggior ragione ora che c'è lei lo segnalo a lei, che l'intervento del presidente Gasparri non era certamente sull'emendamento. presidente Gasparri ha fatto un comizio, ovviamente apprezzato dalla maggioranza, ma che noi abbiamo ritenuto assolutamente fuori luogo rispetto all'emendamento. Era un misto di scherno, irrisione, dileggio, sberleffo,

un giudizio o la valutazione; non solo il voto silente (quando è parlante la maggioranza, apprezziamo), ma ci aspettavamo una risposta sulla proposta emendativa che non è arrivata. Sono arrivati insulti di varia maniera, rispetto ai quali, signor Presidente, siccome ne abbiamo discusso nella Conferenza dei Capigruppo, mi consentirà questo intervento sull'ordine dei lavori di farlo anche per una questione personale. Il senatore Menia, giustificando la sua azione, ha pubblicamente detto che è stato il risultato di un atteggiamento o una mia posizione in Aula, che per la verità, non avevo notato, mentre eravamo riuniti qui velocemente, come si fa spesso durante i lavori dell'Aula, con gli altri Presidenti dei Gruppi di opposizione. In quel momento, probabilmente io, a differenza degli altri miei colleghi che avevo di fronte, ero di spalle all'Aula. Succede e mi pare che sia

Siccome noi siamo tornati in Aula, come lei sa, solo dopo aver avuto la sua garanzia - e per questo l'abbiamo ringraziata - di una convocazione del Consiglio di Presidenza che dovrà valutare e noi speriamo sanzionare il comportamento del

è che la menzogna che normalmente è il rifugio della viltà non sia la strada seguita pubblicamente

Questori di fare una relazione, credo che anticipare qualunque valutazione non sia la strada corretta. Pertanto, senatore Menia, se lei vuole, potrà parlare a fine seduta e credo che il senatore Boccia…

Signor Presidente, se abbiamo completato questo passaggio, ci terrei a intervenire perché è giunta adesso notizia che tre militari della Guardia di finanza sono morti in una esercitazione in montagna. Tre giovani militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza in un drammatico incidente avvenuto nel territorio comunale in Val Masino, in provincia di Sondrio. Ritengo pertanto che nei tempi dovuti e nei modi dovuti, signor Presidente, dovremmo trovare il modo per rendere omaggio ai nostri militari. grazie

sull'articolo e sul disegno di legge. Comunque, signor Presidente, io non possiedo la dottrina giuridica e costituzionale di moltissimi colleghi, per cui farò delle osservazioni di carattere generale, come potrebbe fare un uomo o una donna della strada, come direbbero gli inglesi.

che abbiamo presentato hanno l'obiettivo di far comprendere agli italiani le ragioni della nostra contrarietà al presente disegno di legge e, se possibile, instillare alcuni dubbi nella maggioranza, maggioranza, la quale argomenta come l'obiettivo principale di questo disegno di legge sia garantire la stabilità, facendo scegliere ai cittadini il Presidente del Consiglio e legando la durata della legislatura legislatura a quella dell'Esecutivo. È vero che gli italiani potranno scegliere in questo modo direttamente il Presidente del Consiglio, ma a spese del diritto fondamentale che ogni cittadino ha in un Paese democratico, che è quello di controllare l'operato del Governo attraverso i propri eletti. Io credo che gli italiani, oltre a scegliere una volta sola, abbiano il diritto di controllare continuamente l'operato dell'Esecutivo in modo indipendente e senza condizionamenti. Il controllo dell'operato del Governo si esercita in quest'Aula, anche e soprattutto con il voto di fiducia, anche e soprattutto senza vincolo di mandato e attraverso il contributo di persone autorevoli e indipendenti, come i senatori a vita che voi ieri sera - e uso le parole del Governo - avete avuto la premura di eliminare. Abbiamo dimostrato in questo dibattito e in Commissione come questa legge ridimensioni il potere e le prerogative del Presidente della Repubblica, ma il vero obiettivo è ridimensionare e svilire il Parlamento. Questa legge, alterando il rapporto di pesi e contrappesi, limita in modo drammatico l'indipendenza e il potere di controllo del Parlamento.

Ora chiedo, signor Presidente, per vostro tramite, alla ministra Casellati, stando così le cose, perché rimane la necessità di eleggere i membri del Senato e delle Camere. Se ne può fare a meno. In conclusione, l'elezione diretta è una cambiale in bianco, che si chiede ai nostri cittadini di firmare con il loro voto, privandoli dell'unico potere che hanno, attraverso l'indipendenza e l'autonomia del Parlamento, di controllare l'operato del Presidente del Consiglio. Le vittime saranno proprio quei cittadini ai quali Giorgia vuole dare il potere di scegliere; Giorgia da una parte dà una briciola e con l'altra mano toglie il braccio. Voi avete la maggioranza per approvare questa legge, ma gli italiani sapranno scegliere tra quelli che sono i loro diritti e questo imbroglio di nome Giorgia.

Questo emendamento, che descrive con più puntualità come si svolgono le consultazioni, credo faccia parte di alcuni emendamenti che troviamo qua e là nel fascicolo che chiariscono delle prassi che ormai sono parte inveterata della nostra storia repubblicana e costituiscono la cosiddetta Costituzione materiale, ma che sono parte, appunto, di

quando si ragionava della conservazione dell'organo costituzionale delle due Camere e, quindi, di quell'obbligo che gli studiosi ravvedono in capo al Presidente della Repubblica di fare ogni sforzo affinché non si giunga all'evento traumatico della conclusione anticipata della legislatura e, di conseguenza, della chiamata alle urne del corpo elettorale anzitempo. L'emendamento che stavamo discutendo prevedeva l'obbligo in capo al Presidente della Repubblica di spendersi per trovare nuovi Governi e di sciogliere quindi le Camere soltanto davanti all'impossibilità accertata

il frequente ricambio al Governo del Paese e il frequente numero di crisi di Governo, credo che siamo tutti abituati a vedere come funzionano le consultazioni ed anche il grande pubblico sa che normalmente, una volta caduto il Governo - sia perché il Presidente del Consiglio si è dimesso, sia perché, come diciamo nel nostro gergo, è andato sotto in Aula perché non ha ricevuto la fiducia delle Camere - la matassa torna nelle mani matassa torna nelle mani del Presidente della Repubblica. La prima cosa che il Capo dello Stato fa è quella non soltanto di sentire i Presidenti delle Camere,

del momento della composizione del nuovo Governo. Ha senso pensare che, anche nel momento in cui si debbano sciogliere le Camere perché si è verificato che il nuovo Governo non può essere costituito, il Presidente Repubblica allarghi il *parterre* delle alte cariche dello Stato con le quali si consulta e che quindi questo allargamento, questa maggiore consultazione, questo ampliamento delle persone che offriranno il proprio parere e il proprio consiglio al Capo dello Stato possano essere anche i Gruppi parlamentari. Ciò in particolare a seguito di questa riforma costituzionale, dove abbiamo visto che il Parlamento tende a perdere alcuni dei suoi poteri: è un po' una conseguenza dell'elezione dell'elezione del Presidente del Consiglio. Quindi, in ogni occasione nella quale possiamo dare un ruolo aggiuntivo e valorizzare l'esperienza e la rappresentatività delle Camere, penso sia giusto farlo. È per questa ragione che voteremo a favore di questo emendamento.

perché dicono che devono essere consultati i Presidenti delle due Camere e, in questo caso, anche i Presidenti dei Gruppi. Il punto è il seguente: si vuole giustamente cercare di riequilibrare un ruolo del Parlamento, che a nostro avviso con questa riforma non solo viene umiliato, ma viene pressoché annullato. Questo è un primo punto. La questione su cui voglio tornare, in particolar modo perché ho ascoltato gli interventi del relatore, presidente Balboni, è che - proprio come hanno detto più volte il collega De Cristofaro ed altri - qui avremmo dovuto fare una ampia discussione per condividere perlomeno un lessico istituzionale; non le soluzioni, ma un lessico istituzionale condiviso, perché è questo che non è condiviso. condiviso. Ci sono dei punti che meriterebbero un approfondimento. In particolare, sempre per il suo tramite, presidente La Russa, voglio dire al relatore Balboni, che più volte si è appellato alla questione dei senatori eletti, che il problema è il significato che voi date al concetto di «eletto»: lo sganciate completamente dal concetto di rappresentanza e dal ruolo che devono esercitare gli eletti. Se questi eletti infatti

questo: molti di voi hanno l'idea che il voto, senza il concetto di rappresentanza, senza i poteri che si attribuiscono e senza il ruolo del Parlamento, sia esaustivo perché lo agganciate all'elezione del capo, ma allora non c'è bisogno di modificare dieci o

che fosse discusso, perché - com'è stato detto più volte - qui c'è un dramma delle democrazie moderne: tutte le persone che non vanno a votare, perché non si sentono più rappresentate e non credono più in quel in quel voto, costituiscono un problema che ci riguarda tutti o no? Su questo avremmo voluto coinvolgervi e coinvolgerci, poi le soluzioni possono essere diverse. Non c'è però una parola sul ruolo del Parlamento, né sui pesi e i contrappesi. Vi rendete conto che sono anni che si discute

Ci rendiamo conto che ci siamo anche interrogati se ci sono modi diversi, oltre a quello in cui si vota il Parlamento, ancora con qualche funzione, o altri momenti in cui i cittadini possono essere chiamati a votare, per coinvolgerli di più e non di meno? È un discorso che ci riguarda tutti o no? È da anni che si discute del fatto che, avendo introdotto elementi di maggioritarismo, i pesi e i contrappesi della nostra attuale Costituzione, fondati su un sistema proporzionale, probabilmente non sono più efficaci né validi. E voi ci state dicendo che basterebbe una soglia del 40 per cento, su una percentuale già molto limitata di cittadini che vanno al voto. La democrazia, questo concetto, vi interessa davvero o no? Si possono poi discutere molte soluzioni, ma quest'idea plebiscitaria di consegnarsi a un capo che per voi equivale a democrazia meriterebbe veramente una riflessione in più. È per questo che noi insistiamo: oltre ad ascoltarsi, bisognerebbe tenere anche conto delle cose che vengono dette.

Signor Presidente, nell'intervenire questa mattina, la Ministra a un certo punto, esprimendosi contro alcune opinioni che venivano rappresentate dall'opposizione, ha detto che quella era una norma di raccordo. Credo che bisognerebbe ripartire da lì. Dire che quella è una norma di raccordo, in realtà, è una grande conferma delle cose che stava dicendo l'opposizione, e cioè che proprio per determinare particolari poteri del Presidente del Consiglio bisognava intervenire a ridurre quelli del Presidente della Repubblica negli altri capitoli. Convengo, quindi: è una norma di raccordo, che però manifesta ed esprime esattamente il fatto che l'insieme degli interventi che vengono fatti a partire da un tema, che si chiama elezione diretta del Presidente del Consiglio, ha intenzione di individuare la figura di un capo e non del rappresentante democratico di un Governo. Credo che a molti di noi sia successo, nelle loro vite precedenti a quest'Aula, di dirigere organizzazioni: a me è successo di dirigerne una *pro tempore*, ovviamente complessa, perché rappresentava territori diversi, interessi diversi e condizioni differenti. E ci sono certamente dei momenti in cui si pensa che, in fondo, la semplificazione dei modelli di direzione possa diventare un elemento più facile. Più allarghi la platea teorica, più ti pare che ci sia certezza nella tua condizione dell'espressione di un potere. Ma più allarghi quella platea teorica, più eviti di avere rappresentanza. Fai appello magari ai sentimenti o comunque all'idea di venire direttamente riconosciuto, ma in realtà non sei in grado di rappresentare quell'insieme di diversità. È questa la ragione per cui, per definizione, le democrazie si basano sull'esistenza dei Parlamenti e di eletti che sono eletti con caratteristiche di rappresentanza territoriale, di professione, delle tante cose *(Applausi)*. La rappresentanza si esprime così: si esprime innanzitutto dando chi ti rappresenta la possibilità di esercitare un potere effettivo. E allora il nodo è che qui scompare quel potere effettivo. Scompare il potere effettivo del Parlamento di essere rappresentante, anche perché continuiamo a non capire se c'è un modello elettorale che ricostruisce questa relazione con il territorio - ma, se devi eleggere il Parlamento a strascico, sempre meno sarà la possibilità che autonomamente i territori determinino le loro candidature e sempre sempre più ci sarà bisogno di costruirle in funzione del capo - e perché, ovviamente, il Parlamento non sarà messo nelle condizioni di esprimere una sua opinione, ma dovrà dipendere dall'opinione del capo. capo. Il raccordo non è solo questo. Il raccordo è ciò che c'è dentro questo disegno di legge, ma il raccordo è anche gli atti che vediamo intorno a noi, quelli che stiamo vedendo e che si realizzano. Per poter essere un capo, invece che un rappresentante di una plurale democrazia, si ha bisogno anche che non ci siano due cose, i poteri tra loro suddivisi che si bilanciano. Il primo di cui stiamo discutendo è il Presidente della Repubblica, ma in realtà gli annunci avvengono anche rispetto ad altri poteri. Il secondo bisogno che c'è per realizzare questo disegno è evitare che ci sia il diritto di critica. Anche da questo punto di vista, per esempio, vediamo che si decide che agenzie che sono di aziende pubbliche possono diventare di proprietà di un deputato o di un parlamentare e che si reprime il pluralismo dell'informazione. Il nodo è questo qui. Ma il vero problema di questa modalità, che è abolire il potere legislativo del Parlamento e la sua capacità di rappresentanza, è che questo accentuerà

possibile di coloro che vengono eletti? Io credo di no. Allora da questo punto di vista - e chiudo, Presidente - vorrei anche dire che, nella sequenza di affermazioni che abbiamo visto da parte della Presidente del Consiglio sull'importanza o non importanza di questa...

non è interessante, tanto governerò cinque anni. Il che mi fa pensare che non c'è l'obiettivo di dare stabilità al Governo, perché si pensa di averla già, ma si vuole davvero trasformare il nostro da un sistema parlamentare democratico a un sistema...

Anch'io sono nata e cresciuta da slovena e sono orgogliosa di poter rappresentare la mia comunità in quest'Aula. Non ho l'accento straniero, ma posso dire con piacere: *pozdravljeni sopotnik in prijatelji*.

Signor Presidente, i nostri emendamenti puntano a rimediare ad uno scempio che state colpevolmente facendo. Avete deciso di modificare l'articolo 88 della Costituzione. State, in sostanza, decapitando il Capo dello Stato, rendendolo muto, al servizio del principe, di un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, unico caso in Europa. Il vostro disegno di silenziare e, di fatto, decapitare istituzionalmente il Capo dello Stato lo si trova anche nella modifica, che avete apportato in Commissione, del nuovo articolo 3, sulla disciplina del semestre bianco. L'attuale formulazione dell'articolo 88 della nostra Costituzione prevede, infatti, che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del proprio mandato, salvo che essi coincidano, del tutto o in parte, La modifica voluta dal Governo mira, invece, a prevedere che la regola del cosiddetto semestre bianco non si applichi qualora lo scioglimento configuri atto dovuto. Da sempre il potere di scioglimento è stato esercitato dal Presidente della Repubblica in accordo con la maggioranza delle forze politiche. Si tratta, infatti, non di una prerogativa del Presidente, ma di uno dei suoi atti cosiddetti complessi eguali. Nella storia repubblicana si è fatto dunque ricorso allo scioglimento anticipato solo quando, a seguito delle interlocuzioni tra il Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, risultasse evidente l'impossibilità di formare il nuovo Governo. Tale potere, esercitato con equilibrio nel raccordo tra Presidente della Repubblica e forze politiche, rappresenta uno dei più importanti fattori di indirizzo e gestione delle crisi politiche. Noi contestiamo alla radice il vostro impianto di riforma e i nostri emendamenti hanno l'obiettivo di razionalizzare il potere del Capo dello Stato di sciogliere le Camere, chiarendone i presupposti, senza tuttavia svilirlo e, soprattutto, senza subordinarlo rigidamente alle dinamiche del rapporto fiduciario e, quindi, senza far venir meno la necessaria flessibilità, fisiologica in una forma di Governo parlamentare: quindi - lo ribadisco - in un contesto di ferma e convinta contrarietà alla proposta di revisione della Costituzione presentata dal Governo Meloni. Gli emendamenti di cui sono prima firmataria, in relazione all'articolo 88 della Costituzione, prevedono che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere quando sia acclarata, a seguito di consultazioni delle forze politiche, l'impossibilità di formare un nuovo Governo in grado di ottenere la fiducia. Inoltre, essi prevedono che che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere quando, entro un certo termine, a partire dall'espressione della sfiducia al Governo o dalle dimissioni del Governo stesso, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo. Infine, questi emendamenti prevedono che il Presidente della Repubblica possa o debba sciogliere le Camere quando sono le Camere stesse a chiederlo, approvando una mozione in tal senso, con previsione di varie maggioranze. Ecco, quindi, spiegata la *ratio* degli emendamenti a mia prima firma, che definisce come l'articolo 88 della Costituzione preveda che lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta, con mozione approvata a maggioranza dei due terzi. chiediamo, in caso di scioglimento, che siano coinvolti e sentiti, non solo i Presidenti delle due Camere, ma anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e gli ex Presidenti della Repubblica. Voglio ribadire che state commettendo un pericoloso sbrego istituzionale. La Carta costituzionale sicuramente non è immodificabile, ma quello che state per fare voi la dileggia e la colpisce al cuore.

che mi pare colga lo spirito di un punto abbastanza essenziale, che va esattamente nell'ottica della comprensione in una situazione come questa. Lo ripeterò nuovamente, e non mi stanco di dirlo, che dinanzi a questo stravolgimento della Costituzione - secondo me - è bene ricordare davvero a chiunque ci dovesse ascoltare che, di fronte alla situazione di crisi con la quale conviviamo, la strada che è stata in qualche modo scelta - come diceva anche la senatrice Camusso molto efficacemente nel suo intervento qualche minuto fa

e in qualche modo riguarda lo stato di difficoltà in cui versano le democrazie occidentali più in generale e, in particolare, la democrazia italiana. Dinanzi Dinanzi a tale stato invece di ragionare, nella migliore delle ipotesi comunemente, su quali strumenti poter immaginare per introdurre degli elementi capaci di incrinare

qualche elemento di densità in più rispetto alla crisi che si è consumata in particolare nel corso degli ultimi decenni, si è scelta la strada della semplificazione. Come avviene la semplificazione? Riducendo ancora di più la centralità del Parlamento; processo che va avanti da molti anni e io su questo ho sufficiente onestà intellettuale per dire che non è certamente legato a questa riforma il processo di svilimento e di perdita di centralità politica, politica, che ha riguardato tre decenni di storia italiana. Ricordo che esso ha riguardato purtroppo un pensiero unico; il vero tema attorno al quale noi avremmo dovuto sviluppare una discussione, altro che la propaganda. Avremmo dovuto ragionare se l'indirizzo politico culturale egemone degli ultimi trenta anni, non semplicemente in questo Paese, finalizzato a portare avanti la tesi che tutto dovesse svilupparsi attorno al valore della stabilità, abbia portato con sé un miglioramento della nostra democrazia. Purtroppo penso di no. Penso che questa tesi, che è stata largamente egemone nel Paese e non è figlia semplicemente di questa riforma, avrebbe meritato qui un elemento di approfondimento reale. Penso che la risposta che viene data sia totalmente semplificata e francamente fa anche un po' impressione, anche pensando alla storia di questo Paese. di questo Paese. L'uomo forte al comando ce l'abbiamo avuto in una fase storica ben precisa, come sappiamo. Però poi successe che, quando l'uomo forte al potere cadde...

al posto dell'uomo forte arrivò il Comitato di liberazione nazionale. Il capo del Comitato di liberazione nazionale, differentemente dall'uomo forte, lo sapete che cosa era? Era un *primus inter pares* - guarda caso - la Costituzione italiana, quella che voi andate a modificare, immagina la figura del Presidente del Consiglio, quella che noi abbiamo avuto in tutti questi anni, un *primus inter pares*

del CLN e mi pare una cosa altrettanto negativa passare dal *primus inter pares* che ha segnato la storia democratica di questi decenni, al ritorno dell'uomo forte. Molto, molto negativa.

Stiamo ragionando intorno all'articolo 3, già articolo 2 del disegno di legge. Questo articolo 3, in realtà, soprattutto nel suo secondo comma che noi abbiamo modificato con un emendamento in Commissione, sistematicamente si collega all'articolo 7. Quindi, forse avrebbe avuto più logica coniugare il dibattito all'articolo 7. Infatti, tutti i colleghi stanno intervenendo in realtà non su questo articolo, ma sul tema che richiama l'articolo 7, e cioè sulla possibilità del *Premier* eletto di determinare lo scioglimento delle Camere, non esercitando la facoltà di consentire il passaggio ad un secondo *Premier*. In sostanza, con la modifica che abbiamo approvato in Commissione, abbiamo risposto, signor Presidente, a molte critiche che ci erano state rivolte proprio dall'opposizione, che lamentava come nel testo originario del disegno di legge il Presidente del Consiglio subentrante paradossalmente potesse avere più poteri del Presidente del Consiglio eletto; non ci poteva essere un terzo incarico e quindi davvero il *Premier* subentrante avrebbe - lui sì - potuto determinare *ad nutum* lo scioglimento delle Camere. Abbiamo recepito le osservazioni delle opposizioni e abbiamo modificato il testo; nel testo originario l'ultima parola spetta in capo

Adesso di cosa stiamo discutendo, cari colleghi? Stiamo discutendo di un potere che la Costituzione italiana vigente non concede al Presidente della Repubblica, perché il secondo comma dell'articolo 88 vigente dice che il Presidente della Repubblica non può esercitare la facoltà di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Quindi, questa è una limitazione che la nostra Costituzione impone al Presidente della Repubblica:

i Costituenti hanno inteso negare questo potere negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica? Hanno inteso evitare che il Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del suo mandato potesse sciogliere le Camere, perché evidentemente, di lì a poco, ci sarebbe stata l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e, quindi, i Costituenti volevano evitare che il Presidente della Repubblica, attraverso quest'arma, potesse influenzare il futuro Parlamento. Mi sembra evidente che sia questo il motivo. E infatti, c'è la clausola finale nella Costituzione vigente che recita «salvo che gli ultimi sei mesi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura». Quindi, questa è un'eccezione dell'eccezione: il Presidente della Repubblica potrà sciogliere le Camere anche negli ultimi sei mesi del suo mandato, se chiaramente le Camere stavano comunque per concludere la legislatura. Qual è la modifica che noi introduciamo? La modifica che noi introduciamo è molto semplice. Consentiamo in ogni caso che che lo scioglimento avvenga anche negli ultimi sei mesi del mandato, in seguito a ciò che approveremo con l'articolo 7, sarà un atto dovuto. Sarà un atto dovuto quando, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 che noi voteremo, sarà votata una mozione di sfiducia motivata al Governo in carica, oppure, ai sensi del secondo comma, quando il *Premier* si sarà dimesso e quindi non avrà esercitato la possibilità di consentire il passaggio ad un secondo *Premier.* Pertanto, in realtà non ci si priva di nessun potere, di nessuna prerogativa rispetto a ciò che oggi già avviene in relazione all'articolo 88 della Costituzione. Dico questo per riassumere la questione di cui stiamo discutendo. Mi rendo conto benissimo concluda.

l'autorevole ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e limita i poteri e la sovranità del Parlamento, come hanno detto meglio di me i miei colleghi. Presidente, con i nostri emendamenti abbiamo invece cercato di mantenere intatta e non incarcerata in rapporti di potere sbilanciati l'alta prerogativa costituzionale facente capo al Presidente della Repubblica, oltre a quella che abbiamo già discusso in questi giorni riguardo alla nomina dei senatori a vita. Sto parlando della Sto parlando della facoltà di scioglimento delle Camere. Ci interessa in particolar modo ribadire la centralità del Capo dello Stato che, con la riforma in esame, perderebbe la capacità di influire sulla situazione politica, anche in caso di stallo e crisi di Governo, date le rigidità previste, rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere in alcuni casi. Così facendo si crea un'ulteriore situazione di subalternità del Capo dello Stato rispetto al Presidente del Consiglio, il quale, dimettendosi, potrebbe persino decidere di determinare lo scioglimento delle Camere, in modo da indirizzare l'elezione di un Presidente della Repubblica a lui o a lei gradito. Sarebbe un ribaltone di diversa natura rispetto a quello che continuamente citano gli esponenti dell'Esecutivo, ma sempre

del Presidente della Repubblica, al contrario di quanto ci raccontano da mesi. Questa volontà, finora malamente dissimulata, finisce per danneggiare proprio il Parlamento, depauperandolo ulteriormente delle sue funzioni e poteri. Con gli emendamenti all'articolo 3 riteniamo debba essere rimessa alle Camere e ai suoi rappresentanti la responsabilità di verificare se sia possibile superare una crisi e formare un nuovo Governo, restando all'interno dello stesso Parlamento. Nella nostra Repubblica, signor Presidente, è il Parlamento il luogo in cui si costruiscono o annullano le maggioranze e dobbiamo scongiurare a tutti i costi una verticalizzazione della democrazia rappresentativa, impedendo che il legislatore prosegua nella preoccupante direzione in cui sembra essere avviato, ovvero ridursi ad una svilita appendice dell'Esecutivo. Peggiorerebbe, infatti, quello che appare come un problematico impoverimento della capacità politica e riduzione della partecipazione democratica. È il Parlamento, signor Presidente, a farsi veicolo della sovranità popolare, proprio perché è o quantomeno dovrebbe essere rappresentante della pluralità della componente maggioritaria e delle minoranze. Al Parlamento, dunque, vanno dati sostegno e fiducia nel provare a risolvere al suo interno le crisi di Governo e questo può avvenire solo non spostando *de facto* la facoltà di scioglimento delle Camere perché di questo si tratta nella pratica - nelle mani del famoso uomo solo al potere, costringendo il Presidente della Repubblica, figura garante della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni per il bene comune dello Stato, al ruolo di mero segretario. Davvero si vuole nascondere l'importanza che hanno avuto i Presidenti della Repubblica nella nostra storia repubblicana? Ogni Presidente della Repubblica è stato essenziale per la tenuta del nostro Paese come lo è stata la sua credibilità internazionale anche nei momenti più difficili della nostra storia moderna e non può essere sminuito nella sua funzione in virtù di una riforma che nulla ha di compatibile con la volontà dei nostri Padri e Madri costituenti e con i bisogni del Paese.

per una facoltà in più che viene concessa al Presidente della Repubblica il fatto che gli si imponga, in un periodo in cui non potrebbe farlo, di sciogliere le Camere. Questa non è una facoltà, non c'è nessuna discrezione. Si sta semplicemente dicendo che il Presidente della Repubblica,

Facciamo allora una riflessione sull'uso delle parole, perché le parole sono atti creativi, hanno un grande potenziale creativo, possono possono descrivere mondi reali e renderli più belli, ma possono anche diventare manipolatorie, possono trasformare un terreno abbandonato nel giardino segreto del sultano, che non è quello che vogliono i cittadini. Quello che voi state narrando, le parole che state utilizzando anche in questo provvedimento nascondono un inganno, non dicono la verità. Vi faccio un esempio: prendete la parola «rappresentatività». Sapete dove la state utilizzando? La state utilizzando in quell'articolo di questa vostra riforma, di questa madre di tutte le riforme, in cui si va addirittura a distorcere la rappresentatività. Ebbene, usate l'espressione «rispetto della rappresentatività» quando inserite nella Costituzione un premio di maggioranza che sta a significare che governerà una minoranza che ha vinto il premio per aver raggiunto non si sa quale minimo. Per inciso, avete inserito un premio di maggioranza senza indicarne dato che c'è questa tendenza a usare parole che dicono una cosa diversa dalle intenzioni, perché mai dovremmo fidarci di questa maggioranza? Ancora ad oggi non sappiamo né quale sia la condizione minima

come avvenne ai tempi di Mussolini con la legge Acerbo? Non lo sappiamo, ma non ci fidiamo di chi continua oggi a usare *slogan* per dire che, tutto sommato, si tratta solo di far eleggere ai cittadini il *Premier.* Questa è e continua ad essere una menzogna. C'è una perseveranza nel mentire, perché non si mente soltanto dicendo una cosa diversa dalla realtà, ma la menzogna esiste anche quando si nasconde una parte della realtà; se si presenta a un magistrato la copia di un contratto al quale sono state tolte tre pagine, si sta commettendo comunque un falso,

chiedere, facendo appello al potere del Presidente della Repubblica, di esercitare un suo potere. Qui sta l'inganno, perché il Presidente della Repubblica non ha nessun potere se non quello di mettere un timbro notarile.

si inserisce nel solco di una serie di proposte che, come Gruppo Italia Viva, abbiamo fatto per cercare di dare coerenza all'impianto che è stato presentato dal Governo. Per la verità questo è un elemento del tutto basilare, perché, sia pure nella connessione fra l'articolo 3 e l'articolo 7 di questo disegno di legge a cui faceva riferimento in precedenza anche il relatore, ci pare opportuno dover precisare, in sede di esame dell'articolo 3, che debba valere, qualora questo tipo di impianto dovesse diventare norma, un principio sintetizzato dall'antico brocardo latino *simul stabunt vel simul cadent*. di un elemento abbastanza pleonastico, ma purtroppo in questa circostanza siamo invece costretti a doverlo ribadire: insieme staranno oppure insieme cadranno. Se si ritiene che il Capo del Governo venga eletto insieme al Parlamento e quindi vi sia un unico mandato imperativo del corpo elettorale a due livelli diversi (l'esecutivo e il legislativo), essendo, nel quadro del potere democratico e dell'equilibrio del potere, nella facoltà del legislativo mandare a casa l'Esecutivo, nel momento in cui questo dovesse avvenire bisogna per forza di cose tornare alla fonte primigenia originaria da cui è scaturito questo mandato, e cioè il corpo elettorale. Questo peraltro avviene esattamente in tutti i sistemi in cui vige il mandato dell'elezione diretta del capo di un Esecutivo. Senza andare troppo fuori e per non peccare di provincialismo, vorrei ricordare che questo principio tutte le forze politiche lo hanno assodato e cristallizzato in termini positivi quando si è trattato di introdurre il meccanismo che ha visto gli enti locali e le Regioni passare dall'elezione indiretta all'elezione diretta dei capi dell'Esecutivo. In tali casi vige esattamente questo tipo di equilibrio. Peraltro, suggerirei alla maggioranza di studiare con attenzione un precedente di espressione della Corte costituzionale che, esattamente partendo dall'affermazione del principio che sto cercando di illustrare, ebbe modo di censurare la legge della Regione Calabria - cito la sentenza costituzionale n. 2 del 2004 che introduceva, come si sta facendo in questo caso, l'elemento surrettizio del Vice Presidente come elemento di permanenza e di continuità dell'attività dell'organismo legislativo. In questo caso, quindi, sarebbe bene anche porre una grande attenzione a quello che si sta facendo. Quindi dire, come proponiamo noi nel nostro emendamento, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere significa affermare questo principio, che ieri è stato è stato affermato in maniera molto puntuale e precisa in questa sede dal senatore Renzi, il quale ha sottolineato come questo sia uno degli elementi della

e si è preoccupato di questi aspetti. Noi vorremmo dire che capiamo la preoccupazione del senatore Gasparri, visto che nei sondaggi il suo partito sta scendendo mentre Stati Uniti d'Europa sta salendo. Quanto invece al fatto di scappare, presidente Gasparri, vedremo cosa farà lei, quando il presidente Renzi la aspetterà in tribunale per gli insulti che gli ha rivolto in quest'Aula in una seduta di dicembre 2023.

L'attuale formulazione di questo articolo rappresenta due cose: in primo luogo, raccoglie le osservazioni che sono giunte da molti costituzionalisti nelle audizioni della 1a Commissione.

molti costituzionalisti hanno osservato come il sistema che era stato proposto fosse eccessivamente rigido, oltre alle osservazioni che ha ben rappresentato ben rappresentato prima di me il relatore Balboni rispetto all'ipotesi che il cosiddetto secondo *Premier* avesse potere o facoltà superiori al primo *Premier.*

solo l'ipotesi della decadenza, delineava una rigidità sistemica che alcuni osservatori e alcuni costituzionalisti, anche auditi,

che l'attuale formulazione è proprio frutto della raccolta dei suggerimenti che sono arrivati in sede di Commissione, che hanno portato a una modifica che a nostro avviso avviso crea il giusto equilibrio e la giusta elasticità di sistema per consentire al

Questo in realtà va proprio nella direzione che molti auspicavano, di tutelare comunque la legislatura, salvare in parte la rappresentatività del Parlamento e, nello stesso tempo, garantire quella stabilità che in alcuni casi potrebbe realizzarsi. Come ci hanno ricordato i costituzionalisti, infatti, dev'esserci una necessaria elasticità di sistema nella gestione delle crisi. Crediamo che questo sia il giusto compromesso e rappresenti il giusto equilibrio tra le esigenze di tutelare il Parlamento, la stabilità dell'Esecutivo e i poteri del Presidente della Repubblica.

Signora Presidente, mi rivolgo a lei perché vorrei rispondere, in questa discussione, a quello che ho sentito prima. Sarò un po' duro di comprendonio, però ascolto molto attentamente, in particolare quando il presidente Balboni risponde alle argomentazioni di altri, e cerco di capire. Devo dire che il suo intervento ha confermato *in toto* quello che diceva il presidente del mio Gruppo, cioè, in sostanza, che siamo di fronte al fatto che non è vero quello che lui afferma; in sostanza, non è vero che non si modificano i poteri.

eletto, il che vuol dire che, in sostanza, diamo tutto il potere in mano a una singola persona. Giustamente il senatore Peppe De Cristofaro cercava di spiegare che l'esperienza che abbiamo avuto nel nostro Paese in tal senso non è stata il massimo della democrazia e della partecipazione democratica; anzi, è stata esattamente il contrario.

di una sola persona. Questa discussione non è una questione solo parlamentare. Potremmo fare una discussione più ampia, anche nella società.

per trovare la sintesi, meno si è e meglio è. La democrazia è una cosa complicata e complessa; vuol dire capacità di ascolto, vuol dire modificare le proprie opinioni, vuol dire far partecipare la società. Questo è il dato fondamentale della democrazia. Quello che noi vogliamo difendere è questo principio, non è un'altra cosa. Questo è il dato fondamentale. Se una riforma va in questa direzione, siamo disponibili a discutere; se va in modo contrario, ovviamente abbiamo una contrarietà

sala, ve lo spiegherebbe lui cosa vuol dire questa discussione, che vale in questo Paese, ma vale anche in altri Paesi. Insisto su questo terreno. Ho detto prima questo rischio non c'è solo sul terreno della politica, in Parlamento, ma c'è anche nella società civile. Anche nelle organizzazioni di massa molto spesso si pensa di semplificare le decisioni; le decisioni; sempre di più si va tendenzialmente verso l'uomo solo al comando. E capite bene - e voi lo sapete benissimo, perché lo proviamo tutti sulla nostra pelle - che il livello di partecipazione diventa sempre minore, perché, quando i cittadini sono chiamati solo a ratificare e non a partecipare alla costruzione, sono un elettorato passivo e quindi si distaccano dalla partecipazione. Questa è la nostra preoccupazione

davvero uno sguardo alla sfilza di costituzionalisti che sono venuti in audizione presso la Commissione affari costituzionali su questa modifica costituzionale. Sono quasi una cinquantina. È stato affermato che tanti costituzionalisti hanno ritenuto di darci questo suggerimento, lasciando quasi ad intendere che, quindi, i costituzionalisti fossero d'accordo con questa riforma e che questa avesse soltanto bisogno di alcuni piccoli aggiustamenti. Ma qui c'è una manipolazione palese della realtà e, di conseguenza, la necessità di difendere l'onore e il buon nome dei costituzionalisti. È noto che tutti loro si sono espressi in maniera maniera strenuamente contraria, nel merito e nel metodo, a questa riforma. Ve l'hanno detto in tutte le lingue che i costituzionalisti possono adottare: una lingua tecnica, una lingua alta, una lingua da costituzionalista, che a voi evidentemente risulta incomprensibile e i risultati si vedono. Cosa vi hanno detto i costituzionalisti? Vi hanno fatto notare che, nella prima versione del testo che avevate sottoposto alla Commissione, ciò che voi volevate prefiggervi come obiettivo primario, ossia l'inamovibilità di questo Presidente del Consiglio eletto, che non poteva essere spostato a meno di casi eccezionali, in realtà era un punto

potente di quello eletto dal popolo. Questo non significa che essi fossero d'accordo: che Cheli fosse d'accordo, che Azzariti fosse d'accordo, che De Siervo fosse d'accordo, che Calvano fosse d'accordo. Tutti i cinquantadue

che sono intervenuti. L'articolo che stiamo votando è soltanto il frutto della correzione che avete dovuto apportare una volta che vi siete resi conto di questo errore macroscopico, che per sciatteria e grossolanità avevate avevate inserito nel testo. Pertanto, tutta questa polemica mi sembra davvero assolutamente inutile. La realtà dei fatti è che voi state marciando a tappe forzate. Ribadisco la nostra assoluta contrarietà alla mordacchia che utilizzate, tanto per dimostrare quanto avete a cuore la democrazia; avete messo la mordacchia alle opposizioni, imponendo tempi strettissimi di discussione: due ore scarse. Aggiungo che vorrei sapere quanto tempo è rimasto ancora al mio Gruppo. Quindi, chiedo davvero ai colleghi quantomeno di non mentire sul conto dei costituzionalisti che sono intervenuti in Commissione a dare il loro contributo.

Signora Presidente, questo mio intervento ha lo scopo di illustrare il complesso di emendamenti a mia prima firma e l'emendamento della collega d'Elia presentati all'articolo 3 del disegno di legge in discussione, che regola le prerogative di scioglimento delle Camere nel semestre bianco del Presidente della Repubblica. Prima di iniziare con l'illustrazione, Presidente, faccio una brevissima premessa, solo per ribadire ancora una volta come questa riforma sia un tentativo disperato d'intesa elettorale tra la Lega e Fratelli d'Italia per il sostegno reciproco a due provvedimenti bandiera: l'autonomia differenziata per la prima e il premierato per la seconda. Mi viene in mente una celebre frase di Ennio Flaiano, che recita: la situazione politica italiana è grave ma non è seria. in altre circostanze avremmo gioito come forza d'opposizione dell'attuale stato di confusione in cui vive la maggioranza, ma non possiamo permettercelo oggi. Qui si sta parlando infatti della modifica della Costituzione italiana e del ruolo di garante di garante del Presidente della Repubblica. Vengo rapidamente al merito della questione. e, per il suo tramite, colleghi della maggioranza, il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 3 mira a rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento che la Costituzione riconosce ai partiti politici. L'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare, come è già stato detto più volte, più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione. In questo scenario la figura del Presidente della Repubblica resta l'unica a poter garantire il giusto rispetto dei dettami costituzionali. Uno degli emendamenti a mia prima firma ha l'obiettivo di coinvolgere nelle consultazioni del Presidente della Repubblica per l'eventuale scioglimento anticipato delle Camere anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica. In uno scenario nel quale il Parlamento diventa diretta espressione del Presidente del Consiglio in carica, il rafforzamento delle prerogative del Presidente della Repubblica nello scioglimento delle Camere è un elemento chiave, una priorità assoluta del Gruppo Partito Democratico. Mi permetta poi di sottolineare, Presidente, come le comunità degli italiani all'estero, che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, vengano ancora una volta messe in secondo piano. Le parole, riprese in un editoriale la ministra Casellati affronta la questione del voto degli italiani all'estero, dimostrano il totale disinteresse e la scarsa considerazione che questo Governo ha per gli ormai 7.000.000 di cittadini italiani che vivono fuori dai confini nazionali. La Ministra afferma che la questione del voto degli italiani all'estero verrà affrontata nella legge elettorale e non nella riforma costituzionale, arrivando quindi all'incongruenza evidente di non avere la corretta copertura costituzionale, come segnalato di recente dal costituzionalista di lungo corso Stefano Ceccanti. Abbiamo più volte evidenziato, come d'altra parte ha fatto anche parte della maggioranza, cioè la la Lega, la necessità di conoscere e di esaminare insieme la legge elettorale per fugare i dubbi di illegittimità che abbiamo e temiamo, ma la ministra Casellati ci ha confermato che la scopriremo solo dopo aver votato in prima lettura il premierato. Continuare ad ostinarsi in questo modo è un altro sintomo della confusione e della superficialità nell'approccio della maggioranza ad una riforma così importante. Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, ricordando all'Aula e a chi ci ascolta da casa che questo disegno di legge è il capriccio di un Governo che ha un unico obiettivo: ridurre la la partecipazione democratica. Tutti gli sforzi che il Gruppo PD sta portando avanti attraverso il lavoro di approfondimento fatto e le proposte avanzate vanno esattamente nella direzione opposta. Noi, come Partito Democratico, abbiamo sempre messo al al primo posto la Carta costituzionale e la tutela dei diritti in essa sanciti. Respingiamo dunque convintamente il vostro tentativo di snaturare il Parlamento e il ruolo dei rappresentanti delle istituzioni. Grazie, senatrice La Marca. Voglio approfittare di questo suo intervento per congratularmi con lei per la laurea *honoris causa* che le è stata conferita in *humane letters*.

la nostra convinzione circa la scelleratezza di questa riforma. Infatti, signora Presidente, emerge in maniera sempre più chiara la scarsa cultura costituzionale che possiede questa maggioranza, perché non può essere diversamente se si insiste nel dire che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, o, che l'attività parlamentare non viene limitata; se si insiste nel dire questo e se si insiste nel fare il gioco delle tre carte, che evidentemente piace tanto, per nascondere un chiaro e palese stravolgimento di quella che è l'architettura istituzionale. A pensare questo, signor Presidente, non siamo solo noi. Addirittura il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Zuppi, si è pronunciato in questo senso. Vi vado a leggere le sue dichiarazioni: «quando si toccano gli equilibri istituzionali» è necessaria «molta attenzione», preoccupazione che sembra non avere sfiorato minimamente questo Governo. Il cardinale ancora ha sottolineato che «occorre molto spirito della Costituzione» e qui mi ricollego a quello spirito, a quella cultura costituzionale di cui sopra. Quindi, occorre molto spirito della Costituzione, che «non è un problema di lettera ma di capacità di pensare qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte», «questo è indispensabile». Ma a voi sembra normale che sia un uomo di chiesa ad intervenire per farvi capire cosa significa spirito costituzionale? Tutto questo, anzi anche questo è sconcertante, Presidente; quindi ogni tentativo utile per raddrizzare questa riforma che si sta mostrando sempre più storta,

perché consentono agli avversari politici di guardarsi in faccia, di vedere le rispettive reazioni e di guardarsi negli occhi. E davvero queste giornate di dibattito per noi sono state un po' spettacolari, perché guardando i vostri banchi

Parlo di voi, non perché dimentichi i nostri problemi, ma perché vorrei fare brevemente un ragionamento, perché il tema ci riguarda tutti. Le coalizioni in questo Paese devono essere una scelta o una costrizione? Non Non devono essere una costrizione sotto il partito più forte del momento; le coalizioni devono rappresentare forze politiche che rappresentano delle diversità. In questo momento Forza Italia ha un *trend* positivo nei sondaggi,

quale ragione. Se la ragione è quella che pare di leggere soprattutto dalla giornata di oggi, in cui contemporaneamente il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere e la Camera approva la questione pregiudiziale sull'autonomia differenziata; se il tema, cioè, è lo scambio,

e Berlusconi prima e Salvini poi erano al di sopra il 30 per cento. Vi avrebbero mai concesso in quel momento di fare una riforma di questo tipo, consegnandosi nelle mani del partito più forte della coalizione? Fratelli d'Italia avrebbe mai concesso a Berlusconi o Salvini una riforma di questo tipo? Perché state facendo questo?

e la prosecuzione della vita delle coalizioni e dei Governi, un conto è costruire una gabbia in cui poi imprigionarsi dentro e le cui chiavi appartengono soltanto a chi la guida, a chi comanda in quel momento.

Alla presidente del Consiglio Meloni, che vedo molto impegnata in campagna elettorale, vorrei dire che, anziché parlare e invocare maggiori poteri per il Presidente del Consiglio, provi a usare quelli che ha, che non sono pochi; si dimostri capace di usare quelli che ha per affrontare i problemi degli italiani e governare questo Paese, che sono più che sufficienti. Presidente, gli inviti alla riflessione che vengono da esponenti che hanno un'esperienza politica solida vanno rispettati e ascoltati, quindi la mia risposta non è né di insulto né beffarda. Prima sentivo addirittura parlare di querele per il dicembre 2023; non so se siamo stati querelati per avere condiviso, ad esempio, le posizioni di Renzi nel conflitto di attribuzione, perché quando uno ha ragione noi la diamo perfino a Renzi; forse abbiamo sbagliato, dovremmo essere meno generosi. Dico questo tanto per ricordare la storia parlamentare. Per quanto riguarda il merito della vicenda, non c'è nessuno scambio. Forse qualcuno è rimasto distratto negli ultimi trent'anni. Il presidente Berlusconi, sull'elezione diretta del *Premier,* sul presidenzialismo, su una formula di democrazia diretta ha fondato la sua storia politica, purtroppo inappagata sotto questo profilo. Non sto qui adesso a ricordare le riforme. Anche noi abbiamo approvato una riforma della Costituzione che non vinse il *referendum* confermativo. Un'altra l'ha approvata la sinistra, sulla quale Renzi si è giocato la sua gloria e la sua carriera politica.

neoeletti, è un fatto positivo e quindi non sono abituati a questi riti. Ho visto riti ostruzionistici della sinistra tante di quelle volte che poi la sinistra pretenda che io abbia anche una faccia baldanzosa; se volete, faccio la faccia baldanzosa quando fate ostruzionismo, ma capisco chi è più nuovo a questi riti. Io non sono affatto rassegnato, anzi sono presidenzialista - lo abbiamo detto più volte - anzi in una maniera ancora più piena, vorrei poteri ancora più ampi, ma il premierato è già un punto di equilibrio, quindi non c'è alcuno scambio. Fornirò ai colleghi che ci fanno queste domande copie dei programmi

chiaro che la Lega vuole l'autonomia, è un fatto identitario che poi il centrodestra ha condiviso, perché abbiamo fatto un'alleanza. Siamo stati alleati con la Lega nel 1994, poi ci fu un periodo di divergenze e l'alleanza si è riformata nel 1999; sono venticinque siamo alleati, che abbiamo vinto e perso elezioni, che abbiamo formato Governi nazionali, che governiamo Regioni sempre più numerose grazie agli elettori e quindi siamo alleati e sappiamo che la Lega sui temi dei territori ha una particolare attenzione e priorità: non è un mistero. che tiene molto all'elezione diretta del *Premier* o addirittura avrebbe voluto del Presidente della Repubblica, sui temi della giustizia ha anticipato molti altri (c'è qui il vice ministro Sisto, che ha partecipato

saranno scelti con sorteggio, le correnti lottizzate non saranno padrone delle nomine delle procure della Repubblica; questa è la ragione dello sciopero annunciato. annunciato. Sono baldanzosissimo, voglio rassicurare la Presidenza, ma anche il collega Franceschini sa il rispetto che porto per la sua persona. Dopodiché noi siamo a favore, sì, dell'elezione diretta della carica apicale di Governo da molto tempo, ma su questo fornirò documentazione così potrà essere più sereno.

semplicemente di attuare il programma di Governo. Ve l'ho già detto in sede di discussione generale, ma forse siccome la discussione generale si svolgeva con l'Aula più vuota di quanto sia ora, non mi avete giustamente ascoltato e quindi ve lo ripeto. Qui non si contesta il fatto che il premierato e l'autonomia differenziata fossero entrambi nel programma, perché lo sappiamo che erano entrambi nel programma, ho letto il vostro programma e so che era così. Qui si contesta che il premierato e l'autonomia differenziata erano entrambe nel programma nonostante si fondassero su due concetti totalmente antitetici, che sono, quelli sì, figli di uno scambio politico. Come si può negare questo elemento? Fratelli d'Italia fino a qualche anno fa presentava disegni di legge che volevano abolire le Regioni e consideravano la riforma del Titolo V del 2001 una violenza nei confronti della Costituzione repubblicana: basta andare a vedere i Resoconti dell'epoca. Questa è la cosa che si contesta oggi: pur essendo vero che queste due cose sono contenute nel programma di Governo, si fondano però su due logiche politiche totalmente incompatibili. Non c'è niente da fare, la potete raccontare come volete, ma se una di queste due riforme, il premierato, accentra totalmente i poteri nelle mani del Primo Ministro che verrà, mentre l'altra, l'autonomia differenziata, li decentra al punto tale che quello stesso Primo Ministro con i poteri accentrati non potrà legiferare, per esempio, su scuola o sanità perché decideranno tutto i Presidenti delle Regioni, ci spiegate una volta per tutte questo vostro programma di Governo su questo punto di fondo come si terrà assieme? Come si fa a non vedere che questo è esattamente figlio

sarà ingigantito da questa riforma che state proponendo. Non c'è niente da fare, delle due l'una. In una prima ipotesi avremo tre, quattro, cinque candidati *Premier* rappresentativi di tante coalizioni diverse e quindi non ci sarà il bipolarismo coatto. A quel punto, succederà molto banalmente che chi prende più voti, siccome deve diventare Presidente del Consiglio e lo diventa sulla base dell'articolo della Costituzione modificato che dice che gli dovrà essere garantita la maggioranza dei seggi, prenderà un premio di maggioranza totalmente spropositato. Quindi senza bipolarismo coatto vi sarà un premio di maggioranza totalmente sproporzionato. Nell'altro caso, invece, succederà esattamente quello di cui stiamo discutendo, cioè che il bipolarismo coatto sarà determinato non da una libera scelta, libera scelta, ma esattamente dalla necessità di dover vincere le elezioni, e questo penso determinerà un danno molto grave al nostro Paese. Se già oggi ne vediamo le conseguenze più evidenti e se già oggi vediamo tutti i limiti del sistema, immaginatevi cosa potrebbe succedere con questo tipo di meccanismo. Io non sono nemmeno contro il bipolarismo; credo che sia anche una cosa di cui dobbiamo discutere seriamente e penso che abbia portato anche qualche elemento di giovamento al Paese, purché però il bipolarismo sia figlio di un processo storico. Se il bipolarismo invece è la tanto discussa e famosa fusione a freddo (alla fine questo è), allora porta solo danni e nessun giovamento. La situazione di oggi, già

guardiamo ai fatti. Lei ha votato per il conflitto di attribuzioni perché c'era, mentre noi abbiamo votato per proteggerla da un'iniziativa propagandistica infondata, cioè priva di qualsiasi fondamento almeno apparente quando si trattava di lei. Secondo me, è giusto che noi interpretiamo questo ruolo nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, perché siamo chiamati a far quello e non a dare voti politici. Quindi questo, evidentemente, ci accomuna. Torno Torno su un punto sollevato dal collega De Cristofaro, come al solito molto correttamente, e cioè che alla fine noi abbiamo una responsabilità, quella di consegnare a questo Paese istituzioni meglio funzionanti di quelle che abbiamo oggi. Il tema è che oggi le istituzioni non funzionano e hanno problemi di funzionamento molto seri, è inutile che ci giriamo intorno: basti guardare quello che succede con l'eccesso della decretazione d'urgenza, a quanto spesso votiamo la fiducia o a quanti disegni di legge di iniziativa parlamentare diventano legge in questo Paese; noi saremmo in teoria i legislatori, ma ricordatemi un disegno di legge che sia nato da questi scranni. Siamo arrivati ad approvare una legge che istituisce il premio per il miglior pasticcere d'Italia, che era di iniziativa governativa: il Governo cioè si è riunito per licenziare un disegno di legge premio al miglior pasticcere d'Italia, quindi le possibilità di legiferare non esistono. Allora, in un sistema nel quale il legislatore non legifera e l'Esecutivo legifera anche quando non c'è un caso di necessità ed urgenza, il Parlamento funziona farraginosamente, come vediamo anche nelle Commissioni: quante volte in Commissione la maggioranza va sotto, perché c'è una festa di compleanno? Questo accade perché abbiamo un numero di parlamentari incongruo rispetto ai meccanismi istituzionali. La questione allora è che noi dovremmo riformare la Costituzione per dare a un Paese del G7 come l'Italia, un Paese fondatore dell'Unione europea, istituzioni funzionanti, ma purtroppo invece facciamo riforme - e qui dissento dal senatore Gasparri che non consegnano un quadro coerente e unitario che mette il Paese in condizione di funzionare meglio. Torno infatti al collega De Cristofaro, che ha ragione da vendere, quando chiede come mettiamo

in cui non eravamo in grado di sapere chi veniva vaccinato in un posto e chi in un altro; abbiamo un turismo sanitario che non finisce più, perché se uno è nato a Lamezia Terme e uno a Meda, Meda, in provincia di Monza, i livelli sanitari e dell'assistenza sanitaria non sono assolutamente comparabili. Non avrebbe più senso allora fare un disegno unitario, piuttosto che farsi scambi che sono chiaramente quelli di

costituzionalizzato la legge elettorale e non siamo in grado di votare per una legge elettorale che non conosciamo è perché l'accordo non si è ancora realizzato. Allora dire "questo a te, questo a me e quest'altro e qualcun altro" non significa governare il Paese, ma governare un'accolita, un gruppo di persone o un'associazione privata, di gente che si è simpatica; da qui ad assolvere la responsabilità di governare il Paese, però, scusatemi, ma ce ne corre. Signor Presidente, ringrazio anche il senatore Franceschini che ci ha dato la possibilità di intervenire, così almeno lo ricordiamo per l'ennesima volta, perché sembra veramente che sia difficile far capire come stanno le cose: questa maggioranza politica che governa il Paese si regge non solo, ma anche sulla base di un patto politico chiaro. La Lega vuole l'autonomia; Fratelli d'Italia vuole il premierato; Forza Italia spinge di più sulla giustizia. È tutto scritto in un programma elettorale che abbiamo depositato quando ci siamo candidati alle elezioni politiche, che condividiamo tutti e che il centrodestra condivide da tanti anni, perché la riforma del 2005 fatta dall'allora ministro Calderoli Calderoli contemplava il Senato federale, quindi la distribuzione di più poteri ai territori, l'elezione diretta del *Premier* e la riforma della giustizia. Quindi è il progetto politico del centrodestra, che viene sempre avanti negli anni, a seconda dei Governi che ci sono, con coerenza. *(Applausi)*. Guardi, lo dico sinceramente, lo dico a lei e lo dico a tutti. Lei tra l'altro ha

Le alleanze e i campi larghi si costruiscono sulla base dei patti politici; se non ci sono i patti politici, non ci sono le alleanze. E il centrodestra questo patto politico l'ha saputo fare, infatti governa questo Paese.

fatevene una ragione. Questa è una maggioranza politica. Voi siete un campo troppo stretto. Signora Presidente, anch'io ringrazio il collega Franceschini per aver alzato un po' il livello del dibattito, il che ci consente di fare alcune riflessioni al di là del merito del singolo emendamento. La digressione sul tema dello scambio tra le varie proposte politiche delle forze di centrodestra mi appassiona meno, nel senso che è abbastanza evidente che c'è un Governo sostenuto da una maggioranza fatta da diverse forze politiche, che hanno ciascuna legittimamente alcune ambizioni come forza politica e che stanno assieme in un programma. Incidentalmente ricordo che il premierato non è parte di quel programma di Governo, dove, in modo forse più pulito dal punto di vista della della Carta costituzionale, si proponeva l'elezione diretta del Presidente del Repubblica, cioè un presidenzialismo puro, che avrebbe portato un altro tipo di dibattito in quest'Aula. Però volevo entrare nel merito di alcune delle considerazioni fatte dal collega Franceschini sull'origine e sulle motivazioni con cui, legittimamente e in modo ambizioso, questa maggioranza propone questo tipo di riforma: la governabilità, il tentativo di legare il Governo alle forze politiche che hanno vinto le elezioni, scongiurando Governi tecnici e ribaltoni, e una stretta connessione tra il voto dei cittadini e gli eletti, il Presidente del Consiglio in questo caso. Quindi una partecipazione più diretta

Si fa l'esempio di come storicamente in questo Paese si siano succeduti decine e decine di Governi con durate molto limitate. Però, vedete, nella Prima Repubblica, in quella che viene in modo giornalistico definita Prima Repubblica, la governabilità esisteva non tanto per la continuità effettiva di un Governo, ma erano in qualche modo la postura politica e il disegno politico delle forze che erano maggioranza che consentivano consentivano una continuità dei Governi, a prescindere da chi era il Presidente del Consiglio e da chi erano i Ministri. Tanto che all'epoca era molto più importante fare il Capogruppo di una forza politica che stare al Governo o addirittura fare il Presidente del Consiglio, perché la governabilità in qualche modo era legata più allo stare insieme, sulla base di leggi elettorali proporzionali, di alcune forze politiche che avevano sempre la maggioranza e che davano continuità all'azione di Governo, a prescindere dal Governo e dal Presidente del Consiglio. Sul tema della governabilità è la Seconda Repubblica che ha fallito quella missione, sulla base di una spinta maggioritaria che in qualche modo il Paese aveva. ha portato, invece, come diceva giustamente il collega Franceschini, a far stare insieme in modo forzato componenti politiche che poi, una volta al Governo, non riuscivano a governare. La durata di questi Governi ha dato instabilità, non di quelli formati con la legge proporzionale e sulla Costituzione esistente, che davano una stabilità del sistema Paese anche nei confronti dell'estero. Sul tema dei ribaltoni basterebbe molto meno e questa riforma non ci consente di dire che, per forza, non ci saranno mai maggioranze diverse che sostengono un altro Governo. Questo perché, nel momento in cui io posso dare un altro incarico a un secondo Presidente, non è scritto da nessuna parte che quel secondo Presidente, seppur espressione della maggioranza che ha vinto le elezioni per uno spostamento di alcuni parlamentari, potrà ottenere una fiducia da forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni. Il terzo elemento: l'espressione diretta dei cittadini nei confronti degli eletti. Non è certamente la mia forza politica che si schiererà contro un'elezione diretta, ma è l'impianto costituzionale in cui si inserisce che non ci convince. Perché non passiamo, invece, ad un sistema di elezione con le preferenze, dove i cittadini possono decidere, finalmente, chi entra qui dentro? Io credo che quella sia la modalità giusta per dar voce ai cittadini. che stiamo facendo, il combattere per non avere tempi contingentati, il tentativo di alzare il livello della discussione per fare emergere quello che qui dentro succede, non è legato al fatto che riteniamo illegittimo ciò che state facendo. sono molto preoccupato dal mosaico che si compone tra l'autonomia differenziata, il premierato e la riforma della giustizia, ma di questo avremo modo di parlare. Il nostro dibattito qui non è sulla legittimità di ciò che state facendo; è sul fatto che lo riteniamo profondamente sbagliato.

molto bene i termini della questione. Dopo di lui, però, il senatore Romeo ha confermato quello che da questa parte si è sempre detto: che c'è un patto ed è un patto di maggioranza per fare determinate cose. Io non ho niente da dire su questo. Sono figlio di una cultura di Governo, per cui capisco che chi governa

le faccio volentieri e poi starà a questa parte trovare gli equilibri per andare avanti insieme. Tanto insieme non siamo comunque o, perlomeno, non troppo insieme. Io ho piacere che si possa finalmente parlare, ma ho la sensazione che il testo proposto sia assolutamente blindato così com'è. Da questa parte sono arrivate delle proposte, a mio avviso anche sensate. Però, se da parte della maggioranza c'è la volontà di portare avanti quel testo lì, così com'è, qui si parla a vanvera. Questo volevo dire e questo ho detto.

voluto pronunciarla con la Presidenza del senatore La Russa, ma vale lo stesso. Ieri è stata una giornata abbastanza particolare e io ho capito quanto segue - lo dico a me stesso - anche facendo un po' leva sugli Uffici del Senato. Il Presidente del Senato - o la Presidente del Senato - non deride, il Presidente non sbeffeggia, il Presidente non schernisce, il Presidente non usa sarcasmo, il Presidente non chiosa, il Presidente non parteggia, il Presidente non trasforma quest'Aula nel bar sport. *(Applausi)*. Presidente Malan - naturalmente mi rivolgo a lei per il tramite della Presidente - lei ci ha spiegato che il Presidente della Repubblica, se ho capito bene, può svegliarsi male al mattino e sciogliere le Camere. È un'interpretazione curiosa, che peraltro il presidente Balboni ha negato, ma mi attengo su essa e sono anche agghiacciato dal pensiero che il Presidente della Repubblica, se è all'estero, può essere sostituito che a sua volta il Presidente supplente magari può svegliarsi male e sciogliere le Camere solo mandando un messaggino ai Presidenti delle Camere, in questo caso all'unico Presidente che resta, avendo l'accortezza di farsi rispondere. È un'interpretazione però, oltre che curiosa, molto rivelatrice, e io la dico così: il vostro problema sono le prerogative del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non lo avete votato, non vi fidate di lui, non lo apprezzate, non lo rispettate. Farete precipitare questo Paese in una disputa referendaria e trascinerete per i capelli il Presidente della Repubblica nella mischia, suo malgrado e nostro malgrado. Anche e soprattutto per questo perderete. Lo sapete e infatti, a parte la baldanza - come dice il senatore Franceschini - di questi giorni, sarete voi stessi a mettere questo ircocervo istituzionale su un binario morto. Sarà comunque un peccato non aver potuto ascoltare l'opinione di alcuni illustri senatori in questa discussione. Il presidente Zaffini, ad esempio, non si è retto e ieri, con la sua stentorea voce, ci ha detto che l'opposizione non può bollinare gli interventi della maggioranza. Per mio limite non ho capito non ho capito nemmeno a quali interventi della maggioranza si riferisse. Certamente ho capito che lo ha detto dopo che il presidente Balboni aveva "censurato", non bollinato, gli interventi dell'opposizione, denunciando ogni parola cruda, ma detta "parlamentarmente", Presidente. Cito le belle parole di Giacomo Matteotti. Ha censurato tutti, presidente Balboni, tranne che la ministra Casellati, che ha mandato a quel paese un senatore. Ha avuto una censura selettiva, diciamo così. Si è lamentato perché la senatrice Maiorino ha detto che la maggioranza è asservita al Governo. Io le suggerisco la rilettura, con una riflessione terminologica, del vocabolario: vi sono due parole, una con un'accezione negativa (servo) e un'altra che dovrebbe avere un'accezione positiva (servitore). Si dice, ad esempio, positivamente di un servitore dello Stato, che, con la vostra riforma - a proposito di quello che ha detto la senatrice Maiorino - può essere servitore del Governo, e sarà uguale Rivendicando di essere un uomo libero, presidente Balboni, lei ha detto qui che non è asservito a nessuno, nemmeno al Governo, né alla Presidente del Consiglio. Allora io le voglio dire che anche da questa parte del Parlamento siedono uomini e donne liberi. Liberi anche di difendere la memoria e l'esempio di chi, anche rappresentanti di quest'Aula, ha avuto la libertà davvero conculcata, le vite violentate, strappate via, gli aggrediti, i carcerati, i confinati, gli uccisi nel tempo più buio della nostra storia. Da quel sacrificio nasce l'equilibrio della Carta costituzionale, su cui avete giurato, ma verso cui, in fondo, come sul presidente Mattarella, avete una certa antipatia. Grazie solo a questo, presidente Balboni, voi oggi siete uomini liberi anche di insultare la loro memoria. Meno liberi di fare di questa madre di tutte le riforme, una riforma su cui discutere. La Presidente del Consiglio ha detto che non si dimetterà, eppure è la principale delle riforme a cui è legata questa maggioranza. Altro sarebbe stato se fosse stata affidata alla discussione parlamentare. Delle altre voci che non ho ascoltato vorrei citarne alcune: per stima; quella del presidente De Carlo, la cui squillante voce abbiamo sentito sulla carne sintetica, sul premio al maestro della cucina, ma non sulla riforma della Costituzione; quella del senatore Rastrelli, le cui assertive arringhe abbiamo sempre apprezzato, impreziosite da molte citazioni, a volte in latino, a volte in *latinorum*: nemmeno una parola oggi. Ma una menzione speciale, l'ultima, la debbo fare del senatore Menia. I suoi interventi sono spesso pensosi, profondi, sentiti, a tratti lacrimevoli, spesso sulla storia, a volte su una personale protostoria parallela, anche sulla pseudo-storia, ma niente sulla riforma costituzionale. Ha persino rinunciato a parlare quando lo ha interrotto il presidente La Russa: scatti ferini sì, ma nessuna parola. In conclusione, signora Presidente, vorrei dire che sinceramente capisco la frustrazione di chi è asservito a un *Diktat:* stare in silenzio, subire e votare. *(Commenti).* In fondo è solo l'antipasto di come volete ridurre la Repubblica parlamentare: una Repubblica in cui conta la parola di uno solo o ma il vostro non sarà mai il silenzio degli innocenti.

radicata evitare riferimenti al Presidente della Repubblica in carica, rispetto al quale tutti ci sentiamo vincolati al più alto rispetto istituzionale. *(Generali Signora Presidente, torno un po' sul tema precedente, anche perché si rischia di fare confusione. La forma di governo e il rapporto tra centro e periferia non si escludono: si può tranquillamente parlare di forma di governo e di rapporto tra centro e periferia e, quindi, di autonomia. Venendo all'autonomia, che è stata più volte tirata in ballo, vorrei semplicemente rammentare a tutti noi che dovremmo sapere come funziona, che non è una concessione, ma è semplicemente un diritto. Mi spiego: l'articolo 5

la Repubblica riconosce il diritto al lavoro. Cosa deve fare la Repubblica? Deve attuare queste cose nella Costituzione effettiva, nella Costituzione materiale, cioè

Lo stesso vale per l'autonomia: c'è un diritto all'autonomia che è riconosciuto e che è nostro dovere mettere in campo, e c'è un dovere di contribuire al benessere della Nazione. C'è sempre un equilibrio in Costituzione, però - attenzione l'autonomia non è una concessione a una parte politica, ma è un diritto dei cittadini riconosciuto in Costituzione. vorrei anche esprimere un invito a non cadere in una retorica della intangibilità delle parti - consentitemi di chiamarle così - meccaniche della Costituzione. Io sono uno di quelli che sottoscrive il fatto che la nostra Costituzione è un testo meraviglioso che contiene princìpi altissimi, che sono stati d'esempio a tanti altri Costituenti di Repubbliche più giovani della nostra. E noi dobbiamo essere affezionatissimi al cuore al cuore dei valori repubblicani, alla forma repubblicana, alla nostra cultura della pace, della democrazia, al fatto che la Repubblica è fondata sul lavoro, al principio di uguaglianza, al fatto che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza dei cittadini. Tuttavia non confondiamo, non facciamo

Sappiamo, avendo tutti noi letto i lavori preparatori e avendo studiato la storia di questa Carta costituzionale, che le decisioni sono state spesso di compromesso, dettate, dettate, naturalmente, anche dalla necessità di arrivare a un testo condiviso tra culture molto differenti, in uno scenario internazionale neanche lontanamente comparabile con quello di oggi. oggi. Per cui - lo dico ai colleghi dell'opposizione - non entriamo in una sorta di contemplazione di un testo dandogli una sacralità che non ha in tutti i suoi luoghi. C'è una parte frontale, visiva, e c'è una parte di *back office*, che deve essere funzionante proprio per consentirci di consegnare al Paese quei valori che sono proclamati nella I Parte della Costituzione. il principio per cui dobbiamo fare un lavoro migliorativo, che dobbiamo mettere mano alle tante cose che non vanno, prendendo atto semplicemente che la realtà continua a stiracchiare il testo costituzionale, perché poi la realtà non si fa ingabbiare e quindi nei decenni la nostra Repubblica ha preso anche strade che non assomigliano a quello che leggiamo. Vi sfido a leggere il procedimento legislativo come descritto in Costituzione e a chiederci, colleghi e colleghe, se assomiglia neanche lontanamente a quello che facciamo tutti i giorni: davvero leggiamo i testi due volte, poi c'è la navetta che torna indietro? Sappiamo come legiferiamo: ormai questa Camera ratifica, il 50 per cento delle volte, provvedimenti discussi altrove; dobbiamo chiamare i colleghi della Camera per chiedere, per favore, di presentarci gli emendamenti che qui non abbiamo il tempo o la possibilità di presentare.

di adottare una retorica per cui tutto va bene e non si tocca niente, perché semplicemente non è così.

spiegare questioni anche piuttosto elementari, ma è evidente che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Vorrei allora, tramite lei, signor Presidente, provare a spiegare al collega della Lega che mi ha preceduto che l'autonomia di cui si è parlato è ben diversa da come è stata dipinta in quest'Aula. Naturalmente, lo faccio più a vantaggio di chi eventualmente dovesse ascoltare questo mio intervento che a vantaggio della maggioranza che ovviamente, tra incapacità e non volontà di comprendere, continuerà a non capire. Lo faccio utilizzando non le mie parole, ma le parole di uno dei tanti costituzionalisti che non solo sono venuti in Commissione, ma continuano - ahimè - a far scorrere fiumi d'inchiostro sulle pagine dei giornali, ma evidentemente tutto invano. Uno di loro scrive: in secondo luogo per l'autonomia differenziata. Non è il principio in sé a farci storcere la bocca: se una Regione rivendica ulteriori competenze che corrispondono alla specifica vocazione del proprio territorio, ai suoi tratti peculiari, nulla di male ad ad accendere il verde del semaforo. In via eccezionale, e con una richiesta motivata», cosa che non è prevista, invece, nel disegno di legge Calderoli. «Però se tutte e quindi le Regioni ordinarie possono ottenere tutte tutte e ventitré le materie in ballo, allora l'eccezione si converte in regola, e la nuova regola è lo sfascio, l'anarchia. Con buona pace dell'unità degli italiani evocata dall'articolo 5 della Costituzione», che in maniera mistificatoria è stata tirata in ballo proprio in quest'Aula. Queste sono le parole di Ainis, uno dei tanti costituzionalisti che hanno cercato di spiegarvi anche il perché il premierato non va bene. Allora sfatiamo, sempre attraverso le parole di Ainis, perché il vostro premierato non va bene: «Qualcuno può affermare che l'elezione diretta del Capo del Governo costituisca una bestemmia? No». Quindi sfatiamo anche questa menzogna. Non è la questione dell'elezione diretta di per sé che è irricevibile: «No di certo, dal momento che funziona nelle due democrazie più antiche, negli Stati Uniti e in Francia. Ma se in Italia il *Premier* eletto ha un potere di vita o di morte sulle Camere, se prosciuga le funzioni di garanzia attribuite al Presidente della Repubblica, se torreggia tal quale un gigante in un paese di nanetti, allora sì, c'è di che allarmarsi». Ecco perché vi stiamo ripetendo in tutti i modi di fermarvi e di bloccare lo sfascio della nostra Costituzione.

ed è articolato sulle Regioni. Oggi è stata introdotta invece l'autonomia differenziata: questo è il dato. Il problema è che ciò presuppone il fatto che i cittadini nel nostro Paese non abbiano i servizi e le

sostanziale. Come qualche esperto ci ha spiegato, c'è una specie di secessione dei ricchi, così come abbiamo cercato di spiegare che c'è il voto di censo, perché sempre più

Questo è nel piccolo quello che succederà nel grande livello. Non potete venire a spiegarci che l'uno compensa l'altro, ossia che il premierato compensa la questione dell'autonomia differenziata, perché o c'è l'uno

pubblica e universale. Perché oggi è pubblica, ma non è universale? Proprio perché è stata spezzettata in venti Regioni. spezzettata in venti Regioni. O prendiamo atto di questi fatti e cerchiamo di intervenire per modificare, oppure imbrogliamo i cittadini e le cittadine, perché non saremo in grado di dare un sistema

qualche minuto fa il presidente Boccia lamentava il fatto che un esponente della maggioranza fosse intervenuto un po' fuori tema, non attenendosi all'emendamento che era in votazione. Mi chiedo come siamo riusciti ad arrivare a parlare dell'autonomia differenziata in relazione a un emendamento che parla dello scioglimento delle Camere. Anche questo è un mistero che il senatore Boccia immagino censurerà, come ha censurato prima l'intervento del collega della maggioranza. Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per rassicurare, tramite lei, il collega Fina Fina che anch'io sono intervenuto parlamentarmente. Non è che intervenite solo voi parlamentarmente, colleghi: visto che siamo in Parlamento, anche il senatore Balboni interviene parlamentarmente. Penso che siamo tutti sullo stesso piano.

considera concetti positivi, mi dispiace, ma non li considero così e non sono d'accordo con lei. Al collega che poco fa ha detto che il Presidente del Consiglio con la nostra riforma avrà il potere di nominare e revocare i Ministri,

compete al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Il potere è però del Presidente della Repubblica ed è un potere in più rispetto alla Costituzione vigente, perché - come sapete - su chi è titolare chi è titolare del potere di revocare i Ministri c'è stata una lunga discussione in dottrina e non si è mai giunti a un'interpretazione unanime. Alla senatrice Rossomando, che si e ci interroga su cosa intendiamo per «eletti», rispondo che intendiamo che gli elettori vanno a votare e scelgono da chi essere rappresentati: semplicemente questo. Certo, oggi

cento di noi: questa è la ragione per cui Fratelli d'Italia, ma il centrodestra in particolare, quando si arriverà a discutere della nuova legge elettorale, proporrà un sistema nel quale il potere di scegliere gli eletti venga riconsegnato agli elettori e non a tre, quattro, cinque o sei *leader* di partito. Ci sono due strade, i collegi uninominali oppure le preferenze: si valuterà e si discuterà, come ha garantito il ministro Casellati; su questo ci sarà un confronto, anche e soprattutto con le forze di opposizione. Ultima questione: vede, signor quando abbiamo discusso dei senatori a vita, l'opposizione ha trascinato nella polemica senatori a vita che non sono assolutamente in discussione, perché - come sappiamo anche se la riforma sarà approvata, i senatori nominati resteranno giustamente in carica con tutte le loro prerogative e continueranno ad essere senatori di serie A come quelli eletti, e anche di più. Però, senatore Boccia, non è che non condividere un intervento, tra l'altro garbatissimo, di un senatore a vita - mi riferisco alla senatrice Cattaneo, che ha tutto il mio rispetto e credo di averglielo sempre dimostrato in ogni sede non è che, se io non condivido un suo giudizio o una sua interpretazione, le manco di rispetto. Anzi, credo sia esattamente il contrario, perché mi metto sullo stesso piano di un senatore che può avere legittimamente idee diverse dalle mie. Credo che questa si chiami dialettica democratica, non si chiama mancanza di rispetto. Certo, capisco che, se

Chiamare in causa il Presidente della Repubblica, nei confronti del quale abbiamo tutti il massimo assoluto rispetto, in una riforma che tutti sanno che, quando entrerà in vigore, il mandato dell'attuale Presidente della Repubblica sarà ampiamente scaduto, è un'operazione scarsamente elegante,

ha votato diversi Presidenti della Repubblica. Da Ciampi in poi li ho votati tutti; anzi, Ciampi l'ho votato, gli altri no, per la verità. Ma, nel momento in cui sono stati eletti, sono stati considerati da me e da tutto lo schieramento che rappresento i Presidenti della Repubblica di tutti gli italiani, di chi li ha votati e di chi non li ha votati. Questo è l'ABC della democrazia. *(Applausi)*. Guardi che lei parla con una persona che, anche se dispiace al collega Fina, è un uomo libero. Non perché voi non siate liberi; ma io non mi sono mai permesso di dire ai colleghi dell'opposizione che sono asserviti, mai mi sono permesso di dire questo. Per me, certo che i colleghi dell'opposizione sono uomini liberi. Dario Franceschini mi conosce da mezzo secolo e credo di avere sempre rispettato i miei avversari. Il problema, Presidente, è che i miei avversari non rispettano me: è questo il problema. *(Applausi)*. Per cui sono costretto a spiegare che, come sono uomini liberi loro, si dà il caso che siamo uomini liberi anche noi. Tutto qua. qua. Alla luce di tutto questo, credo che faremmo tutti un servizio alla democrazia e alla dignità dei nostri lavori parlamentari se rimanessimo un po' di più al tema e se divagassimo un po' di meno. *(Applausi)*.

e se è ancora valida quella norma, che abbiamo più volte chiesto di rivedere, secondo la quale sono compresi nei tempi anche gli interventi sull'ordine dei lavori. Stiamo comunicando a ciascun Gruppo il tempo rimanente. Come è stato detto in Conferenza dei Capigruppo, è conteggiato anche il tempo

Presidente, intervengo perché il 3.1177 è un emendamento soppressivo. È una presa di posizione impegnativa ed è - come accennavo anche in fase di illustrazione - il tentativo di mettere in collegamento

lo scioglimento è praticamente sempre atto dovuto. Quello che veramente spiazza, nella lettura del testo che stiamo qui a votare,

La filosofia di questo disegno di legge è proprio di evitare che salti la coerenza tra il voto popolare e l'assetto di Governo del Paese. Questo è il frutto, naturalmente, di un sistema puramente proporzionale, quale era stato immaginato al momento della scrittura della Costituzione; è una sorta di delega in bianco al Parlamento. Noi, in questo momento, funzioniamo così. Il popolo elegge il Parlamento, il Parlamento rappresenta il popolo; a quel punto, il Parlamento ha le mani libere e questo significa che l'unico legame di consequenzialità tra il voto e l'assetto istituzionale del Paese sta nel fatto che, se io ho votato Mario Bianchi o Giovanna Rossi, quella persona è diventata parlamentare e, da quel momento in poi, Mario Bianchi e Giovanna Rossi hanno soltanto una responsabilità politica. Tale responsabilità si traduce nel fatto che, tra cinque anni, dovranno rendermi conto del loro operato e io, elettore, deciderò se meritano ancora la mia fiducia o se non la meritano più. Questo è il sistema come funziona oggi. Naturalmente, questo significa che, per esempio, nel 2018, quando il 4 marzo abbiamo votato, l'esito elettorale ha chiarito chi erano i parlamentari, ma non ha dato segno della possibilità di formare

il corpo elettorale non ha avuto più alcun controllo di quello che succedeva. Abbiamo avuto un Governo gialloverde, formato da una polarità e un pezzo di una seconda polarità; poi abbiamo avuto un Governo giallorosso, formato dalla medesima polarità iniziale, il MoVimento 5 Stelle, e dall'altra polarità, quella di sinistra; poi si è terminata la legislatura con un ulteriore Governo, secondo me il migliore dei tre, che era un Governo di unità nazionale. perché la delega dell'elettorato dava carta bianca ai parlamentari di cambiare idea, anche in modo ampio: tant'è che noi, giustamente,

si deve tornare alle urne e il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere. Succede, invece, come poi vedremo nell'articolo 7, che non è sempre così. Questo introduce un elemento di incoerenza

Non si sta risolvendo il problema democratico che sta nella usurpazione sostanzialmente totale del potere legislativo da parte dell'Esecutivo. a stabilizzare e a costituzionalizzare questo problema, come avete dimostrato nella misura in cui non avete voluto modificare l'articolo 77 della Costituzione. Voglio provare però a introdurre un'altra tematica, che sembra stia sfuggendo alla maggioranza. maggioranza. Voi state concentrando tutti i poteri all'interno del Palazzo del Governo, dove si prenderanno le decisioni. Avete pensato mai alle ricadute sulla rappresentanza territoriale? La presidente del Consiglio Meloni è venuta nel mio territorio, ha fatto una corsa con i bersaglieri, ma non si è accorta dei problemi che aveva intorno quel territorio. Ha fatto una bellissima corsa, ma non si è accorta che ci sono tantissimi tantissimi cantieri fermi, che il sindaco sta cercando di risolvere problemi che questo Governo ha creato, non si è accorta che non si riesce ad andare avanti con la ricostruzione delle aree sismiche. sismiche. Questi problemi li può vedere un parlamentare che vive nei territori, non li può vedere un Presidente del Consiglio. Non è manco colpa sua. Può venire a fare una sfilata, ma non conosce i territori. Parlamento: il parlamentare sta vicino ai territori, può essere interpellato dalla gente. Il Presidente del Consiglio può farsi vedere dalla gente, si può fotografare, ma non conosce quei problemi.

aveva bloccato la ricostruzione delle aree sismiche. Un vostro parlamentare ha dovuto dire al suo Governo che stava sbagliando e stava mettendosi in difficoltà. Se non ci fosse stato un vostro parlamentare, non un vostro Ministro, ancora qui avremmo avuto problemi a mandare avanti

monocorde, un monologo interno al Palazzo? Il Governo non può conoscere i problemi delle infrastrutture. Ecco perché si fanno le stupidaggini. Come fate a spiegare ad alcuni territori che hanno carenze infrastrutturali che sarebbero risolte con pochi milioni di euro e poi magari concentrate tutte le risorse - 13 miliardi, se non sbaglio - sul Ponte dello Stretto; poi bocciate gli emendamenti sulla perequazione infrastrutturale dei territori. dei territori. Questi errori li commettete perché non state sui territori. Venite soltanto a fare propaganda elettorale, ma non conoscete i territori. E poi vi siete dimenticati delle aree di crisi industriale complessa? Le aree di crisi industriale complessa sono problemi che divergono da una Regione all'altra e questi problemi li conoscono il Parlamento e i parlamentari. Il Governo che cosa può fare? Può fare interventi che ancora non risolvono i problemi di quelle aree che sono tipizzanti di ogni area territoriale; possono riguardare le infrastrutture e solo problemi di natura geografica che il Governo non conosce. Ancora, i disegni di legge dei parlamentari che fine hanno fatto? Siamo invasi da decreti legge, o tutt'al più disegni di legge di origine governativa. Il Parlamento è già scomparso. Voi lo state cancellando definitivamente. a parlare il senatore De Cristofaro efficacemente - secondo me - ha detto che il Parlamento è scomparso. E lo faccio anche sulla base di una serie di dati che adesso le leggo, che il presidente Boccia ha giustamente enunciato nella riunione dei Capigruppo che abbiamo fatto oggi pomeriggio, ma che reputo giusto diffondere anche qua per capire di cosa stiamo parlando. Io ho fatto quella domanda a lei - e naturalmente ringrazio gli Uffici per la solertissima risposta - sui minuti che mancano a ogni Gruppo per sapere perlappunto quando poi i tempi saranno esauriti: da una parte perché volevo sapere effettivamente quanto tempo ci rimane dall'altra parte, anche per evidenziare la cosa che sta accadendo in quest'Aula negli ultimi giorni e settimane. Noi stiamo discutendo della riforma costituzionale con trenta ore di dibattito, con tempi contingentati; fra un'ora di interventi, naturalmente, a me sarà tolta la voce; fra una cinquantina di minuti di interventi sarà tolta la voce al Presidente e ai senatori del Partito Democratico; fra un'oretta e qualcosa sarà tolta la voce ai senatori del MoVimento 5 Stelle e questo accade per l'appunto non su un normale provvedimento, ma su una riforma costituzionale. Colleghi, soltanto per soltanto per avere un metro di paragone e per sapere di cosa stiamo discutendo, quando in quest'Aula il Senato affrontò, nella XVII legislatura,

Se in questo caso noi abbiamo avuto soltanto quattro sedute di discussione generale prima del voto degli emendamenti e due sedute in cui discutere il totale degli emendamenti, ai tempi ai tempi della riforma Renzi avemmo otto sedute di discussione sul complesso del progetto di riforma, quindi esattamente il doppio, e ben 15 sedute aggiuntive per l'esame e il voto degli emendamenti. *(Applausi)*. Peraltro, sappiamo anche che in quel caso il senatore Calderoli presentò un numero di emendamenti leggermente superiore - diciamo così a quelli che sono stati presentati dalle opposizioni. Ricordo anche alle senatrici e ai senatori che il contingentamento del canguro, con il quale ci stiamo raccapezzando da qualche settimana a questa parte, all'epoca

si sono capite le ragioni del dissenso e lo ha capito il Paese); io non lo giustificavo neanche in quel caso -capiamoci - perché considero il canguro, le tagliole e strumenti esattamente funzionali a quello che è successo negli ultimi decenni, e cioè allo spostamento del potere decisionale sempre di più dal Parlamento al Governo. Non è che questa cosa è nata per caso. Non è che i Regolamenti parlamentari sono stati modificati per caso, perché c'è il destino cinico e baro. Ciò fa parte esattamente della cosa che stiamo cercando di dire, cioè che da molto tempo a questa parte, da molti decenni a questa parte, questa modalità e questo andazzo stanno determinando una progressiva riduzione di potere del Parlamento, che arriva in questo caso al paradosso incredibile che discutiamo la riforma costituzionale in prima lettura in quattro sedute e con il canguro deciso al primo secondo di gioco (così si direbbe, se parlassimo di sport). Però capite bene che, siccome non parliamo di sport, di sport, ma di Costituzione, questo ci lascia molto, molto perplessi. Figuriamoci cosa succederà se sciaguratamente dovesse passare il premierato, ma non succederà perché gli italiani, che sono molto saggi, lo bocceranno sonoramente nelle urne.

è evidente che siamo in un contesto molto particolare, in cui si vuole giocare con le parole, modificandole senza un'adeguata riflessione.

su questa proposta di modifica della norma elettorale. Quello che ci manca è molto semplice, è il concetto generale: dove vogliamo arrivare. Non vogliamo arrivare soltanto alla modifica della Costituzione, ma alla modifica della Costituzione abbinata alle leggi che seguiranno, perché il concetto complessivo è dato dalla modifica costituzionale e dalle leggi che seguiranno. Se non sappiamo come saranno le leggi, anche la modifica costituzionale è un po' fine a sé stessa. Sarebbe molto meglio, invece, ragionare insieme, poi è chiaro che la maggioranza valuterà e deciderà con i numeri che le sono propri, ma sarebbe bene ragionare insieme anche di dove vogliamo arrivare. Io, per esempio, anche perché dalle mie parti funziona così, sono un acceso sostenitore dei collegi uninominali, dove l'eletto risponde alla propria gente dell'elezione e torna dalla propria gente a confrontarsi sul da farsi, cosa che non avviene con l'attuale sistema elettorale. Sono dell'avviso che anche da noi si dovrebbe introdurre finalmente una modifica tale per cui chi cambia bandiera va a casa, perché

tra le diverse forze di maggioranza, cioè tra coloro che vogliono la modifica della Costituzione, coloro che vogliono l'autonomia differenziata e coloro che vogliono una riforma della giustizia. Così finiamo per avere tre prodotti malfatti. più benfatti possibile, perché chiaramente è mio interesse di cittadino che le norme approvate da questo Parlamento siano le migliori possibili, ma ho forti dubbi che questo accada e se non accade è proprio perché c'è questa ostinazione

Signora Presidente, intervengo in dissenso, ma il mio dissenso non è tanto rispetto all'emendamento di specie, non me ne voglia il collega De Cristofaro. Il mio è un dissenso più generale rispetto al clima, rispetto al clima, al contesto e al testo. Io credo che in questa discussione non stiamo dando una bella immagine del nostro Parlamento e temo che i cittadini italiani lo puniranno con un altissimo astensionismo e ognuno di noi si dovrà prendere le proprie responsabilità, se il partito più grande in Italia continuerà a essere il partito dell'astensione.

La mia preoccupazione è che il messaggio che stiamo facendo passare ai cittadini italiani è che il Parlamento si possa sciogliere per inutilità. Continuo, nei miei interventi, a ribadire quanto invece sia importante, come hanno sottolineato le opposizioni, salvaguardare le prerogative delle funzioni parlamentari e la dignità del Parlamento, riconoscere che nella nostra Repubblica parlamentare, se il Governo è ospite di quest'Aula, è perché in qualche modo sono i parlamentari che gli devono riconoscere la fiducia e devono esercitare l'iniziativa legislativa, della quale sono stati espropriati. Qui il tema dello scioglimento delle Camere non dipende dal *quorum*, ma dal senso che diamo alla funzione che ricopriamo.

perché dobbiamo pensare che un *Premier*, un Presidente del Consiglio possa essere più legittimato dal voto diretto degli italiani e non riconosciamo la stessa democrazia e la stessa legittimazione ai parlamentari che sono stati eletti. Lei fa riferimento a una legge elettorale che verrà dopo, ma come si può pensare di mettere insieme, nel momento in cui andiamo a votare, con i tempi contingentati che ci vengono dati, una riforma costituzionale sulla base di una riforma elettorale che oggi non esiste? È questo il dissenso, signor Presidente, non solo rispetto all'emendamento, ma rispetto al fatto che pensare che una maggioranza possa modificare da sola la Costituzione, il che è un errore grave e imperdonabile per tutti.

Signora Presidente, facciamo una prova. Supponiamo che la riforma costituzionale così come l'avete immaginata vada a buon fine a buon fine e che anche la legge elettorale che ci avete detto approverete con premio di maggioranza che inserirete in Costituzione vada a buon fine, con l'accordo, ovviamente, della sola maggioranza, perché noi non siamo d'accordo. Proiettiamoci quindi alle nuove elezioni, in cui ci sarà un Parlamento formato presumibilmente dal 55 per cento di parlamentari che sono stati eletti con la nuova legge elettorale e con una nuova Costituzione vigente. Il nuovo articolo 88 della Costituzione reciterà: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere», quindi quello che state sostenendo adesso è che il Presidente mantiene il potere di scioglimento delle Camere. Il secondo comma prevede che non possa esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto e quindi vi riferite alla modifica entrata in vigore allora, tramite l'articolo 7.

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». Questo viene modificato ulteriormente. «Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio Voi avete modificato anche questa parte, che sarà quindi vigente in maniera diversa. Potrà succedere che nella prossima legislatura il Presidente della Repubblica si alzerà al mattino,

compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Succederà

il Presidente della Repubblica andrà a sciogliere le Camere perché è impazzito, voi lo metterete in stato di accusa e avrete la maggioranza per farlo. Allora di che cosa stiamo parlando? State mentendo agli elettori, perché non esiste che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere liberamente, come avete sostenuto fino ad non esiste e non è scritto da nessuna parte. Vi invito a fermarvi. Fermatevi, perché state facendo una cosa obbrobriosa.

sconcertante, è una mancanza di rispetto verso il popolo italiano, verso le istituzioni e verso la Costituzione davvero inenarrabile, una cosa senza precedenti. Prima sono state elencate le ore di discussione che hanno comportato tentativi di modifica costituzionale e questa è la dimostrazione plastica della degenerazione che stiamo vivendo e del fatto che siamo già davvero a un livello bassissimo di rispetto delle Istituzioni e del nostro stesso ruolo. Lo sottolineo perché quello che state facendo, anche se continuate a negarlo, è togliere completamente ai parlamentari qualunque potere di rappresentanza e di autonomia. L'unica scelta che sarà lasciata ai parlamentari, infatti, sarà se seguire comunque il *Premier* eletto in qualunque circostanza, qualunque cosa accada, oppure determinare la propria morte politico-istituzionale, perché le Camere dovranno essere sciolte. Questa non è governabilità: è una rigidità

ad altri cittadini e cittadine di entrare in queste Aule o di legiferare. Faccio allora nuovamente presente, come ho già fatto in altre circostanze, che avete ben cinque Ministri nella vostra squadra di Governo che non sono mai stati eletti da nessuno, eppure legiferano attraverso i decreti-legge. *(Applausi)*. Mentite quindi agli italiani, quando dite che soltanto il voto popolare può far governare questo Paese, che oggi è già

non è possibile che siano concessi pochi minuti alle forze di opposizione per gridare il proprio disappunto contro questa mostruosità che state cercando di mettere a terra.

una riforma costituzionale così importante meritasse una discussione più ampia, con l'utilizzo del contingentamento e dei cosiddetti canguri in una fase successiva. Francamente io, come molti di voi sanno, sono un reduce della campagna del 2016, nel senso che all'epoca ero il Sottosegretario per le riforme costituzionali; quelle quelle sedute di cui parlava il collega De Cristofaro credo di averle fatte tutte qui, in quest'Aula del Senato, nonostante fossi deputato all'epoca e mi sembrava una cosa normale, quando si mette mano a un pezzo della Costituzione così importante. Certo, nel 2016 erano molti di più gli articoli; ma le variazioni e le modifiche che stiamo deliberando in questo modo vanno a incidere in modo ugualmente importante, forse addirittura più importante, di quanto non succedesse nel 2016. Ebbene, credo che sarebbe stato il caso di dare

un mio disagio. Non credo che, quando si parla di una riforma costituzionale, si possa farla breve. Fa parte un po' del gioco; io mi rendo conto, essendo stato in maggioranza, che c'è una pressione a raggiungere l'obiettivo quanto prima possibile. Però se questo è concepibile su disegni di legge ordinari, quando si mette mano proprio al funzionamento e alle regole del gioco, che devono devono unire tutte le parti, non lo è. Si può dissentire nel merito delle questioni, ma si deve riconoscere tutti insieme come è fatto il campo di gioco, quali sono le regole del gioco, chi è l'arbitro. Quando si tratta di mettersi d'accordo su questo, credo che non ci sia limite di tempo che tenga. Così come penso che sarebbe importantissimo porsi in un atteggiamento di ascolto più ampio. Devo dire che in parte l'atteggiamento di ascolto annunciato dalla ministra Casellati si è visto, ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo non lo abbiamo visto. Tant'è che appunto ci sembra che questo disegno di legge, alla fine, non ci consegni delle istituzioni meglio funzionanti e una meccanica del processo legislativo e della gestione del potere esecutivo più equilibrata, più efficace, più capace anche di dare risposte brevi brevi e rapide davanti a un tempo che corre e che ci chiede di essere capaci di elaborare soluzioni molto più rapidamente, nel mondo globalizzato nel quale viviamo. Io intervengo in particolare per annunciare il mio voto favorevole a un emendamento successivo questo, che sarebbe però dichiarato decaduto se l'emendamento in votazione venisse approvato: quello che dice che, per poter sciogliere il Parlamento, il Presidente del Consiglio deve verificare che non ci sia un'altra possibilità di formare un Governo. Ora, in linea di principio io penso che questo, se vogliamo essere coerenti, non dovrebbe essere permesso mai. Il Presidente della Repubblica, in un sistema come quello disegnato dalla ministra Casellati, nello scioglimento. Se il Governo viene a mancare, essendo il Governo stato eletto con il Parlamento, dovrebbero andare via insieme. Ma dato che, come sappiamo, in questo disegno di legge è previsto un Presidente del Consiglio di scorta, allora io credo che, quando

Signora Presidente, ho dimenticato di dirlo prima: ieri c'era stato un paventato boicottaggio nei confronti del Gruppo delle Autonomie, perché si era rotto il microfono. Ringrazio gli addetti del Senato, che l'hanno riaggiustato in tempi rapidissimi; c'è un'efficienza straordinaria, che va sottolineata. Riprendo quello che ha detto il collega Scalfarotto, perché effettivamente questo emendamento che andiamo a discutere e, probabilmente, a vederci bocciato è migliorativo del testo proposto. Io vorrei rifarmi ad una una citazione di Massimo d'Azeglio, un politico italiano vissuto tra il 1798 e il 1866, che è stato senatore quando senatori a vita erano Manzoni e Carducci, giusto per citare due esempi particolari di senatori a vita di alto profilo. Sì, va bene, era il Senato del Regno, ma sempre senatori a vita erano. Massimo d'Azeglio diceva che l'assoluto è il peggior nemico della buona politica, come l'assenza dell'aspettare è la sua più fedele alleata. porsi in maniera assoluta a difendere un testo blindato è evidentemente in contrasto con questa massima di Massimo d'Azeglio, che io ovviamente condivido in pieno. Quanto all'aspettare, adesso si aspetterà, io confido che questa attesa al *post* elezioni europee consenta qualche ripensamento rispetto al testo di questo provvedimento. Avremo alcuni giorni e sicuramente ci sarà modo di riflettere, anche da parte della maggioranza, e valutare se ci sono degli aggiustamenti da apportare. che è necessaria, potrà, se la maggioranza vorrà, essere usata per migliorare questo testo. Questa attesa è stata provocata dall'opposizione, grazie ai suoi numerosissimi emendamenti, che hanno portato a fare l'accordo per cui

intervenire su questo testo. Sono convinto, infatti, che questo testo sia migliorabile anche nell'ottica della maggioranza. Non è migliorabile solo nell'ottica dell'opposizione, che peraltro ha anche visioni abbastanza diverse al suo interno. La maggioranza è riuscita a compattarsi, ma non è perché si è compattata che allora bisogna rimanere fermi. Cerchiamo Cerchiamo di fare il bene del Paese, cerchiamo di fare il bene del popolo italiano e, se si devono aggiustare alcune cose che meritano di essere aggiustate, io confido che questa maggioranza abbia le capacità di farlo.

della riforma e noi, su questo tema, vogliamo essere molto chiari. Quando ci siamo presentati al confronto con il Governo abbiamo detto chiaramente per noi questa era una riforma irricevibile, perché toccava il cuore dell'equilibrio dei poteri, andando a indebolire il Presidente della Repubblica. Voi vi rincorrete in affermazioni in cui provate a giustificare il fatto che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati. colpite al cuore quello che è il garante, l'arbitro della Costituzione, in un momento in cui i cambiamenti profondi nella società, come la transizione ecologica e digitale, polarizzano le società e c'è bisogno di di garanti, di arbitri, ma anche di persone che tengano insieme il Paese e ne garantiscano la coesione sociale. Lo dimostrano gli Stati Uniti, dove lo scontro fortissimo fra Biden e Trump ha dimostrato tutta la necessità di avere una figura in cui si riconoscano la maggioranza dei cittadini. Voi, invece, indebolite questa figura. Quello che ci preoccupa di più, però, e lo voglio dire chiaramente in quest'Aula è la mancanza di un terreno comune, della capacità di definire delle regole condivise, non solo sulla Costituzione, ma anche nella gestione, nella conduzione di una riforma così importante. Si può fare tutto: si può discutere, si può litigare, ma non ci si può dividere sulle regole. *(Applausi)*. Nella discussione che facciamo, abbiamo bisogno di riconoscerci in un terreno comune.

che voi ci avete concesso - uso questa parola - l'allora riforma Renzi, la riforma della Costituzione, ebbe ben otto sedute di discussione e 15 sedute aggiuntive. Il contingentamento e il canguro ci furono, come avete ricordato voi, ma furono applicati solo dopo ben dieci sedute. *(Applausi)*. Voi invece avete fatto subito ricorso a questo strumento.

Chi mi conosce, lo sa, vengo dalla carriera diplomatica, sono persona mite, in politica, anche nei momenti più duri, provo prima a sorridere.

davanti a una maggioranza sorda, davanti all'incapacità di trovare un terreno comune, io penso che un messaggio, un segnale, un simbolo nei confronti di una regola che abbiamo sempre rispettato tutti qua dentro. E quindi con il gesto, che certo non ha a che fare con la violenza verbale o fisica,

Colleghi, vi invito a riprendere posto. Metto ai voti

Signor Presidente, in queste lunghe, frustranti giornate in cui siamo inchiodati in quest'Aula a fare questo esercizio di resistenza, alla fine ho fatto una riflessione, in particolare quando arriviamo a valutare gli emendamenti sulla composizione del Parlamento e sul legame tra Presidente del Consiglio e Parlamento. Fondamentalmente, si vuole istituzionalizzare una situazione che già di fatto è così, nel senso che, sulla base di un contratto sinallagmatico tra le forze di maggioranza, cui io do una cosa a te e tu in cambio dai una cosa a me, tutti siamo legati a doppio filo al Presidente del Consiglio per garantire la tenuta di questo Governo. Con questa riforma, si vuole vincolare istituzionalmente la maggioranza del Parlamento al Presidente del Consiglio, che può decidere se, come e quando sciogliere le Camere e mandare tutti a casa. A questo punto vi chiedo: collegato con il premio di maggioranza, quindi, il Presidente del Consiglio avrà i propri parlamentari, che potranno - come ora - vincere tutte le votazioni; a questo punto, a cosa serve il Parlamento? Qual è il ruolo dei parlamentari? Non serve assolutamente a nulla, quindi suggerisco alla maggioranza di riflettere se in questa riforma non sia addirittura il caso di eliminarlo, il Parlamento, perché i parlamentari non serviranno a nulla. *(Applausi)*. Il Presidente del Consiglio si crea i propri uffici tecnici e governa per cinque anni da solo, perché non ha bisogno di sentire nessuno e non ha bisogno dell'appoggio di nessuno, quindi è assolutamente un uomo o una donna solo al comando e il Parlamento, con questa riforma, diventa totalmente totalmente inutile, come lo è oggi. Signor Presidente, penso che la senatrice Sironi abbia perfettamente ragione, nel senso che c'è da porsi perlomeno il problema su cosa bisognerà fare di questo Parlamento. Ribadisco quello che ho detto prima, cioè che adesso ci sono alcuni giorni su cui riflettere. Qui richiamerei un episodio storico interessante soprattutto in questo edificio, che ricordo questo edificio, che ricordo essere stato per decenni proprietà del Vaticano, che vi aveva stabilito la sede della polizia vaticana, da cui Madama, come viene chiamata oggi la polizia municipale: ricordo che nel 1294 il papa Celestino V fece il gran rifiuto, abdicò e venne sostituito da Bonifacio VIII. Ebbene, si dice che Bonifacio VIII, il cardinal Caetani, prima che Celestino V si dimettesse, avesse trovato un marchingegno per cui, attraverso dei sistemi a tubo, faceva pervenire a Celestino V, mentre dormiva nel suo letto, delle voci che sembrava venissero dall'aldilà e pare che fosse lo stesso Caetani a dire: «Celestino, dimettiti, Celestino!». E lui, convinto che fosse Dio, alla fine si dimise

alla vocazione turistica di Roma, che è quello che la tiene ancora in vita. Bonifacio VIII ha quindi avuto la sua ragione storica per diventare Papa. Ma perché dico questo? Perché adesso ci sono alcuni giorni e hai visto mai che nelle orecchie del presidente Balboni o della ministra Casellati che dormono non arrivi una voce dall'alto che dica «Pentitevi, fate qualcosa di meglio!»: questa è l'unica cosa in cui possiamo sperare perché questo testo venga migliorato.

Invito i senatori Segretari a controllare.

Il Senato è in numero legale.

In quel caso c'è stato un celeberrimo scambio tra il capitano dei Carabinieri e il *boss* della zona, che ha definito, secondo una scala, gli uomini in cinque classi: uomini, mezzi uomini e via dicendo, e comunque l'ultimo era - non so se è pertinente per quest'Aula - un quaquaraquà dal punto di vista politico.

Mi riferisco all'inserimento, in base all'articolo 81, di un disegno di legge sulla riforma, il testo unico sulle isole minori. Qua dentro c'è il presidente Romeo, che ha preso un impegno pubblico, suffragato dal Ministro di riferimento, per la procedura accelerata d'urgenza, in quanto il disegno di legge era stato approvato nella scorsa legislatura. In quest'Aula il Presidente di turno ha avallato la richiesta del presidente Romeo, che ha sovvertito l'inserimento nella Conferenza dei Capigruppo; 8 marzo 2023, in quest'Aula. Pertanto, Presidente, nella qualità

Pertanto vi chiedo in virtù di questo. E poi il ministro Calderoli, ai primi di gennaio di quest'anno, è stato chiamato a rispondere in Aula. Anche in questo caso Calderoli ha detto: «Da qui a pochi giorni avrete già pronto il disegno di legge di iniziativa governativa». Voi continuate a far calpestare il ruolo dei parlamentari e dei senatori in maniera, dal nostro punto di vista, indegno.

Gli isolani, le isole minori italiane, non sono un orpello. È stata una presa in giro. E ci sono tanto di prove: dall'8 marzo 2023 ad oggi soltanto chiacchiere. Due Ministri della Repubblica che prendono in giro gli italiani.

a giudicare con il voto alle elezioni europee e avranno elementi in più per valutare chi votare e chi no. Chiedo, quindi, ai Capigruppo delle altre opposizioni di esprimersi: se per loro è per loro è più urgente trattare un disegno di legge in via prioritaria e d'urgenza o continuare a trattare questo obbrobrio normativo, che offende l'Italia e la Costituzione.

sull'ordine dei lavori perché ho una curiosità. I due posti aggiuntivi sono posti che servono al Governo o sono posti per i senatori? Se sono posti del Governo,

io continuo a insistere su questo dato. Ovviamente, noi siamo di fronte al fatto che, in sostanza, stiamo costruendo un sistema in cui il potere è tutto in mano a una persona.

cercando populisticamente di descrivere l'elezione diretta del *Premier*. Anche i senatori e i deputati dovrebbero essere eletti dal popolo; però con quale legge elettorale. Se, ad esempio, si tratta di una legge elettorale proporzionale, o di una legge elettorale proporzionale con preferenze; no, questo non si sa e non è dato sapere.

I Padri costituenti - vorrei ricordarlo a tutti - hanno fatto una Costituzione in cui prevedevano che questo Parlamento rappresentasse

la Costituzione italiana, che è nata dalla Resistenza e dalla lotta partigiana antifascista - sottolineo antifascista - è stata fatta e nello stesso tempo si sono preoccupati di fare in modo che tutte le opinioni fossero rappresentate, cosa che voi state negando.

Siamo seri tra di noi: in tutti i Paesi, visto che è stata più volte sottoposto la questione (a me non fa né caldo né freddo se uno mi dice che Putin ha nominato i senatori a vita perché non è mai stato mio amico;

Per noi delle minoranze linguistiche questo è il punto più dolente della riforma. Nel loro ruolo di garanti della Carta costituzionale, i Presidenti della Repubblica si sono più volte dimostrati importanti difensori delle minoranze linguistiche. Penso agli anni nei quali le autonomie speciali sono state messe sotto attacco o a quei Governi che non mostravano troppa simpatia per la minoranza di lingua tedesca. In tutte queste circostanze la Presidenza della Repubblica ha giocato un ruolo importante nel richiamare gli Esecutivi ai loro doveri costituzionali e al rispetto degli accordi internazionali che sono alla base della nostra autonomia. Un Presidente con poteri limitati e che, con ogni probabilità, sarà individuato tra le figure di stretta vicinanza del Presidente del Consiglio, perché non avrà bisogno del voto delle opposizioni per essere eletto, cessa di essere una figura terza. Diventa a tutti gli effetti una figura ombra del Presidente del Consiglio e quindi una figura che risponde a una logica politica di parte. Smetterà di essere una figura *super partes* di tutela dei princìpi costituzionali: un pericolo e una minaccia, perché un Paese non lo si governa solo con la forza della decisione, ma anche con quei contrappesi, con le figure terze, con le autorità di garanzia, che sono l'essenza stessa della democrazia.

Signor Presidente, stiamo provando fin dall'inizio a spiegare che il nostro approccio su questo disegno di legge vuole essere il più possibile laico e il meno possibile In conseguenza di questo, avevamo anche stabilito una modalità sulla base della quale il nostro voto sui vari articoli si sarebbe voluto attenere il più possibile al merito delle questioni, rimandando la valutazione di carattere politico più generale al termine del nostro lavoro. Ciò non è stato reso possibile sull'articolo 1 per le note vicende di cui abbiamo abbondantemente discusso ieri e sulle quali non torno, anche perché prendo atto positivamente della decisione del Presidente del Senato di investire l'Ufficio di Presidenza di tutto ciò. Tutto questo invece rimanda all'esigenza di dover affrontare il voto dell'articolo 3, in considerazione del fatto che abbiamo votato a favore dell'articolo 2, essendo stato un recepimento di una nostra proposta in sede di Commissione, in un quadro più sistemico, perché inevitabilmente, nel momento in cui si affronta il potere del Presidente della Repubblica, questo non può che tenere conto di un quadro d'insieme. Quest'ultimo rischia di confermare l'elemento di confusione a cui abbiamo cercato di fare riferimento nel corso di queste discussioni. Rimando a tal proposito, ancora una volta, all'intervento del senatore Renzi di ieri, perché la maggioranza, nel tentativo di venire incontro o di rispondere inconsciamente, surrettiziamente, inconsapevolmente alle preoccupazioni della opposizione circa la natura e il potere del Presidente della Repubblica, ha pensato di rispondere, tra l'altro con un pregevole lavoro del senatore Pera di cui voglio dare atto, con un articolo successivo, in cui gli atti e le controfirme del Presidente della Repubblica vanno nella direzione di un potenziamento. Quindi, qui ci troviamo in una sorta di sbilanciamento. Con un articolo, i poteri del Presidente della Repubblica vengono ridotti, con l'altro, su un altro versante, i poteri del Presidente della Repubblica vengono aumentati e la bilancia comunque la si veda è fuori asse. È inevitabile che questo sia considerato considerato dal punto di vista oggettivo, ma mi richiamo ancora una volta all'autorevole - e sotto questo aspetto condivisibile - intervento del senatore Pera in discussione generale. Il senatore è venuto a dirci che non tutto può essere rimandato alla legge elettorale; noi abbiamo presentato un ordine del giorno in cui ponevamo questo tema come un elemento discriminante la maggioranza ha ritenuto di bocciare questo nostro ordine del giorno. Il senatore Pera ha messo in fila una serie di questioni che sono oggettivamente piombo all'interno della prosecuzione di questa riforma: di questa riforma: la questione del voto degli italiani all'estero; il tema della possibile discrasia tra il voto alla Camera e il voto del Senato, mantenendo l'impianto diverso tra Camera e Senato sul premio di maggioranza (nazionale alla Camera alla Camera e regionale al Senato), circostanza che ha già ampiamente creato problemi in passato, e modalità con la quale il premio di maggioranza si va a configurare. Queste cose sono tutte impregiudicate, sono ancora tutte aperte, sono ancora tutte da sciogliere, però si è partiti dal Presidente della Repubblica; cioè, anziché affrontare e risolvere queste problematiche che darebbero un elemento di organicità, si parte parte da una diminuzione dei poteri della più alta magistratura del nostro Paese. Questo non significa che non si possano mettere in discussione il ruolo, la natura e la funzione del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica in Germania ha una funzione e un equilibrio e in Francia ne ha tutt'altro, così come in Austria, dove ha addirittura un ruolo di garanzia e viene eletto direttamente dai cittadini. In quei contesti, però, c'è un elemento di organicità che consente di affrontare anche consente di affrontare anche una possibile riforma dell'istituto della Presidenza della Repubblica. In questo caso, invece, si parte da questo punto di vista, colpendo la Presidenza Repubblica e lasciando aperto tutto il resto. È una cambiale in bianco che non ci sentiamo di dovervi dare.

disegnando un Parlamento eletto a maggioranza, a strascico di una sola persona: il Capo del Governo eletto; considerate, peraltro, che non per caso si chiama Capo del Governo, che è un potere, mentre il Parlamento dovrebbe esercitarne un altro, quindi c'è già una commistione, davvero quantomeno segno della vostra imperizia costituzionale. Il Parlamento viene eletto a maggioranza, a strascico di una sola persona, il Capo del Governo;

Qual è la funzione di questo Parlamento? A cosa serve un Parlamento siffatto? Qual è l'indipendenza e l'autonomia di pensiero di chi, certamente eletto dal popolo, ma sicuramente non con non con le preferenze (perché vorrò vedere se davvero metterete nella legge elettorale le preferenze), entra in queste Aule? In che modo è autonomo, indipendente e rappresenta il popolo? È evidente, rispondo io alla collega Sironi: non serve a

il potere di scioglimento delle Camere, il potere di nomina del Presidente del Consiglio e, davvero per *surplus* di spregio, avete tolto anche la possibilità di nominare i senatori a vita. Cosa rimane a fare il Presidente della Repubblica? Cosa arbitra? Andrà ad arbitrare le partite di calcio la domenica, perché qui non servirà più a niente. Davvero avete la faccia di di bronzo di mentire palesemente alle persone, perché la verità è che avete in spregio la democrazia e la partecipazione popolare. A voi piace soltanto la folla acclamante, magari possibilmente guardandola da un balcone, come ai vecchi tempi.

è così si che si innerva e si vivifica alla democrazia. Avete bocciato tutti gli emendamenti che rafforzavano lo strumento del *referendum* e delle leggi di iniziativa popolare. Questo significa volere la partecipazione delle persone, avere rispetto del popolo, che a voi manca completamente. Siccome ho deciso in corso d'opera che farò una mia battaglia per difendere e tutelare il buon nome dei costituzionalisti che rischiano di essere infangati, li menzionerò uno per uno.

non è affatto, come il Governo afferma, limitata dal momento che viene a colpire il cuore del nostro governo parlamentare - sembra porsi come obiettivo primario, forse più che l'efficienza del Governo (che già oggi dispone di poteri adeguati e di una forza talvolta eccessiva), il conseguimento di una vittoria culturale di portata storica diretta a cancellare l'originaria ispirazione fondativa del nostro impianto repubblicano. Ispirazione che, nel clima politico e culturale europeo e mondiale che si respirava nel secondo dopoguerra in antitesi con i regimi autoritari che avevano condotto alla guerra, si riassumeva nella visione di una democrazia a potere diffuso che collocava al centro della Costituzione non lo Stato e i suoi poteri, ma la persona e le sue libertà e che, di conseguenza, per garantire il pluralismo politico ed il garantismo istituzionale, collocava il Parlamento in posizione centrale. Rispetto a questo quadro introdurre, come oggi si vuol fare, l'elezione popolare diretta della persona investita della guida del potere esecutivo non significa quindi tanto riformare quanto ribaltare uno dei criteri ispiratori di base del nostro modello costituzionale, un modello che ha inteso in primo luogo evitare il primato dell'Esecutivo fondato sulla concentrazione del potere nelle mani di un solo organo o di una sola persona (...). Se questo Se questo disegno di legge che il Governo persegue con tanta tenacia condurrà alla fine» - qui c'è una profezia e credo che vi convenga ascoltarla, perché non la faccio io, ma la fa qualcuno che di democrazia e di Costituzione ne capisce ne capisce - «come oggi si pensa, alla prova referendaria, la divisione di fondo che verrà ad emergere nel nostro Paese non sarà, dunque, quella tra chi vuole e chi non vuole le riforme vogliamo riforme costituzionali in grado di migliorare la funzionalità del nostro governo parlamentare), bensì tra chi vuole una riforma orientata a ribaltare l'ispirazione originaria della Costituzione vigente e chi vuole, invece, con la riforma, conservare le basi del modello democratico su cui la nostra Repubblica è stata fondata». A questo andate incontro.

reticente dibattito e confronto abbiamo capito perché tanta difficoltà da parte dei senatori di maggioranza nell'entrare nel merito e nel risolvere quelle che sono oggettive contraddizioni o, peggio, insostenibili torsioni del nostro modello democratico. Abbiamo spiegato perché la riforma determina una concentrazione del potere in una sola carica che non ha eguali e non ha precedenti storici. abbiamo anche insistito molto per far sì che ciascun senatore prendesse la parola, spiegasse, dicesse che in effetti sarebbe bene apportare questa correzione o quest'altra, e invece niente: sempre e soltanto il silenzio. La spiegazione, purtroppo - lo abbiamo detto - ha trovato conferma ogni giorno: è uno scambio consumato in una sede extraparlamentare che ha fatto sì che i paladini dell'autonomia differenziata non potessero intervenire, pur essendo palesemente critici, per correggere le distorsioni più gravi, che non potessero far valere quei principi di ragionevolezza che pure a volte nei corridoi abbiamo sentito condividere. Lo stesso copione lo abbiamo visto durante la discussione sull'autonomia differenziata: il principale partito di Governo non perdeva occasione di di testimoniare il proprio imbarazzo e cercare in qualche misura di raccontare che quella riforma era stata corretta, era stata rivista, era stata mitigata, insomma che non c'era nessun rischio di vera autonomia.

C'è un qualche filo che lega queste tre riforme? C'è un qualche aspetto che le tiene insieme? C'è un qualche profilo politico e culturale che ne spiega la ragione e spiega perché alla fine questo compromesso questo compromesso non solo al ribasso, ma in danno del Paese, si è potuto realizzare? In realtà c'è, e lo abbiamo ascoltato anche nelle ultime ore. Il tratto comune a queste tre ipotesi di riforma è innanzitutto una insofferenza, un'ostilità, una avversione al pluralismo, che significa avversione alla separazione del potere. *(Applausi)*. Tutte e tre le riforme sono tre modalità per concentrare il potere. Anche l'autonomia differenziata, onorevoli colleghi, è in realtà una forma di concentrazione del potere. Nella potere. Nella riforma del premierato tutto si concentrerà nell'elezione del Presidente del Consiglio e il Parlamento sarà ad esso sottoposto. Con la riforma dell'autonomia differenziata, per come l'avete scritta, non sarà il Parlamento a determinare i livelli essenziali delle prestazioni; non sarà il Parlamento a stipulare con le Regioni le intese che poi dovranno essere formalizzate nella legge, farà un DPCM, cioè il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione; tutta la attuazione dell'autonomia differenziata avverrà tra esecutivi. Il Presidente del Consiglio

in tutto e per tutto dalla volontà del Presidente del Consiglio. Saranno i DPCM a decidere cosa trasferire, che cosa è il livello essenziale delle prestazioni, come si adeguano i livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché il Parlamento per voi è un problema... la prego di concludere. non soltanto il potere chiamato ad applicare la legge, ma anche il potere chiamato a porre un limite all'arbitrio e agli abusi del potere che la politica è naturalmente portata a compiere. L'intera impalcatura costituzionale si regge su questo su questo grandissimo principio fondante: la separazione e la limitazione del potere, il che significa primazia del Parlamento, del pluralismo e dei diritti, e la netta separazione delle funzioni. Voi, con queste tre riforme, state concentrando il potere in una sola figura e state cercando di sottoporre al potere politico anche il potere giudiziario. Questa è la vera ossessione che anima tutta la vostra azione.

a spiegare ai suoi elettori quello che sta succedendo, perché poi questo *Premier* non sappiamo neppure se e quali materie sarà disposto a cedere, però su questo se la vedranno i colleghi della Lega. Adesso però, signor Presidente, non posso nascondere una profonda preoccupazione. Nei tanti interventi del ministro Casellati non ho sentito spendere parole sul problema che ho più volte sollevato: qui non si è parlato mai dello Stato di diritto.

Un altro dovere di verità è poi quello di spiegare ai cittadini e anche a noi parlamentari che ve lo stiamo chiedendo, colleghi, come pensate che questa riforma possa essere compatibile con i valori condivisi non soltanto a livello europeo. Come pensate che questa riforma possa considerarsi compatibile con i valori indicati nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea? È inaccettabile, questo silenzio. State girando intorno a un problema che è unico ed è di democrazia. allora che il Governo spendesse qualche parola su questo, ma soprattutto che ci dicesse se, una volta che non c'è più l'equilibrio tra i vari poteri, l'Italia la possiamo ancora considerare una Repubblica democratica. Possiamo considerarla democratica, se ci sarà un *Premier* che può mandare a casa il Parlamento e non potrà essere sfiduciato, se il Parlamento non torna a casa e non si torna al voto? Dateci queste risposte, Ministro: una sola risposta ci potrebbe essere sufficiente per aprire una riflessione, però su questi temi non si può rimanere in silenzio.

e il successivo 4.1002 non hanno alcuna portata modificativa e, quindi, confermano il testo dell'articolo 4 proposto dalla maggioranza. Quindi, ringrazio i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che, pur formulandolo in modo diverso, confermano esattamente che non è soggetta a controfirma tutta una serie di atti del Presidente della Repubblica. Semplicemente loro dicono che la controfirma è atto dovuto,

in relazione alla nomina dei giudici della Corte costituzionale. Quindi, a proposito di atto dovuto, in questi emendamenti si parla proprio di atto dovuto. Che si dica che l'atto non è soggetto a controfirma o che si dica che la controfirma è atto dovuto - mi rivolgo a lei, Presidente - credo che sia esattamente la stessa cosa. Quindi ringrazio il MoVimento 5 Stelle per aver espresso, seppur con una formulazione diversa, esattamente gli stessi contenuti proposti dalla maggioranza.

io noto che questo è l'articolo 4, giusto? Noi abbiamo già votato a favore dell'articolo 2 e credo che voteremo a favore anche dell'articolo 4. Lo dico con soddisfazione, perché questo è un articolo pieno di buonsenso, che mi sembra dica delle cose chiarificatrici che approfondiscono in modo pensato il ruolo del Presidente della Repubblica. Si dice che il Presidente della Repubblica - come sappiamo - è irresponsabile, per cui c'è sempre bisogno della controfirma. Però ci sono degli atti - diciamoci la verità - che promanano direttamente dalla volontà del Presidente della Repubblica, che sarà pure irresponsabile in teoria, però

positivo nei confronti del lavoro della maggioranza per esprimere un enorme rammarico. Su alcune questioni si è ragionato. che questo è il secondo articolo su quattro, quindi sul 50 per cento degli articoli che abbiamo trattato finora c'è stata un'apertura. Perché questa apertura si è voluto che fosse soltanto cosmetica? Perché il metodo del buonsenso, il metodo del contenuto, il metodo dell'ordine, dell'approfondimento, del chiarimento, dell'esplicitazione di prassi già consolidate che passano in Costituzione non lo si è applicato anche ad altre questioni, che sono veramente sostanziali? Noi abbiamo

di connazionali all'estero che votano con un voto che non è proprio uguale a quello degli altri, ma fa eccezione all'articolo 48 della Costituzione,

dubbio. Sull'uguaglianza invece dubbi non ce ne sono. Gli italiani all'estero, per eleggere un parlamentare, devono essere tanti di più di quanti devono essere gli italiani per eleggere un parlamentare in Italia. Allora, questi cinque milioni di elettori all'estero saranno computati ad "uno vale uno" - come dicevano un tempo i colleghi del MoVimento 5 Stelle - oppure saranno considerati persone che hanno soltanto un diritto di tribuna, come oggi? oggi? Forse, noi dovremmo ragionare non più di voti, ma di seggi? Stabilire che è eletto direttamente Presidente del Consiglio chi ottiene più seggi? Allora, però, dovremmo capire qual è la legge elettorale che trasforma i voti in seggi, ma noi questo non lo sappiamo. lo sappiamo. Quando ci siamo messi al tavolo, abbiamo individuato questioni come questa della controfirma del Presidente della Repubblica, che però è piccola cosa. Diciamo la verità: si tratta di decidere quando non ci sarà bisogno della controfirma, ma noi sappiamo che spesso la controfirma è atto dovuto. Quindi, è un elemento più estetico che sostanziale. Se, infatti, il Presidente della Repubblica decide alcune cose, in in alcuni casi chi deve controfirmare è tenuto a controfirmare. Nel confermare, ancora una volta, che noi come Gruppo eravamo aperti e desiderosi di un confronto; nel confermare che, quando questo confronto c'è stato e ha prodotto dei risultati, noi li apprezziamo, tant'è che votiamo a favore dell'articolo 4, pensiamo di dover lasciare agli atti di questo Senato che il fatto che la maggioranza abbia limitato la sua apertura solo a questioni estetiche e cosmetiche è veramente una grande occasione persa per il nostro Paese.

Scienze forestali, sono un alberologo e qui ritengo di essere l'unico, mentre ci sono tantissimi avvocati. Nella mia esperienza di amministratore pubblico, io ho potuto constatare in più occasioni che, quando gli avvocati mettono mano agli atti, normalmente li allungano. Quando io divenni sindaco della mia città, ritrovai 146 regolamenti elaborati da coloro che mi avevano preceduto, o meglio dai loro giuristi, che complicavano enormemente la vita agli uffici e mi premurai di farne sintesi, riducendoli a una ventina. Qui io vorrei sottolineare che l'articolo 89 della Costituzione, che andiamo a modificare con questa proposta, è lungo sei righe, di cui tre nel primo capoverso e tre nel secondo. Invece, la proposta fatta nel documento è di undici righe. Io so per esperienza che, quando si allungano i testi di legge, si dà spazio agli avvocati per poter intentare cause. In questo Senato oggi ci sono quarantatré avvocati. Sono di gran lunga la categoria più rappresentata e nulla mi toglie dalla testa che qui ci sia anche una certa componente mentale di vantaggio personale, o perlomeno di vantaggio per la categoria: complichiamo un po' le norme, che così lavoriamo tutti un po' meglio. Non credo che sia una cosa che corrisponda ai bisogni del nostro Paese. Io sono convinto che dovremmo semplificare le norme e qui non lo stiamo facendo. Vorrei solo sottolinearlo e magari richiamare la maggioranza a un ripensamento.

stiamo discutendo, sostanzialmente, è una domanda. Che Aula è quella il cui destino viene messo nelle mani del potere esecutivo? Che dignità c'è per una senatrice o un senatore nel sapere che, a seconda di quelli che saranno la sua scelta saranno la sua scelta e il suo voto, potrà essere cacciato via dal *leader* e con il *leader*? Siete troppo bravi, troppo preparati, troppo attenti per non aver capito questo interrogativo di fondo; per non aver capito che non ci potrà mai essere in quest'Aula un confronto libero e sereno, una critica autentica, un contrasto, uno scontro in questo dibattito se noi, comunque, saremo sempre accompagnati dal pensiero che potremo restare qua solo finché lui o lei lo vorrà. Colleghi, questo è il punto e questa è la domanda che noi vi poniamo. Noi staremo in quest'Aula solo fino a quando il *leader*, il *Premier* lo vorrà. Quando si stancherà di voi, il *Premier* vi caccerà via. Di questo dovete essere consapevoli! Un'Aula può essere contrappeso al potere esecutivo se è indipendente rispetto ad esso. Il potere esecutivo propone e l'Aula deve avere la forza e la dignità di poter dire no, questo io non te lo voto. Questo è essere senatori e senatrici. La forza di poter dire al *Premier* no, questo provvedimento noi non te lo votiamo e non la paura, il timore, quella condizione di subalternità che ci si infila nel cervello. Attenzione a non spingere troppo, senatore. Attenzione, a non spingere troppo, senatrice, perché, se spingi troppo, ti caccerò e ti rimanderò a casa. Questo è il Senato che volete!

quando salgono al Governo perseguono un obiettivo solo. E quell'obiettivo è il Parlamento. Non è un caso

e uccidere il pluralismo all'interno delle Aule parlamentari! *(Applausi)*. Questo è il primo obiettivo di un dittatore. obiettivo di un dittatore. Dobbiamo imparare dalla storia. Dobbiamo fare attenzione perché qui siamo tutte persone perbene. Ma tra cinque o dieci anni, quando ci saranno i vostri figli, quando ci saranno i vostri nipoti, noi non sappiamo. Ci sarà la *leader*, può essere la vostra Giorgia *(Applausi)*, ma può essere anche una persona che calpesterà i vostri diritti di senatori e di senatrici. *(Applausi)*. Noi dobbiamo fare attenzione, signori, e ve lo diciamo con il cuore in mano. Questa vostra riforma sta alterando gli equilibri tra potere esecutivo e potere legislativo, perché li lega entrambi al medesimo destino. E noi non possiamo avere lo stesso destino che ha il potere esecutivo, perché noi siamo popolo! Noi siamo popolo! *(Applausi)*. Siamo i rappresentanti del popolo e per quanto lei possa... ad essere i veri e autentici rappresentanti del popolo!

Signor Presidente, debbo dire che l'intervento del collega senatore Licheri, con la consueta *verve* la passione che gli sono proprie - e credo che, indipendentemente dal merito delle questioni, vada sempre apprezzato e riconosciuto un collega che crede in quello che dice e ha passione nelle posizioni che esprime all'interno di quest'Aula rimanda ad una questione non banale. Noi diamo una lettura un po' diversa crediamo che bisogna sempre essere molto attenti a gridare "al lupo al lupo" rispetto al rischio dell'affermazione di una deriva totalitaria; non foss'altro per il fatto che, a furia di gridare "al lupo al lupo", alla fine le difese cadono e, quando le cose si realizzano davvero, non scattano più le necessarie barriere immunitarie. Indipendentemente da queste che possono anche essere sfumature a mio giudizio - il tema di fondo che ha posto il collega Licheri deve essere smontato da un'iniziativa della maggioranza. Questo è il punto politico: il senatore Licheri e altri pongono un tema sulla natura della libertà dell'esercizio del parlamentare, ora per allora. Questo, per la verità, è già stato sufficientemente conculcato dalla deriva personalistica e totalizzante interna a tutti tutti i partiti, nessuno escluso. Diceva De Gasperi, nel 1948, commentando l'articolo 49 della Costituzione, che, se vogliono vedere il livello di democrazia di una Nazione, dobbiamo andare a vedere il livello di democrazia dei partiti che rappresentano quella Nazione in un Parlamento e la modalità con la quale selezionano le persone che concorrono poi alle elezioni politiche o amministrative. Guardate, colleghi, questo punto è stato irrisolto per cinquant'anni in questo Paese per motivi storici che qui non riprendo, perché li conosciamo tutti, sia di destra che di sinistra. Dopodiché è stato irrisolto dall'arrivo sulla scena dei partiti azienda e dei partiti personalistici. Guardate che, se noi non sciogliamo questo nodo - e voi avete la responsabilità di doverlo sciogliere, proprio per rispondere a questo tipo di sollecitazioni e, più in generale, per costruire un impianto che regga noi rischiamo di trasferire sul piano dell'ingegneria costituzionale problemi che sono attinenti alla definizione dei processi politici. Aldo Moro insegnava che è sempre un errore trasferire sul piano della geometria istituzionale problemi che la politica non riesce a risolvere autonomamente, perché questo è uno dei problemi per i quali le riforme istituzionali ed elettorali nel nostro Paese hanno portato ad una sterilità. I processi politici non hanno saputo governare, affrontare e risolvere, nel caso specifico, il problema della democraticità della selezione della classe dirigente, oltre che il livello di accesso alla partecipazione e al concorso della vita democratica dei singoli cittadini. Se, infatti, il cittadino X, appartenente ad una determinata Regione o abitante in un determinato Comune, decide di concorrere alla vita democratica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, iscrivendosi ad un partito, cosa fa se trova le porte delle sezioni chiuse o si trova i *blog*, rispetto ai quali si può entrare soltanto accedendo in un certo modo, o se si trova a dover votare soltanto una lista bloccata, prendere o

voi oggi avete questo onere e questa responsabilità. Se lo lasciate cadere, non potrete poi lamentarvi se vi diranno le cose che avete ascoltato pochi minuti fa.

ho sostenuto e sostengo che è necessario riflettere e ripristinare, ad esempio, il finanziamento pubblico ai partiti, che spesso ormai vivono delle rimesse dei

più volte da ciò che pensa Tino Magni, c'è un problema di fiducia, scatta un meccanismo per cui a quel punto lo si mette da parte. È una cosa semplicissima, più semplice di quanto si possa spiegare. Succede così.

basta che uno parli bene, e se razzola male non fa niente. Basta che parli bene, che sia in grado di essere - come si dice - trascinatore con le parole e poco con i fatti. Insisto che questo problema vuol dire affrontare

c'è proprio un rifiuto a discutere nel merito, con un'ottica che, pur con un'alternatività, vada in questa direzione.

credo che non esista precedente - magari mi sbaglio - di una riforma costituzionale in cui un articolo passa senza che nessun Gruppo dichiari niente. Mi pare una sottovalutazione e anche una mancanza di rispetto nei confronti del testo. Visto che votiamo, credo sia il caso di assumerci la responsabilità e di spiegare, lasciandolo per iscritto, perché votiamo in un certo modo. Ho già avuto modo di dire in parte quale sarà il nostro orientamento e di spiegarlo, e lo ribadisco in questa sede. È una proposta che abbiamo accolto anche favorevolmente quando è stata presentata in Commissione. Ci sembra una giusta proposta che vada in una direzione assolutamente condivisibile. Ci sembra anche che quella irresponsabilità del Presidente della Repubblica di cui si parla nella Costituzione fosse un poco limitativa e anche molto formale e non davvero sostanziale. Sappiamo bene che il Presidente del Repubblica assume delle decisioni, sono decisioni importanti, pesanti, alle quali il Paese guarda con estrema attenzione e gratitudine, perché i nostri Presidenti della Repubblica hanno dato sempre grande prova di essere persone del calibro necessario a ricoprire un incarico così alto. E, quindi, ci è sembrato molto giusto che il presidente Pera proponesse questo emendamento in Commissione e che il Governo lo facesse proprio. Lo abbiamo votato allora e lo votiamo anche adesso.

posizioni non necessariamente allineate alla propria maggioranza. E credo che il senatore Pera ci abbia dato un esempio preclaro di questo atteggiamento e penso che di questo dobbiamo ringraziarlo tutti. Però peccato che tutta questa volontà di collaborare, tutta questa partecipazione e questo ascolto non si siano poi realizzati su questioni molto più importanti. Ho già fatto riferimento prima ad alcune problematiche che ci sono, ma abbiamo ad esempio

Parlamento e Governo vengono eletti insieme, quella tradizionale dialettica che vediamo tra il Congresso americano e il Presidente degli Stati Uniti, o tra il Parlamento francese e il Presidente della Repubblica francese, in questo caso non ci sarà. Evidentemente la mancanza di questo rapporto dialettico tra legislativo ed esecutivo va blindata con delle norme che garantiscano che quegli organi, come la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, che devono mantenere il bilanciamento delle garanzie, siano eletti e nominati nel modo più giusto. ha trasformato la democrazia ungherese in una democratura utilizzando le regole che c'erano. Nel momento in cui lui ha potuto nominare la Corte costituzionale, se ne viene fuori molto difficilmente: se approvi una legge incostituzionale, ma la Corte costituzionale l'hai nominata tu, è difficile che te la dichiari incostituzionale. *(Applausi)*. Il tema è che dobbiamo chiedere al Governo di utilizzare, se non in questa sede almeno nella prossima lettura, quello che mi consentirete di chiamare il metodo Pera, per andare a mettere le mani nei punti deboli di questa riforma per il bene del Paese. Alla fine, quando si fanno le regole, si fanno soprattutto

abbiamo il Senato e i senatori che stanno portando avanti un lavoro molto partecipato, un grande confronto; il tentativo con le proposte emendative di raddrizzare, di correggere o di frenare questa riforma; dall'altra parte, abbiamo una *Premier* che dice: voi voi lavorate e poi, se la riforma va o meno avanti, chi se ne importa, pazienza. Qui, signor Presidente, emerge tutta la presa in giro che si nasconde dietro questo provvedimento, ossia distogliere l'attenzione dai problemi veri del Paese e catalizzarla su una riforma che, se poi va avanti o meno, al vostro capo, a donna Giorgia, poco alla fine importa. Quindi ci chiediamo: ma di che cosa vi state preoccupando e occupando? Signor Presidente, qui si racconta la storiella che si deve dare importanza alla volontà del popolo sovrano, e questo provvedimento è la risposta ai bisogni e alle preoccupazioni del popolo sovrano? Ma perché non vi occupate delle cose serie? Mi chiedo se i dati che leggete e i giornali che leggete Parlate di povertà che diminuisce e di *export* che aumenta. Ma dove? Quando? Sarebbe stato bello vedere la stessa passione per argomenti come ridurre le liste d'attesa o sarebbe stato bello parlare seriamente di lavoro. *(Applausi)*. Il lavoro che voi dite che sta aumentando è semplicemente il lavoro povero, il lavoro precario. 3 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Come si fa chiamare questa riforma madre di tutte le riforme? Questa riforma, insieme a quell'altro capolavoro dell'autonomia differenziata, segnerà la morte di tutte le riforme. Altro che madre! Presidente, tramite lei e la Ministra, chiedo veramente di osservare questa riforma da un'altra prospettiva, perché è necessario approfondire tutte le sue conseguenze. Con essa praticamente nessuno, neanche il Parlamento, potrà dare il suo contributo su temi controversi come il fine vita, come l'autodeterminazione delle donne. Con una politica orientata alla "capocrazia", questo succederà, signor Presidente: per voi esiste solo un modo di vivere, il vostro, che ci riporterà al Medioevo e ai racconti dell'ancella. Signor Presidente, il nostro voto è contrario.

È chiaro che il Presidente della Repubblica è stato un riferimento fondamentale e lo è per le Autonomie e abbiamo paura che la sua possibilità di intervento nella vita del Paese venga modificata. Mentre si parlava qui, mi è venuto in mente l'affresco di Cesare Maccari che si trova nell'omonima sala Maccari, in questo Palazzo, che raffigura Cicerone, che

tutti si schierano: perché i senatori sono tutti schierati dietro Cicerone e Catilina è da solo dall'altra parte? Nel Senato romano, che non era a emiciclo, non si votava, ma ci si spostava dietro l'oratore che si riteneva corrispondente al proprio pensiero. Tutti si misero quindi dietro Cicerone, perché così funzionava allora. E qual è oggi la figura di riferimento del panorama politico italiano che può coagulare il consenso di tutti i cittadini? Ovviamente, il Presidente della Repubblica, se agisce in maniera corretta, ma finora abbiamo avuto Presidenti della Repubblica che sono riusciti in questo intento. Ribadisco allora ancora una volta la richiesta di pensarci, pensarci e pensarci: non è che questo

Signor Presidente, volevo ricordare con il mio intervento il Magnifico rettore, professor Anelli, una figura importante nel mondo dell'università, che ci ha lasciato la settimana scorsa. È stato il mio professore di diritto privato alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza. Il 16 maggio era qui con noi nella Sala capitolare per la *graduation day* e il *welcome day* dei due master di innovazione della pubblica amministrazione dell'Università Cattolica. una persona profonda e di straordinaria cultura, che ho avuto occasione di conoscere ed apprezzare durante i suoi tre mandati e durante i miei diciott'anni di docenza a contratto e di collaborazione con l'università. I suoi interventi erano sempre rivolti ai giovani, favorendo il dialogo con loro e spronandoli a intraprendere sempre un percorso di vita non influenzato da stereotipi o da influenze esterne, ma guidato da onestà, trasparenza, schiettezza, senso pratico e soprattutto concretezza. L'università, diceva il professor Anelli, deve pensarsi sempre più come un luogo di costruzione del senso profondo delle cose, come una comunità che progetta la vita, una vita autentica. Signor Presidente, esprimo il pensiero mio e quello del Gruppo Lega, ma interpreto anche quello di tanti colleghi di quest'Assemblea che vogliono unirsi a me per esprimere cordoglio e vicinanza alla mamma, ai suoi cari, ma anche a tutta la comunità dell'Università Cattolica in tutte le sue sedi, al Policlinico Gemelli e all'IRCCS. Per suo tramite, signor Presidente, concludo, rivolgendomi al magnifico rettore, professor Anelli, per dirgli grazie. Riposi in pace.

Anch'io, da studentessa della Cattolica, non ho avuto il professor Anelli come mio docente, ma la sua fama di grande giurista era già presente all'epoca e devo dire che tutti lo ricordano come il rettore che ha guidato l'Università Cattolica in un momento molto difficile, per tre mandati per tre mandati indubbiamente non facili, che si sono confrontati con un mondo che è cambiato incredibilmente. Il magnifico rettore aveva proprio il desiderio che l'università parlasse e rispondesse ai tempi e ricordava sempre che l'università non era una *start-up*, ma non era neppure solo pura e semplice conoscenza; era luogo di confronto, di ricerca e di crescita, lo spazio di democrazia per eccellenza, un laboratorio dove poter far pratica, appunto, di libertà e di democrazia. È chiaro che la sua tragica scomparsa ha lasciato tutti attoniti. La collega Murelli ha rappresentato bene l'emozione e la commozione che tocca chi lo ha conosciuto, che tocca

della libertà dell'università, dell'indipendenza del sapere e di quella capacità di costruire tasselli di democrazia nella quotidianità.

Presidente, sono costretto a contestare la Presidenza in questo caso, perché, vede, quando ad un senatore viene detto che è bugiardo, menzognero, vile, viene fatta un'aggressione e chiede di parlare e avrebbe potuto fare come ha fatto il Capogruppo dei DS

Dicevo che, quando ti accusano di queste cose e tu fai finta di non capire, tu segui il Regolamento (articolo 87, comma 2). Ebbene, parlerò a fine seduta. Ti mettono dopo le commemorazioni e dici: no, io non penso di avere dignità minore di chi prima, abusando della fiducia della Presidenza, che non ritiene di togliergli la parola, parla di cose già passate e, come dire, accusa di una serie di fatti un senatore che ha tutto il diritto di rispondere e di replicare. Vede, *in cauda venenum*. Per davvero, in questo caso.

Avrei potuto rispondere subito, quindi, durante la seduta, avrei potuto utilizzare falsamente un intervento su un emendamento, avrei potuto fare un intervento sull'ordine dei lavori.

*sic et simpliciter*, perché *ipse dixit*, *senator* Boccia, accettare e tacere. Sui fatti di stamane, la Presidenza aveva già detto quello che c'era da dire. Era stata sospesa la seduta e la di aver incaricato i senatori Questori di rendere una relazione sui fatti accaduti in Aula per una valutazione del Consiglio di Presidenza. Ebbene, devo dire che su tutto questo abbiamo i video, abbiamo tutto quello che serve. Sarò contento di contribuire anch'io, con qualche cosa che vi dirò adesso. una nota personale. Prima qualcuno ce l'aveva con chi si siede a quel tavolino. Sapete cosa mi dispiace sia accaduto al Senato, come alla Camera, dopo il Covid-19? Non abbiamo più gli stenografi in Aula. Gli stenografi raccoglievano tutto quello che accadeva in Aula. Quindi, gli insulti, le frasi, ogni sospiro, ogni respiro, ogni applauso veniva descritto, decrittato e ad ognuno veniva attribuita ogni parola. Tutto questo non succede più. Io sono andato a leggere il Resoconto in corso di seduta: non si capisce niente. che voi capite tante cose, avete capito anche che io non dico menzogne di alcun tipo e ascoltate un attimo anche quello che ho da dirvi. La mia premessa è questa: sì, prima ero pesantemente irritato. E lo sapete perché ero irritato? Ero irritato dallo strabismo della Presidenza di turno, che non si era resa conto, per una decina di minuti, che il sempre impeccabile e professorale senatore Boccia era rimasto ostentatamente seduto lassù, con le terga da queste parti, sul tavolino, senza che nessuno osasse richiamarlo. che ogni tanto sono fumantino, alzo la voce e di richiami ne becco parecchi, penso che il Capogruppo dovrebbe comportarsi in modo conveniente e non sconveniente. Io vengo richiamato per tante cose da questi *arbitri elegantiarum* - toglietevi la giacca - e vi dirò che cosa è accaduto. Aveva appena finito di parlare il senatore Licheri, che è bravo nella sua oratoria, spesso provocatorio, ma questo fa parte del contesto: sono uso a queste cose. Lo so, è logico che ci si possa dire e raccontare tante cose. Però, dopo giorni che ti senti dare del ladro di democrazia, dello sciatto, del barbaro, del vergognoso, dell'imbecille, dell'asservito, dell'ignorante, del totalitarista, del *quaquaraquà*, del mezz'uomo, si alza anche il livello. livello. Mentre aveva appena iniziato a parlare il senatore De Cristofaro e da questa parte si rumoreggiava, perché continuava l'eco di quello che era accaduto prima, a dirigere con ampi gesti delle braccia e delle mani, lo sfottò a questi banchi

Non dico chi lo ha fatto: *nomina sunt odiosa*, però questo è accaduto. Non sempre sono pensoso, calmo, nostalgico, lacrimevole. Divento anche fumantino, come si nota. E molto fumantino sono sceso nell'emiciclo, dove mi ha intercettato l'amico De Poli,

a leggere i giornali *on line*, io scopro di avere fatto una rissa col senatore Croatti: non me ne ero accorto, personalmente*.

e, visto che abbiamo il VAR, sarà ancora più facile accertare tutto questo. Però, uno: non ho aggredito nessuno, anche perché, per aver fatto un'aggressione, ci dev'essere un aggredito. Dovete dirmi chi è l'aggredito; non ho capito, non me ne sono accorto: forse De Poli. Non sono un bugiardo e uso guardare la gente negli occhi. Non sono un vile, perché vile è chi lancia il sasso e poi nasconde il braccio. Quindi, a quelli che mi insegnano l'educazione, consiglio di rimettersi la giacca. A quelli che vorrebbero che fossi cacciato, mi dispiace: *hic manebimus optime*.